Fratelli d'Italia ha presentato questa mozione per portare nella discussione parlamentare e all'attenzione del Governo il tema centrale del settore siderurgico, che è considerato strategico e su cui è costruita la competitività di tutto il sistema industriale italiano. L'acciaio in Italia non solo ha una lunga tradizione, ma rappresenta l'eccellenza e la flessibilità tipiche del *made in Italy*. Per queste ragioni, la siderurgia italiana mantiene un ruolo di primo piano non solo nel contesto economico nazionale, ma anche in quello europeo e globale, essendo la seconda potenza produttiva a livello continentale, dopo la Germania, e la decima a livello mondiale. In Italia ci sono quattro siti di rilevanza nazionale: Trieste, Piombino, Terni e Taranto, tutti coinvolti in opere di ristrutturazione tecnologica, industriale e ambientale. A parte il sito friulano, gli altri tre lo sono con *partnership* straniere, con poca predisposizione alla tutela degli interessi nazionali. Le gravi crisi esplose negli ultimi anni all'Ilva di Taranto, alla Lucchini di Piombino e alla AST di Terni mettono in discussione la vitalità dell'intero settore della siderurgia, esponendo l'intera economia italiana a un rischio di sistema di enorme portata, che non sembra essere preso nella giusta considerazione dal Governo. Nel caso di Terni, la ThyssenKrupp ha espresso l'intenzione di voler uscire dal settore; nel caso di Taranto, ArcelorMittal ha dichiarato l'impossibilità di eseguire non solo il piano ambientale, ma anche l'attività industriale, dopo provvedimenti che hanno tolto lo scudo penale, invocando persino l'esercizio del diritto di recesso. Nel caso di Piombino, la JSW ha atteso fino all'ultimo momento possibile la presentazione del proprio piano, alimentando le tesi di coloro che, fin dall'inizio, hanno sostenuto che gli investimenti della multinazionale indiana avessero l'obiettivo di eliminare un concorrente più che quello di aumentare la loro presenza in Europa. situazione è ancora più critica se si considera che proprietà e *management* hanno due direzioni e obiettivi divergenti: da una parte, si chiedono investimenti di Stato; dall'altra, si parla di

la realizzazione di un piano strategico per la siderurgia che definisca nel dettaglio il fabbisogno di acciaio del nostro Paese e le condizioni di mercato su cui i produttori devono muoversi, prevedendo la ristrutturazione del comparto in un'ottica di maggiore competitività. luogo, con riferimento al sito di Taranto, chiediamo un elemento molto importante, ossia di accelerare l'attuazione del piano ambientale e del piano industriale, assicurandosi che ArcelorMittal rispetti gli impegni assunti affinché lo stabilimento *ex* Ilva possa davvero diventare il più grande polo siderurgico *green* d'Europa. Qui voglio specificare un altro passaggio per noi importante, forse non ben compreso, ma fondamentale: chiediamo anche di ricostituire lo scudo penale per il periodo di attuazione del piano, alla luce degli sviluppi giudiziari in corso a Taranto, per evitare che le gravissime responsabilità del passato - che, lo sottolineo, vanno sicuramente accertate e perseguite con la massima severità, sul piano sia penale sia civile - non ricadano però anche su chi oggi si impegna invece per la salvaguardia della salute e dell'ambiente, operando la necessaria riconversione industriale e il risanamento ambientale. Chiediamo di confermare il programma di investimento previsto per la AST di Terni nel corrente anno 2021 e di valutare l'impegno di Cassa depositi e prestiti o di Invitalia, ove fosse richiesto. Chiediamo di convocare tempestivamente un tavolo per valutare la fondatezza del piano industriale presentato dall'acciaieria di Piombino, che, come emerge dalle poche notizie trapelate, appare del tutto generico e privo di garanzia. Chiediamo, cosa molto importante e fondamentale, di prorogare l'estensione, anche al settore siderurgico, del *golden power*, con l'obiettivo di garantire livelli occupazionali e la produttività, non essendo stata prorogata dal precedente Governo. ultimo punto, chiediamo di utilizzare anche le risorse del *recovery fund* e il ruolo propositivo di Cassa depositi e prestiti e Invitalia al fine di riaffermare il ruolo strategico della siderurgia italiana. Signor Presidente, concludo

ringraziare il collega Urso, che questa mattina ci dà modo di discutere di un tema assolutamente necessario, indispensabile e strategico per il nostro interesse nazionale. Nei "rari sprazzi di lucidità", il collega Urso riesce a

e posso trasmettere il grande senso di impotenza delle istituzioni locali nei confronti di tematiche che volano alte sulla testa del Governo regionale, tanto da non riuscire neanche ad afferrarne i momenti salienti. Lo stesso potrebbe accadere nel momento in cui lo Stato si trova a interfacciarsi con processi che rischiano di vederlo come banale spettatore: è del tutto evidente che in questo tipo di trattative deve avere strumenti utili a far a far valere la sua presenza e l'intera filiera delle istituzioni (ivi comprese quelle regionali) ha il dovere e il diritto di partecipare a tali processi, con la possibilità di incidere ed essere protagonista al fine di vigilare e controllare. Certamente il mercato risponde a logiche che a volte devono essere integrate da un'azione politica delle istituzioni di presenza sul territorio, in termini di controllo del rispetto dei parametri ambientali, ambientali, del mantenimento dei livelli occupazionali e dei programmi di investimento presentati dalle grandi aziende multinazionali, che a volte invece travalicano l'esigenza di confrontarsi con le istituzioni. Rispetto a tutto ciò la mozione pone puntelli precisi, quindi ribadisce la necessità di un piano siderurgico nazionale, di agire con di agire con lo strumento della *golden share,* che dev'essere evidentemente trasformata in legge, visto che è scaduta quella che era stata posta. In alternativa, si deve anche considerare una vecchia proposta di Fratelli d'Italia, espressa anche sul territorio dalla nostra presidente Giorgia Meloni, cioè la possibilità di acquisto da parte di Invitalia o di Cassa depositi e prestiti di una piccola quota tale per cui lo Stato possa almeno vigilare sull'andamento di una trattativa che non può essere lasciata semplicemente alle dinamiche di mercato, cioè alla domanda e all'offerta.

alla ArcelorMittal di Taranto un lavoratore, Riccardo Cristello, è stato licenziato perché aveva pubblicato su Facebook un *post* che invitava a seguire una *fiction* televisiva riguardante il tema dell'inquinamento di una città non meglio identificata, da parte di una fabbrica non meglio identificata. Gli è bastato questo per essere licenziato. Imporre ai lavoratori di nascondere le proprie opinioni e non manifestarle è fascismo aziendale. Un licenziamento così ingiusto e abnorme è il segno inequivocabile che in questo frangente di crisi, non solo sanitaria ed economica, ma anche sociale e democratica, i più forti si sentono invulnerabili e contano sull'impunità nelle prepotenze sui più deboli, perché l'aura che emana da questo Governo è proprio quella della predominanza del grande sul piccolo, del forte sul debole e del capitale sul lavoro. La razza padrona fiuta subito l'aria, stringe la morsa e comprime diritti che fino a poco tempo fa sarebbero stati inviolabili. Per contrastare questa deriva, domani sarò a manifestare con l'Unione

Per produrre senza inquinare occorre investire e cambiare tecnologie e mentalità. Certamente costa molto, ma è su questo, sulla bonifica di Taranto e delle tante realtà simili, che occorre spendere i soldi del piano di ripartenza, non in armi o in ponti sullo stretto di Messina. però non ascoltate, siete sordi e ciechi. Il piano acciaio noi ce l'abbiamo ed è una ricerca e produzione di nuova generazione, costi quel che costi, liberandoci delle vecchie scorie con tutti i soldi che sono necessari.

Signor Presidente, stamattina, spero non nella distrazione generale, si discute uno dei temi più significativi per il Paese, perché parliamo non

hanno perso il lavoro). Si tratta di un elemento importante, ma altrettanto importante e significativa è la centralità che l'Italia vuole avere nel sistema europeo e internazionale relativamente all'acciaio. venduto, o svenduto - non lo so, cercate voi di meglio interpretare quello che è accaduto - a gruppi stranieri. Ciò ha riguardato Taranto e Piombino, con ArcelorMittal o Jindal. I nostri impianti,

dell'acciaieria piombinese. Ci sono 1.800 persone che non sanno quale sarà il loro destino, una comunità intera che guarda a quell'azienda come possibile ipotesi di sviluppo e un Paese e una Regione che fanno conto su quell'attività, fino ad oggi ci siamo occupati poco e male. La prospettiva è allora quella contenuta in un fantomatico piano industriale che ancora non abbiamo visto.

C'è l'ipotesi di una partecipazione di Invitalia all'azienda piombinese, che però è ancora per aria, perché giustamente le prospettive legate al piano industriale sono evanescenti. Sembra quasi che ci sia la volontà di far chiudere l'azienda e trasferire la produzione altrove, probabilmente perché produrre acciaio nel mondo costa molto meno rispetto a quello che costa nel nostro Paese. Abbiamo sottoscritto però un accordo di qualche miliardo tra Ferrovie dello Stato e Piombino per la realizzazione delle rotaie, senza di fatto un oggettivo vincolo di permanenza sul posto di questa commessa, che domani l'imprenditore indiano potrebbe prendersi e trasferire nei propri impianti indiani, abbandonando la città di Piombino, senza guardare alla prospettiva del futuro dell'azienda, delle persone, delle famiglie, dell'economia italiana e della centralità del Paese all'interno dell'economia dell'acciaio.

Vogliamo capire l'esercizio del *golden power,* perché probabilmente non c'è stato, e comprendere a posteriori l'opportunità di tanti imprenditori dell'acciaio italiano ancora oggi disposti a partecipare quell'azienda, rendendola nuovamente nazionale e portando avanti la prospettiva dell'acciaio italiano nel mondo, con una visione occupazionale di rilievo, per la centralità del nostro Paese in quello scenario, che ormai abbiamo abbandonato da troppo tempo. *(Applausi)*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Urso per averci dato oggi l'opportunità di riparlare in Aula di un tema così importante, così come ringrazio il Governo, che da quando si è insediato sta lavorando alacremente per far ripartire l'Italia, dopo un lungo anno di *lockdown* il momento di ricostruire il Paese, non sono con le infrastrutture, il turismo, l'agricoltura e lo snellimento della burocrazia, ma anche con un piano industriale che faccia tornare l'Italia ad essere protagonista in Europa. L'Italia ha bisogno di un'industria sana, che rispetti il diritto al lavoro, il diritto all'ambiente e il diritto alla salute. È necessario un piano industriale diverso e aggiornato, perché l'obbligo è quello di far lavorare le aziende. Il settore siderurgico costituisce un elemento fondamentale delle attività produttive e rientra in questo piano. Noi della Lega siamo consapevoli di quanto sia importante produrre acciaio in Italia, ma siamo anche consapevoli di quanto sia importante tutelare la salute. Per questo motivo, il problema dev'essere affrontato a tutto tondo e, chiaramente, non solo con una mozione. Non è infatti un caso che uno dei primi *dossier* su cui il ministro Giorgetti ha iniziato a lavorare sia stato quello allo stabilimento di ArcelorMittal, incontrando da subito il commissario dell'*ex* Ilva, il governatore della Puglia, Emiliano, il sindaco di Taranto, i sindacati e Confindustria Puglia. Inoltre, egli ha proposto di effettuare una verifica di fattibilità tecnico-economica, per puntare a una riconversione energetica del sito dell'ex Ilva. Tale possibilità è prevista nel quadro del Next generation EU, con la riconversione energetica di questi impianti, per produrre acciaio con bassissimo impatto Taranto vive momenti di grandi tensioni sociali, legati alle incertezze per il mantenimento dei livelli occupazionali, da un lato, e alle legittime aspettative di tutela della salute, dall'altro. È il momento di intervenire in favore di questa città, dei suoi abitanti e di questa Regione, non concentrandosi più sui racconti di un domani non realizzabile. Corre l'obbligo di dare finalmente concretezza a scelte di buonsenso, capaci di infondere fiducia anche nelle aziende dell'indotto, che, da più parti e a più riprese, chiedono interventi urgenti in favore della produttività. È inderogabile una significativa accelerazione, sia sul piano ambientale, sia sul piano industriale. Vigileremo affinché ArcelorMittal rispetti tutti gli impegni assunti con il Governo: lo dobbiamo a un pezzo importante della storia industriale italiana e ai tanti lavoratori che di questa storia fanno parte. L'ambizione è quella di trasformare l'attuale sito produttivo

di questo eccezionale progetto. Le risorse messe a disposizione dell'Europa attraverso il *recovery fund,* il decisivo intervento della Cassa depositi e prestiti e i 400 milioni di euro di Invitalia devono essere gli strumenti attraverso i quali costruire solide basi, sulle quali poter riaffermare il ruolo strategico della nostra siderurgia in Italia Per far questo è necessario evitare che le pesanti e gravi responsabilità del passato ricadano su chi intende impegnarsi attivamente per salvaguardare l'ambiente e la salute, garantendo il risarcimento dei luoghi e la riconversione industriale, nonché prorogare l'estensione del *golden power*, unico argine in grado di garantire gli attuali livelli occupazionali del settore siderurgico. Signor Presidente, l'ingresso dello Stato non servirà per fare la solita politica assistenziale, perché il Sud non ha bisogno di questo, ma per far crescere e sviluppare non solo

rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, la mozione sottoposta alla valutazione dell'Assemblea pone importanti questioni in merito al punto di svolta in cui si trova il settore siderurgico nazionale, sul piano economico, della salute pubblica e ambientale. In un contesto internazionale sempre più agguerrito, la situazione in Italia sta peggiorando di anno in anno, con decine di migliaia di lavoratori che rischiano il proprio posto di lavoro. Non possiamo restare a guardare che uno dei punti di forza della nostra industria perda un pezzo alla volta. Occorre con urgenza la formulazione di un piano nazionale strategico per la siderurgia da parte del Governo, che prenda in considerazione tutte le attuali criticità per proteggere questa importante parte del PIL nazionale. È un piano indispensabile, poiché, oltre alla salvaguardia dei posti di lavoro, dobbiamo anche rispondere alle istanze di salvaguardia della salute dei cittadini nei territori in cui sono presenti stabilimenti siderurgici, in cui i dati statistici di incidenza delle patologie tumorali sono molto superiori alla media nazionale. Il primo pensiero va alla drammatica situazione di Taranto, dove per decenni la salute pubblica è stata sacrificata sull'altare del profitto, a tutto vantaggio di pochi proprietari, favoriti da una classe politica asservita al al loro potere economico, come le indagini giudiziarie hanno portato alla luce. Da cittadina umbra non posso non menzionare le acciaierie di Terni, all'interno di un'area classificata come sito di interesse nazionale (SIN), ovvero altamente inquinata e da bonificare, a cui si aggiunge la presenza di due inceneritori, che complica ulteriormente la criticità ambientale della conca ternana. Purtroppo, devo notare l'atteggiamento dell'amministrazione regionale, che ha sostanzialmente fermato il pieno funzionamento del registro dei tumori, importantissimo strumento per avere l'incidenza delle patologie tumorali nella popolazione in un'area geografica. Non possiamo scordarci dell'ambiente. Ecco perché serve essere consapevoli del fatto che le acciaierie emettono una grande quantità di CO2. I dati del 2018 del *report* «Acciaio sostenibile - Indicatori 2018 e iniziative» rivelano che, per ciascuna tonnellata di acciaio, sono state prodotte in media 1,83 tonnellate di CO2. quindi arrivato il momento di fare scelte coraggiose, imprescindibili per il futuro di tutti noi e delle generazioni che verranno, e orientare le acciaierie di cui non possiamo fare a meno - verso la necessaria transizione ecologica, con aziende responsabili, che mettano in campo una reale visione a medio e lungo termine, sia dal punto di vista industriale, sia per la conversione *green* del settore. Questo è fondamentale anche per una città come Terni, dove i lavoratori attendono ancora risposte chiare. Il dovere costituzionalmente riconosciuto di proteggere la salute dei cittadini è direttamente collegato alla salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso, a partire dall'emissione nell'aria e nell'acqua, tenendo presenti le disposizioni dell'Unione europea, che prevedono il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 (quanto previsto nel *green deal* europeo). Da legislatori e decisori siamo chiamati a una grande responsabilità, per iniziare a guardare a questo settore con un'ottica diversa. Dobbiamo proteggere l'industria siderurgica nazionale, ma dobbiamo spingere le imprese a investimenti in nuove tecnologie e impianti che permettano di produrre acciaio con il minore inquinamento possibile nel ciclo di produzione delle scorie residue nelle emissioni in atmosfera; è fondamentale però che la stessa industria si attivi verso lo stesso obiettivo. Il *World steel association* (cioè tutte le industrie dell'acciaio nel 2018) ha infatti sottoscritto il *Sustainable development charter of the world* *steel industry*, ma ad oggi questo cambiamento non sembra ancora attuato. La tecnologia ci viene in aiuto. Ecco perché serve passare velocemente alla decarbonizzazione del settore. Dobbiamo promuovere l'economia circolare al riuso del materiale in quanto al 100 per cento riciclabile e adottare soluzioni per il riciclo delle scorie attraverso la creazione di nuovi materiali. Anche per questi motivi, è stato pensato il nuovo Ministero della transizione ecologica che, in sinergia con altri Ministeri, sarà chiamato a svolgere un ruolo importantissimo per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e neutralità climatica previsti dai sopra richiamati piani europei e normative collegate. *(Applausi).*

a nome del Governo ringrazio i proponenti la mozione, anche per la disponibilità a trovare una convergenza rispetto al

l'insieme del sistema dell'acciaio. Vorrei ricordare che Ilva e Piombino sono questioni nazionali relative a un certo tipo di acciaio, Terni è un'altra questione. È come confrontare la viscosa e la vicuña, parlando di tessile. Vi è, quindi, la necessità di salvaguardare tutta la filiera e naturalmente di trovare le soluzioni opportune, nei primi due casi di ristrutturazione, nel terzo caso di individuazione di un nuovo socio rispetto alle finalità dell'attuale proprietà.

l'attenzione e il potenziale deterrente, rispetto ad alcune situazioni, dell'utilizzo degli strumenti giuridici a disposizione. Ringrazio i proponenti e credo che

Sottosegretario per le considerazioni poc'anzi espresse e per aver contribuito, a nome del Governo, alla stesura di un ordine del giorno che va nella direzione

produrre una discussione sul tema della siderurgia, che caratterizza gran parte dello sviluppo del nostro Paese, per la centralità che il settore siderurgico

a un dibattito di questa natura. Noi abbiamo il dovere, come Parlamento, di contribuire a dare una direzione e una spinta al Governo sul tema della siderurgia. Sappiamo bene che il settore siderurgico è una ricchezza straordinaria, non solo del nostro Paese ma di tutta l'Europa; una ricchezza occupazionale stimabile in 70.000 addetti, sia nel settore diretto che in quello indiretto, il cosiddetto indotto. un settore che caratterizza la vita del nostro Paese e dell'Europa nell'ambito delle costruzioni, della meccanica, dell'*automotive*, degli elettrodomestici. Sul nostro territorio riconosciamo la centralità di tre siti straordinariamente importanti (Taranto, Piombino, Terni), caratterizzati in questa fase da problematiche piuttosto rilevanti, su cui torno tra poco.

ormai imperante bisogna assolutamente rilanciare un piano di industria sostenibile, come veniva detto prima e come e come si dice nella riflessione che l'ordine del giorno pone al Parlamento. Innanzitutto ciò dovrà essere fatto puntando sulle risorse del *recovery plan.* In questo senso, abbiamo visto come quel piano può avere una grande centralità, soprattutto per quanto riguarda le risorse da destinare a tutto il processo di transizione

all'indomani della crisi che c'è stata con ArcelorMittal relativamente a problemi sorti nella gestione del sito e alle questioni concernenti la cancellazione dello scudo penale.

nessuno si può sottrarre, inclusi il Governo e l'Unione europea. Abbiamo il tema di Piombino, un altro dei siti di grande valore strategico per questo Paese, caratterizzato dalla presenza dell'azionariato Jindal, che in questi anni non ha in questi anni non ha dato l'impressione di voler spingere il polo industriale di Piombino verso un rinnovato sviluppo. È sembrato quasi più un tentativo di limitare la concorrenza di questo stabilimento nel panorama mondiale. Di fatto, Jindal, comprandolo, lo ha sottratto alla concorrenza verso le proprie produzioni con altri siti mondiali. Appare più questo il problema di Piombino piuttosto che questioni che attengono alle valutazioni che invece sono da fare sullo sviluppo di un sito così importante. Da ultima, ma non per importanza, vi è la questione dell'acciaieria ternana, che avverto personalmente

L'acciaieria ternana ormai da molti anni è sottoposta a *stress* - soprattutto i lavoratori - per i continui cambi di assetto societario. L'anno scorso la proprietà attuale, ThyssenKrupp, che l'aveva riacquistata per motivi attinenti all'intervento dell'Europa in tema di *antitrust* dai finlandesi di Outokumpu, ha annunciato la dismissione dell'*inox* (ovvero della produzione di acciaio su Terni) e non

si pone una riflessione che deve coinvolgere necessariamente le istituzioni europee perché, come l'Europa intervenne per bloccare la cessione ai finlandesi di Outokumpu dell'acciaieria ternana per questioni relative alla concentrazione di azionariato all'*Antitrust*,

possano essere sostenute anche in campo europeo. Noi pensiamo di no e quindi il tema deve essere sicuramente posto all'attenzione del commissario europeo per la concorrenza e il Governo deve spingere in questa direzione. Sostanzialmente

tavoli europei per la definizione di una politica industriale comune. Questo sicuramente è il primo punto e il più rilevante. Siamo convinti che sia importante adottare un nuovo piano di azione che dia una visione di lungo periodo per quanto riguarda la politica siderurgica in Italia. Pensiamo però che sia fondamentale fare questo attraverso un passaggio che poi è indicato bene negli impegni per il Governo: la soluzione di tutti i tavoli di crisi. Le situazioni dei tre principali stabilimenti

e linfa ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché sono quelli che potranno garantire i necessari passaggi di riconversione ecologica verso una produzione industriale sostenibile, che può dare nuova linfa alla siderurgia italiana.

Fratelli d'Italia ha presentato la mozione che ha dato occasione al Parlamento e a quest'Aula di discutere di una questione fondamentale per l'assetto della politica industriale, sociale e ambientale di questo Paese. L'ha fatto con convinzione, in un momento particolarmente delicato per il settore, come dimostra il fatto che il Governo ha convocato i sindacati per domani e il fatto che c'è grande agitazione nelle sedi e negli stabilimenti del settore siderurgico italiano, a Taranto, a Genova, a Piombino, a Terni. Ma, soprattutto, c'è tanta agitazione e preoccupazione nei settori che utilizzano l'acciaio italiano. L'altro giorno un quotidiano importante e certamente non vicino a noi ipotizzava che ci fosse una strategia internazionale di cui gli stabilimenti italiani fossero oggetto per aumentare il prezzo dell'acciaio in Europa, come dimostra l'andamento del prezzo dell'acciaio di questi giorni, facendo uscire fuori dalla competizione proprio gli utilizzatori del settore in Italia, che sono gran parte della nostra industria ferroviaria, automobilistica, degli elettrodomestici e quant'altro. Ringraziamo il Governo e le altre forze politiche per aver compreso l'importanza della questione e aver convenuto nella realizzazione di un documento finale unitario: un ordine del giorno che recepisce gran parte delle nostre indicazioni,

Lo ringraziamo quindi nel merito, perché stiamo parlando di una cosa fondamentale per l'economia italiana, ma lo ringraziamo anche nel metodo, è quello che noi vogliamo attuare in questa fase della legislatura, come ha detto sin dall'inizio Giorgia Meloni nel motivare la nostra posizione rispetto al Governo, quella di un'opposizione patriottica e quindi costruttiva e collaborativa, tanto più quando si tratta di argomenti e di decisioni che vanno prese oggi per non pregiudicare il futuro del Paese, anzi per costruirlo insieme. Poi, quando noi saremo noi saremo al Governo, ci ritroveremo in una condizione migliore, se abbiamo collaborato insieme in Parlamento a indicare le vie giuste su cui il Paese si deve indirizzare. Nel merito si tratta quindi di un argomento strategico su cui lo Stato - l'abbiamo detto - deve intervenire non come Stato interventista, ma come Stato stratega nel delineare quale sia il fabbisogno dell'acciaio in Italia, per sostenere la propria industria nel delineare quali devono essere gli attori. Tutti siamo infatti consapevoli che gli stabilimenti di Terni, Piombino e Taranto, oggi in mano ad aziende straniere, nei prossimi anni vedranno altri attori, perché siamo consapevoli che costoro stanno uscendo da tali aziende per motivi diversi: TyssenKrupp per una strategia internazionale abbandona l'acciaio; Piombino perché di fatto non vediamo un impegno reale, come era stato assicurato dall'azienda indiana che aveva acquisito lo stabilimento; l'Ilva perché voi che avete governato in questi anni siete più consapevoli di noi di quali fossero i reali intendimenti del soggetto che è intervenuto e di come si possa operare. Però oggi si può fare qualcosa, anzi si può fare molto, anzi si può fare tutto, oggi più che mai, utilizzando proprio le risorse del *recovery fund*, e non solo

automobilistica e manifatturiera italiana, che è la principale voce delle nostre esportazioni proprio perché ha potuto usufruire in questi anni di un prezzo competitivo e di un acciaio che è migliore di quello prodotto in altri stabilimenti europei. Lo sanno tutti, a cominciare dai militari europei che operano all'estero e che, quando si ritrovano in un mezzo protetto dall'acciaio italiano *(Applausi)*, sanno bene che quell'acciaio protegge meglio di quello prodotto in Francia. Ecco perché noi sappiamo quanto fondamentale sia e oggi delineiamo una strategia che prevede un piano per la siderurgia, una logica unitaria (non lo spezzettamento tra i tre tavoli di Piombino, dell'Ilva e di Terni, ma una logica complessiva), e nel contempo la riproposizione del *golden power*, che era stato inserito con un emendamento nostro e credo della Lega alla Camera nel decreto-legge liquidità dell'aprile scorso,

con un documento unitario, ben consapevole che su questo il Parlamento non si deve dividere. Noi per primi non intendiamo dividere le altre forze politiche, nemmeno quelle della maggioranza: il nostro intendimento era unire,

risolvere; lo dobbiamo ai tanti lavoratori e anche a coloro che hanno pagato in termini sanitari, talvolta con la vita, l'inquinamento della siderurgia di Taranto. Noi dobbiamo risolvere il problema e non meramente denunciarlo, né tantomeno dobbiamo lasciare che sia la magistratura a dettare le regole della politica industriale e ambientale in questo Paese. È la politica e il Parlamento che lo debbono fare, e in questo la magistratura non può, a nostro avviso, svolgere un ruolo di supplenza del Parlamento; ovviamente deve indagare e colpire in maniera chiara i colpevoli. Per questo l'estensione del *golden power* è importante: in un momento in cui probabilmente i soggetti stranieri intendono uscire dal Paese, dobbiamo indirizzare chi ne prenderà il posto per costruire una siderurgia che si regga sulla strategia dello Stato, anche sull'intervento pubblico - che sia Invitalia o Cassa depositi e prestiti - che può essere importante per il momento di supplenza per condizionare poi le scelte e indirizzarle verso l'interesse nazionale nel settore. Ma cito anche i privati italiani, perché abbiamo un'industria siderurgica e un *management* di prim'ordine in Italia, che va coinvolto nella logica di un piano nazionale e nella gestione industriale di queste aziende: si può fare se insieme costruiamo una politica nazionale che sia di esempio anche su altri settori. In queste ore alla Camera si sta discutendo di Borsa italiana. Anche in questo caso, essendo un settore fondamentale, Giorgia Meloni ha voluto che ci fosse un dibattito aperto in Parlamento, con delle convergenze tra maggioranza e opposizione, nell'interesse supremo del Paese, su decisioni che - prese oggi - possono pregiudicare o salvare e costruire l'interesse nazionale dei prossimi anni. Su questa linea proseguiremo anche sulle altre questioni fondamentali, con la consapevolezza che in questo scorcio finale di legislatura dobbiamo proporre e costruire un rapporto corretto con la maggioranza e con il Governo, nella convinzione che in questo campo è sempre più necessario condividere le scelte.

perché non si può cambiare una politica sulla siderurgia, sull'acciaio o sulla finanza allo stormir dei Governi. Queste sono scelte nazionali

e in tutto il mondo. Il Covid ci ha fatto dire spesso che niente sarà come prima, ma questo dipende essenzialmente dalla nostra capacità di guardare in modo diverso alla realtà, di proiettarla nel futuro in un modo più consapevole rispetto a tanti temi che oggi abbiamo scoperto essere essenziali, come la sostenibilità ambientale. L'Europa si è data, con grande coraggio, degli obiettivi ambiziosi di cambiamento; il *recovery plan* non è soltanto una grande iniezione di risorse, ma è un percorso di trasformazione dell'economia, del sistema produttivo dell'Europa e quando si fanno queste valutazioni, credo che debbano essere individuati i settori strategici. Questo è il tema fondamentale. Oggi, con la discussione che abbiamo affrontato, soprattutto con l'ordine del giorno che ci apprestiamo a votare unitariamente, dichiariamo di avere questa consapevolezza. È vero che ci sono delle crisi aziendali e ci sono tavoli di crisi che vanno assolutamente risolti, ma non è una risposta emergenziale quella che vogliamo dare, bensì una risposta che contenga una progettualità, che dia un senso e un percorso complessivo al nostro Paese, in un quadro di strategie europee che dobbiamo assolutamente richiamare e cercare di ottenere. ottenere. Le soluzioni rispetto a questi ambiti strategici non stanno più soltanto nella ricerca delle condizioni che localmente possono determinare una via d'uscita, vanno ricercate e trovate in una prospettiva che all'intero settore siderurgico riconosca un ruolo fondamentale. Il settore siderurgico per l'Europa è assolutamente decisivo proprio perché sono venute a crearsi delle nuove condizioni, ad esempio l'industria automobilistica ha fatto dei cambiamenti, delle fusioni, ha fatto dei passi di avanzamento importanti, tutto quello che ne consegue. Le filiere legate all'acciaio sono assolutamente importanti per il nostro continente e sono legate, come è stato anche detto, a produzioni di grande qualità. È chiaro che oggi nel mondo ci sono delle grandi disomogeneità dal punto di vista produttivo. Non è un'eresia parlare di *dumping*

a tali disomogeneità, noi dobbiamo fare delle scelte strategiche come Unione europea e l'acciaio sta al centro. Non può arrivare un'altra pandemia e colpire un'Europa che ancora non sa quali sono i settori strategici sui quali dobbiamo aver fatto un percorso di messa in sicurezza. L'Europa non può rischiare di trovarsi sguarnita perché ci sono dinamiche che l'hanno portata ad affidare ad altri soggetti il futuro di determinati settori sul territorio dell'Unione europea.

per il Governo a lavorare in questa direzione, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale ed europeo. se non facciamo crescere questa consapevolezza tra tutti i Paesi e continuiamo a pensare che la soluzione di certi temi stia prima di tutto nel nostro Paese e non sia

L'Europa ha fatto un salto di qualità dal punto di vista della consapevolezza di fronte a questa pandemia. Deve ripetere, secondo me, questo questo salto di qualità in ogni settore che dal punto di vista strategico rappresenta un'infrastruttura fondamentale dell'economia del continente. Questo è un Questo è un punto d'inizio. Normalmente le mozioni cercano di essere precise e di dare degli impegni precisi. possono sembrare un po' sfumati, ma in realtà sono punti decisivi, perché rappresentano gli obiettivi sui quali occorre lavorare in modo determinato da subito, proprio perché

tempestività. Quindi, queste riflessioni strategiche vanno fatte in fretta e vanno condivise a livello di Governo, ma soprattutto a livello di Parlamento, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate: il sistema produttivo, i lavoratori, i sindacati e le popolazioni sulle quali insistono questi grandi impianti. I territori sono assolutamente protagonisti in questo tipo di percorso. Se questo ordine

potremmo valutare ulteriormente l'approfondimento di questi temi. Abbiamo un affare assegnato sulle aree di crisi complessa e sappiamo che diciassette aree di crisi complessa ci sono proprio quelle interessate dagli impianti siderurgici. Al di là dei temi specifici di ciascun sito, credo che il Governo e il Parlamento dovranno lavorare per affrontare i temi di fondo che sono emersi da questa discussione. Certamente, tutti i settori strategici hanno necessità di scelte significative della parte pubblica, da parte del Governo. Ci sono delle trasformazioni che, se le lasciamo al mercato, seguono dinamiche che non danno le risposte che cerchiamo. Quindi, l'indicazione emersa di valutare l'estensione del *golden power* al settore siderurgico è assolutamente decisiva. Noi non possiamo cadere in questa contraddizione dove, da una parte, diciamo

un tema importante, da continuare a sviscerare e approfondire, ma poi, con il Governo, dovremo riuscire ad approdare a scelte precise, incisive e decisive.

che hanno promosso una discussione così importante su un settore strategico come quello siderurgico. Grazie anche per l'impegno a contenere, nei limiti del possibile e per quanto si possa fare, questa discussione dentro un ordine del giorno unitario, condiviso trasversalmente dalle forze politiche.

costruita attraverso linee strategiche condivise trasversalmente dalle forze politiche e dall'intero Paese. Dentro questa cornice, naturalmente, rientra la legittimità, da parte delle forze politiche, di dividersi in relazione alle proprie sensibilità e al proprio sguardo sul mondo. il fatto di costruire un ordine del giorno che ha queste caratteristiche mi conforta, perché vuol dire rimettere al centro la discussione sulla politica industriale e porci la domanda delle domande, cioè che cosa vuole diventare l'Italia nei prossimi venti, trenta anni. Dobbiamo tornare all'ambizione di riformulare domande che abbiamo smesso di farci da molto tempo. Aggiungo soltanto poche considerazioni che tra l'altro sono sottolineature che riprendono alcune riflessioni già sviluppate dai colleghi che mi hanno preceduto. La prima: Ilva, Lucchini, AST sono naturalmente e tecnicamente vicende trattate in tavoli di crisi industriali, non possono essere considerati semplici tavoli di crisi industriali, tanto più se li trattiamo in modo separato, in assenza di una cornice unificante, di un filo conduttore che li tenga insieme, se non usciamo dalla logica emergenziale, se non individuiamo un piano strategico complessivo, se non pensiamo, come invece dovremmo, che tali vicende hanno bisogno di una trattazione unificante. Questo perché c'è un tema che le attraversa, che riguarda l'innovazione tecnologica, riguarda la capacità di aumentare e di far crescere la produttività, che riguarda, per esempio, la possibilità di aumentare la capacità negoziale in relazione alla trattativa sui costi energetici. Stiamo parlando di programmazione che è la premessa per costruire un piano di investimenti sul settore tutto, nella sua complessità e nelle sue articolazioni. Per questo, l'indicazione individuata all'interno dell'ordine del giorno è un'indicazione giusta, che è di metodo, ma anche di sostanza. Non lo dico perché ho sentito echeggiare alcuni richiami patriottici e autarchici: non abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di difendere l'interesse nazionale, ma con la consapevolezza che la scala su cui riportare questa discussione è quantomeno europea. Anche in questo senso, l'ordine del giorno dà un contributo significativo proprio perché sottolinea il tema

abbiamo ragionato di operatori propensi più a operare una sorta di disimpegno sugli investimenti, che ad attivarsi realmente per far ripartire l'attività industriale dei siti di cui stiamo discutendo. Ciò vale sia per Terni (che è stata citata e dove la ThyssenKrupp ha espresso l'intenzione di uscire dal settore), che per ArcelorMittal,

agli indiani di Piombino (lo dico non in senso dispregiativo, ma a sottolineare la nazionalità della multinazionale), che hanno atteso hanno atteso fino all'ultimo minuto per presentare il piano, sostanzialmente dichiarando in modo piuttosto esplicito almeno così la si deve leggere - l'intenzione più di eliminare un concorrente, che di mettersi in corsa attivamente per far ripartire la produzione industriale. Non so se si possa definire così, ma io mi permetto di chiamarlo

Si tratta di un punto importante che ha a che fare con la funzione e il ruolo dello Stato in un settore che non può essere considerato uno come come tanti, perché rappresenta l'ossatura e la spina dorsale di un bel pezzo dell'industria manifatturiera del Paese. Infine, la siderurgia è certamente la storia di un settore industriale, ma anche di luoghi, comunità, famiglie e storie come quelle raccontate nel bel romanzo di Silvia Avallone, che ha un titolo piuttosto esplicativo - «Acciaio» - e racconta la storia di famiglie e ragazzi che hanno vissuto

quindi, di poter continuare a garantire la dignità per sé e i propri familiari) e la consapevolezza di doverlo fare a prezzo della propria salute salute e del depauperamento delle risorse ambientali. Io penso che siamo arrivati in una fase in cui bisogna uscire da questo ricatto e abbiamo fatto l'accento con molta forza sui processi di riconversione ecologica che devono attraversare questi settori. Dobbiamo discutere anche di una parola che per alcuni è una parolaccia

con gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che deve essere la guida per ridisegnare un settore nuovo. Si

un ringraziamento particolare a Fratelli d'Italia, ma soprattutto al sottosegretario Pichetto Fratin, perché ha avuto la capacità di trasformare un'ipotetica discussione fra di noi in un ordine del giorno condiviso da tutti su un settore così importante e strategico.

Il merito è andato ad un personaggio mitico nella siderurgia, Oscar Sinigaglia, cui è stato intitolato lo stabilimento di Cornigliano, che ha avuto meriti enormi, ma anche enormi demeriti I meriti sono stati: aver capito che solo un ciclo integrale poteva permettere di costruire l'acciaio a prezzi competitivi; comprendere che in quegli

per fare i vari stabilimenti. Il grande demerito che ci portiamo dietro ancora oggi è quello di aver deciso di costruire i siti degli stabilimenti sulle coste e soprattutto nelle grandi città. aveva il fine di evitare il trasferimento degli operai e talune difficoltà, ma questo è stato lo sbaglio che ancora oggi ci portiamo dietro. Nel 1953 nacquero quindi lo stabilimento di Cornigliano, quello di Taranto, che poi fu sviluppato nel 1970, quello di Piombino e così di seguito. Solo per dare una notizia ai colleghi, Cornigliano era a Genova, insieme a Nervi dalla parte opposta, la spiaggia dorata dei genovesi, era il luogo di villeggiatura dei genovesi, forse come Bagnoli per i napoletani; pertanto quella distruzione fu disastrosa per Genova. Ancora oggi chi arriva a Genova in aereo purtroppo costeggia l'acciaieria di Cornigliano: invece di avere le belle spiagge di Portofino, ha una schifezza *(Applausi)*. Io purtroppo devo dire a tutti quelli che vengono a Genova che è bellissima, ma non ci credono perché quando arrivano in aereo vedono

Quando ho avuto l'onore di fare il Presidente della Regione la prima cosa che ho fatto è stata una battaglia epocale contro Riva, che è stato un ottimo imprenditore per sé stesso *(Applausi),* producendo enormi utili alle sue casse, ma senza rispettare alcun accordo di programma. Ci siamo

industriale al mondo di acciaio. È in 60 Paesi, ha 200.000 dipendenti, fattura 80 miliardi; noi vogliamo mandarlo via? Perché Sabrina Ferilli ha difeso un operaio?

in cui lo Stato è certamente importante. Lo Stato però deve fare il finanziatore, deve controllare che vengano fatti i lavori di riconversione, deve fare quello che deve fare lo Stato e non l'imprenditore. Non ne siamo capaci storicamente. Inoltre, Governo, se vogliamo che le nostre attività industriali siano competitive, dobbiamo renderle tali, non possiamo pagare l'energia tre volte tanto, non possiamo pagare le imposte quattro volte tanto, non possiamo pagare gli interessi due volte tanto rispetto agli

Non sprechiamo questa occasione, non siamo capaci. I commissari sono solo capaci a farsi lo scudo fiscale per loro, a fare le parcelle, a prendersi uno stipendio, a fare delle *slide* che vanno avanti anni e anni *(Applausi)*, come accaduto con Alitalia. Basta,

le sfide che il Paese dovrà affrontare nei confronti del suo posizionamento all'interno della geopolitica che riguarda la parte siderurgica. Evidentemente ognuno di loro è diverso, ogni sito ha la sua peculiarità, ci sono problemi di piani industriali, occupazionali, di transizione e trasformazione energetica dal punto di vista dell'approvvigionamento per la produzione. il Parlamento ha questo ruolo, il Governo ha il suo e noi, come giustamente ricordava il senatore Collina, attraverso l'esercizio degli affari assegnati sull'area di crisi complessa, nelle

è che nel 2021 questi 40 punti percentuali si sono ridotti a 12. Condivido totalmente le preoccupazioni del senatore Biasotti, quando fa cenno alla difficile localizzazione degli attuali impianti. L'acciaieria di Cornigliano ha 1.200 dipendenti ed è sita effettivamente in una posizione strategica, che probabilmente oggi risulta anacronistica. scacchiere geopolitico dal comparto siderurgico è estremamente importante, anche alla luce della difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime Grazie

mette insieme un'enorme richiesta di produzione di acciaio. ormai storica, del ponte sullo Stretto di Messina fosse assolutamente strategica, anche per la produzione dell'acciaio. Se poi riteniamo, come credo facciamo tutti, anche alla luce dell'ordine del giorno, che questo comparto sia assolutamente strategico,

intanto alla salvaguardia dell'occupazione, che mi sembra un altro tema fondamentale, e in modo particolare alla produttività e allo sviluppo.

È evidente che ogni transizione energetica, in modo particolare in questo periodo, è fondamentale e ce lo chiede l'Europa, con la decarbonizzazione e quant'altro. Mi pongo però il problema che questa transizione, molto spesso, non viene vista come non viene vista come un'incidenza sui costi di produzione, perché tale incidenza ci rende probabilmente meno competitivi all'interno dello scacchiere mondiale.

di indicare la crisi come un'opportunità. In questo momento storico, l'ingente impegno di risorse conseguente alla crisi rappresenta una grandissima opportunità. Da questo punto di vista, mi sento tranquillo se ad affrontare questo argomento all'interno del Governo c'è un Ministero che ha

contempla, all'interno del panorama delle possibilità, anche l'intervento pubblico attraverso gli strumenti che abbiamo, per la ricerca di *partner* realmente efficienti. Per questo motivo, a nome

dalla transizione ecologica dichiarata e in atto, dagli obiettivi dell'Agenda 2030 e da quelli più ambiziosi dell'Agenda 2050, a cui l'Italia ambisce e a cui saranno destinate prevalentemente le risorse del *recovery fund*. Nel programmare la transizione industriale, poi, occorre prendere atto dei cambiamenti avvenuti nell'ultimo ventennio proprio nel settore in esame, dove è necessario abbandonare le nostalgie del passato e orientare le scelte su nuovi paradigmi industriali ed economici. Due sono le realtà che si sono contrapposte nel nostro Paese e che, purtroppo, rispecchiano ancora una volta il divario tra Nord e Sud: la produzione a ciclo integrale a carbone e quella a forno elettrico. Quest'ultima è risultata vincente sui mercati, in forte crescita, con un alto valore aggiunto, sostenibile sul piano economico, ambientale e sociale. nella produzione a forno elettrico l'Italia è prima in Europa e tra i primi a livello internazionale. La realtà produttiva a ciclo integrale a carbone, invece, fondata sull'utilizzo del carbon coke, ha avuto un declino inevitabile, ma anche prevedibile, viste le chiusure degli stabilimenti di Bagnoli, prima, di Cornigliano, Piombino e recentemente di Trieste. Trattasi di una realtà produttiva fuori contesto dai mercati, molto impattante su ambiente e salute pubblica, non accettata sul piano sociale, superata sul piano tecnologico, con un basso valore aggiunto, basata sulle economie di scala, ahimè, non più correnti, correnti, concepita per far fronte alle grandi produzioni di massa non più attuali e con un'elevata incidenza del costo del lavoro. A fronte di questa contrapposizione produttiva, le nostre imprese siderurgiche, i nostri imprenditori italiani hanno già scelto: hanno scelto le produzioni a forno elettrico, su cui ormai si concentra l'82 per cento della produzione nazionale, pari a 23 milioni di tonnellate. La produzione a forno elettrico, divenuta progressivamente di eccellenza, si concentra nel Nord del Paese, dove la classe politica e quella imprenditoriale e sindacale hanno saputo prendere decisioni lungimiranti e coraggiose hanno programmato e realizzato per tempo processi virtuosi di transizione industriale ed economica. Tutto questo però - ahimè - non è accaduto per il Sud e per l'ultimo impianto ancora rimasto aperto, quello di Taranto, dove, nell'anno 2020, la produzione ha superato di poco i tre milioni di tonnellate. Per tale impianto, dopo oltre trent'anni di incompiuta, inefficiente gestione, prima pubblica, poi privata, affidata a soggetti prima italiani e poi stranieri, non si è riusciti a dare soluzioni tecnologiche ed economiche valide per soddisfare le primarie ed essenziali esigenze di corretta funzionalità e le necessarie e indispensabili attese di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica. E, tra tutte, la tutela del lavoro. Ciò è dovuto all'eccessiva dimensione e capacità produttiva dell'impianto, all'obsolescenza degli stessi impianti, alla forte concorrenza internazionale, alla qualità e all'elevato costo di produzione, come dimostrano le perdite di di importanti commesse, tra cui quelle nel settore dell'automobile. La crisi dello stabilimento siderurgico di Taranto non è di origine giudiziaria, risalente a quando, nove anni fa, la magistratura sequestrò gli impianti e perseguì penalmente proprietari e dirigenti. Quella fabbrica, Presidente, venne definita fonte di malattia e morte per chi ci lavora e per chi abita nelle vicinanze! È invece una crisi strutturale, dovuta all'obsolescenza degli impianti, all'assenza di investimenti in ammodernamento tecnologico e di processo, di manutenzioni straordinarie e persino ordinarie;

traguardo che non sarà, per l'ennesima volta, raggiunto. Se nel 2020 ArcelorMittal a Taranto ha prodotto e venduto poco più di tre milioni di tonnellate, Presidente, non è perché l'autorità giudiziaria ha impedito di produrre e vendere di più, ma perché l'acciaio prodotto oggi a Taranto non ha mercato, come dimostra, d'altronde, l'avvio della cassa integrazione per crisi di mercato promossa dalla stessa società nel luglio del 2019, quando l'attuale pandemia era relegata al mondo dei brutti sogni. Sullo stabilimento siderurgico di Taranto, quindi, servono scelte coraggiose, all'avanguardia, sostenibili, come avvenuto in altre parti del Paese, garantendo immediati e ingenti investimenti in grado di riconvertire radicalmente i processi produttivi e di rimettere la fabbrica sul mercato, ma con nuove prospettive industriali ed economiche. Per fare questo è necessario abbandonare il ciclo integrale a carbone, non più sostenibile, orientando la produzione a forno elettrico, sperimentando nuovi processi produttivi innovativi, come quello presente nell'accordo stipulato con Invitalia, che è è a forno elettrico, ampliando l'attività di lavorazione, anche favorendo filiere produttive *post* produzione di acciaio, e prevedendo, nel periodo di transizione, un accordo di programma finalizzato a gestire le linee produttive destinate alla chiusura, alla riconversione e alla riqualificazione e reimpiego delle unità lavorative in esubero. Allo stesso tempo è necessario garantire la città, ancora agli ultimi posti per qualità della vita, sia sulla tutela ambientale, sia su quella della salute. Su quest'ultimo profilo ribadisco con forza in questa sede che la valutazione del danno sanitario contenuta nel decreto Balduzzi-Clini del 2013, oggi ancora in vigore, è un'arma spuntata, superata, inefficace e fuori contesto. Tale decreto, emesso dopo il sequestro penale e la pubblicazione dei dati aggiornati dello studio "Sentieri", fa dipendere la valutazione del danno sanitario dalla circostanza in cui i valori per ciascuno degli inquinanti cancerogeni emessi dalla fabbrica superano i limiti stabiliti dalla legge. Si tratta di un paradosso inaccettabile dopo otto anni. Presidente, chiedo pertanto formalmente di voler sollecitare le Commissioni competenti ad accelerare l'*iter* di discussione di una proposta sul tema, a mia prima firma, che prevede la valutazione integrata del danno ambientale a prescindere dal superamento dei valori limite previsti dalla legge. Si tratta di introdurre la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario in modo da poterla contemplare nel prossimo piano ambientale. In un contesto più generale è è opportuno confermare l'orientamento del Governo Conte II di partecipazione dello Stato nel settore, salvaguardare la riconversione *green* e la diversificazione produttiva dell'impianto ex Ilva di Taranto che contempli soprattutto orizzonti mai sperimentati. La recente mancanza di continuità e decisioni da parte dell'attuale Governo sta provocando incertezze, ritardi, rischi di incidenti in fabbrica, tensioni tra i lavoratori e, persino, licenziamenti di lavoratori per un semplice *post* su Facebook. Facebook. Presidente, le possibili decisioni su tale impianto dipendono da un ricorso per la chiusura dell'area a caldo al Consiglio di Stato, che verrà discusso il prossimo 13 maggio, dal rischio di confisca legato al processo «Ambiente svenduto» e da una sentenza di condanna dell'Italia emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo del 2019

del giorno in esame, con la richiesta di reintrodurre lo scudo penale, offende la civiltà di un Paese

esprimo voto in dissenso rispetto all'ordine del giorno presentato. Ho ascoltato attentamente gli interventi soprattutto di Forza Italia e Fratelli d'Italia, che sono indignati più per il fatto che la Ferilli vuole difendere da una multinazionale che tratta con arroganza il nostro Paese che non per il lavoro e la dignità di una persona. Nell'ordine del giorno si fa riferimento al mantenimento della *partnership* con ArcelorMittal, facendo finta che due anni fa ArcelorMittal non sia arrivata alle minacce di chiudere gli altiforni solo perché avevamo eseguito una sentenza della Corte costituzionale che dice che, qualora si rispetti l'autorizzazione

dovrebbe seguire la legge e trattare con rispetto la città che la ospita. Qui si deve giungere finalmente a una soluzione chiara e definitiva, perché, dopo che tutti i Gruppi, in questo anno così drammatico, si sono sciacquati la bocca sulla salute pubblica e sulla dominanza della salute sull'economia, questo ancora non vale per Taranto e per i tarantini, i possono anche morire, possono anche ammalarsi, possono anche avere dei rappresentanti, come Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che mettono l'acciaio alla salute dei bambini. *(Applausi)*. E ancora si discute in Parlamento di una cosa così scandalosa! Andate a dirlo a Taranto. Quindi, dal momento che ancora una volta su Taranto si prendono delle posizioni fumose, ideologiche e senza alcun riferimento sano e solido sulla salute e sull'economia, noi voteremo contro.

Signor Presidente, colleghi, da quasi quindici mesi Patrick Zaki, studente e ricercatore dell'Università di Bologna, attivista per i diritti umani, è imprigionato nelle carceri egiziane per la sola colpa delle sue idee. Dal 7 febbraio 2020 è sottoposto ripetutamente, senza prove e senza processo, a quella che viene chiamata detenzione preventiva, ma che è a tutti gli effetti una detenzione arbitraria e una violazione dei diritti umani. Patrick è stato picchiato e torturato con scariche elettriche, come denunciato dai suoi legali. Le accuse contro di lui sono pretestuose e, come lui, sono migliaia i "prigionieri di coscienza" (come vengono definiti dalle organizzazioni umanitarie) che sono stati incarcerati in Egitto negli ultimi anni (avvocati, intellettuali, cittadini comuni). La detenzione prolungata è una tecnica intimidatoria che vuole cancellare e far dimenticare vite, storie, volti, nomi, rivendicazioni. Ma la storia di Zaki non deve e non può essere cancellata, perché è una storia importante, più grande ancora del suo destino personale: è una storia di multiculturalismo, di incontro tra mondi diversi che vogliono stare insieme. Zaki è tra le centinaia di ragazzi di tutto il mondo che partecipano al bando per la borsa di studio europea Erasmus Mundus, è tra i pochissimi a vincerla e per questo arriva a Bologna. Zaki ha scelto l'Europa e ha scelto l'Italia, dove studiare e poter essere libero di esprimere le proprie idee e le proprie convinzioni; è diventato parte di qualcosa di universale, la comunità studentesca e universitaria. In una lettera alla madre, qualche settimana fa, ha scritto: «Voglio mandare il mio amore ai miei compagni di classe e agli amici di Bologna. Mi mancano la mia casa, le strade, l'università». questo sentimento di Zaki è ricambiato da una grande spinta emotiva che ovunque in Italia ha portato molti Comuni ad attivarsi per conferirgli la cittadinanza onoraria, come già hanno fatto le città di Bologna e di Milano; la conferenza dei rettori delle università a chiederne formalmente l'immediata liberazione; e oltre 200.000 cittadini a firmare la petizione sostenuta da molte associazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana, come chiesto a gran voce dalla consulta degli studenti

in questa mozione che ho l'onore di presentare e che è sostenuta dalla quasi totalità dei Gruppi parlamentari, ognuno dei quali voglio ringraziare. Una mozione che diventerà un ordine del giorno più ampio che terrà insieme entrambi gli atti che oggi vengono presentati. La reclusione e la sorte di Zaki rende più profonda la ferita del sequestro, della tortura, dell'omicidio di Giulio Regeni. Abbiamo il dovere di non smettere mai di pretendere dalle autorità egiziane verità e giustizia per Giulio. *(Applausi)*. Le vite di Giulio e di Zaki sono legate: entrambi giovani ricercatori, entrambi innamorati dell'Italia e dell'Egitto. E tra i tanti *murales* a loro dedicati, comparsi in questi mesi, ce n'è uno molto bello che li ritrae abbracciati e sorridenti, con Giulio che dice, rivolto a Zaki: «Stavolta andrà tutto bene». Ebbene, abbiamo il dovere di far sì che questo avvenga, di non lasciare nulla di intentato. Questa mozione può salvare la vita di Zaki e dimostrare che per l'Italia lo Stato di diritto è una frontiera irrinunciabile, non derogabile. A dare a questa mozione un significato speciale

il nome di Liliana Segre porta con sé l'enormità della storia, il monito contro ogni discriminazione, contro ogni totalitarismo, contro ogni violazione dei diritti umani e dei diritti civili, contro ogni indifferenza. Solo pochi giorni fa Zaki ha affidato alla sua compagna, nascosto tra le pagine di un libro, «Cent'anni di solitudine», un messaggio scritto in italiano e rivolto a noi, che dice: «Ancora sto resistendo. Grazie per il supporto a tutti». Signor Presidente, quando Zaki saprà che avremo approvato questa mozione, alla presenza di Liliana Segre in quest'Aula, potrà essere orgoglioso dell'Italia, il Paese che ha scelto, e anche noi, signor Presidente, potremo esserlo quando finalmente Zaki sarà di nuovo libero.

Signor Presidente, ho sottoscritto la mozione del senatore Verducci poiché credo fermamente che la concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki sia un atto dall'alto valore simbolico.

e ci è stato segnalato il caso di questo giovane studente. Mi sono mobilitata e ringrazio tutte le colleghe della Commissione straordinaria per i diritti umani, che insieme a me hanno sostenuto questa mobilitazione in Commissione e che mi Commissione e che mi hanno supportata nel mio continuo promuovere iniziative, non ultima quella di costituire un osservatorio permanente sul caso di Patrick. L'osservatorio purtroppo non ha potuto

che la Presidenza si ricostituisca il prima possibile per continuare questo lavoro prezioso della Commissione per i diritti umani, che si inserisce nel solco di una mobilitazione nazionale ed internazionale di cui la mia Bologna si è fatta capofila,

tante iniziative, anche una maratona musicale, per richiamare l'attenzione sul caso di Zaki e per far capire che anche la nostra cultura è presente a fianco di Patrick Zaki. L'impegno costante della Commissione per i diritti umani si inserisce anche in un solco internazionale, perché il 18 dicembre 2020 il Parlamento europeo ha approvato una proposta di risoluzione comune sulle violazioni dei diritti umani in Egitto e successivamente anche il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, il 12 marzo 2021, ha espresso in una nota la profonda preoccupazione

a un certo punto sembrava quasi non potesse più accadere - siamo qui a discutere e ad approvare delle mozioni importanti, non solo quella che chiede al Governo di impegnarsi per farsi per farsi promotore, presso la Presidenza della Repubblica, dell'emanazione di un decreto di concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, ma per spingerci oltre. per spingerci oltre. Infatti, se la concessione della cittadinanza italiana ha un valore altamente simbolico, comunque dobbiamo continuare a perseguire l'obiettivo della liberazione di Patrick Zaki. Patrick ha voglia di tornare nella sua Bologna, nelle piazze di Bologna, insieme agli studenti, a parlare del futuro, a scambiare opinioni sui cambiamenti, a dare vita a quell'incubatore di intelligenze vivaci di cui sono promotori i nostri i nostri studenti quando si incontrano nei contesti internazionali. Il caso di Patrick Zaki porta alla luce una situazione anche più ampia di *academic freedom*, di libertà all'interno delle università, di libertà di ricerca, di libertà nelle accademie, che oggi sono messe in discussione e sono in gravissimo pericolo. Ciò significa mettere in pericolo le istituzioni che diffondono la nostra conoscenza. Oltre al riconoscimento della cittadinanza italiana, che chiaramente aumenterebbe la pressione diplomatica - voglio qui ringraziare la nostra ambasciata al Cairo, che già sta fornendo la massima assistenza al caso e vorrei sottolineare che dopo lo *stop* all'ingresso degli osservatori stranieri alle udienze, la diplomazia italiana sta lavorando per ripristinare il monitoraggio processuale internazionale, al quale l'Egitto non può sottrarsi - il MoVimento 5 Stelle ha voluto presentare una sua mozione in cui

per sollecitare l'immediata liberazione di Patrick Zaki», ma - è questo il punto giuridico fondamentale - valutando la possibilità dell'utilizzo degli strumenti previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984;

che l'Italia si faccia promotore attivo, all'interno di un consesso internazionale come il G7, del tema del rispetto dei diritti umani e della tutela dei difensori dei diritti umani,

l'ipocrisia e portare con coraggio questi temi nei consessi internazionali, per richiamare l'attenzione di tutti e ragionare insieme su come recuperare questo valore altissimo e concreto, non astratto. Dunque,

è stato fatto un lavoro per confluire in un unico ordine del giorno. Al riguardo ringrazio il senatore Verducci e tutte le forze politiche che hanno contribuito a questo sforzo.

Comunico che, in relazione alla avvenuta presentazione dell'ordine del giorno G1, come testé anticipato dalla senatrice

Signor Presidente, colleghi, senatore Verducci,

Noi oggi siamo chiamati ad un atto che è molto particolare; non si tratta solo di esprimere solidarietà alla persona, a Zaki, ad uno studente che a Bologna si è segnalato solo per elementi di positività, di entusiasmo e di impegno. No. Noi oggi siamo chiamati ad un esercizio diverso, colleghi, e la presenza qui in Aula della vice ministro Sereni ci richiama a questo nostro dovere. Noi oggi discutiamo sulla possibilità che la politica estera si misuri con alcune questioni fondamentali che per noi sono beni indisponibili, tra cui, ad esempio,

siamo firmatari di una Convenzione ONU del 1984 contro le torture, le punizioni inumane e degradanti. cioè, come l'Egitto, come Stato, abbiamo firmato un impegno che dovrebbe vincolare i nostri sistemi Paesi. vediamo che questo ragazzo, da quindici mesi, senza una condanna e una imputazione specifica, si trova nelle carceri di un Paese, dove, peraltro, esistono preoccupanti analogie con casi di altre persone - penso al giornalista di «Al Jazeera» -che, da diversi anni, senza imputazioni o condanne stanno nelle carceri egiziane.

Il popolo italiano è unito al popolo egiziano e noi abbiamo la chiara consapevolezza dell'importanza che l'Egitto ha ha nel Mediterraneo. Noi vogliamo collaborare con l'Egitto. Noi sappiamo benissimo che l'Egitto è importante per la stabilizzazione della Libia, per le questioni energetiche del Mediterraneo, sappiamo che l'Egitto è un bastione contro i rischi del terrorismo e della sua espansione nel Mediterraneo. Proprio per questo richiamiamo le autorità egiziane a un rispetto dei diritti dell'uomo, perché non è in nessun modo possibile macchiare tutti gli elementi di positività, che noi vediamo in questo Paese, con un comportamento che è del tutto intollerabile. Noi non vogliamo esportare la democrazia, come diceva il presidente americano Bush, perché sappiamo che la questione è molto più complessa, perché sappiamo che ci scontriamo con Paesi nel mondo che hanno una concezione anche religiosa antitetica alla nostra. Quindi, esportare la democrazia, come se fosse possibile farlo in modo automatico, è un atto che addirittura potrebbe essere anche di arroganza da parte nostra. Ci sono, però, dei diritti inalienabili. Ci sono dei confini oltre i quali il compromesso della politica estera incontra dei limiti e delle barriere. Noi siamo arrivati a questi limiti. Siamo arrivati a questi limiti che per noi non è possibile in alcun modo varcare, perché perché significherebbe complicità con atteggiamenti che noi riteniamo antiumani. Terminando, dico alle autorità egiziane, ringraziando anche l'ambasciata per quello che fa in modo encomiabile, che noi abbiamo una ferita che non è chiusa, ma è aperta, che è quella di Giulio Regeni, vicenda sulla quale non abbiamo avuto una risposta in termini di collaborazioni istituzionali, come pure ci era stato promesso e come pure noi speravamo di avere, come autorità dello Stato italiano, Parlamento e Governo. Colleghi, questo atto di indirizzo per dare la cittadinanza a Patrick Zaki è, dunque, un atto, secondo me, di grande decoro e dignità del Parlamento, che acquisisce un punto fermo tra tutte le forze politiche. Dove i diritti individuali delle persone vengono sistematicamente violati, noi dobbiamo dire una parola di libertà e di verità. Signor Presidente, saluto e ringrazio il Governo e la viceministro Sereni il collega Verducci. È bene fare anche un po' di storia. Il 7 febbraio 2020, più di un anno fa, veniva arrestato al Cairo Patrick Zaki. Il fermo è avvenuto appena lo studente egiziano aveva messo piede in Egitto, dove era tornato per una breve vacanza e per vedere i genitori. Arrivava da Bologna, dove si era trasferito dal settembre 2019 per seguire un *master*. Dopo l'arresto, ventiquattro ore di *blackout*, durante le quali, secondo le denunce di legali e attivisti, Zaki è stato interrogato e torturato. Poi, l'8 febbraio, la formalizzazione dello stato di arresto. Da allora è nel carcere di Tora, in attesa di processo, dopo svariati rinnovi di custodia cautelare con accuse che vanno dalla propaganda sovversiva al terrorismo, solo per alcuni *post* sui *social*, che peraltro la sua difesa sostiene essere falsi. I reati che gli sono stati contestati sono quelli di istigazione, proteste e propaganda per il terrorismo sul proprio profilo Facebook, cioè di aver pubblicato notizie false con l'intento di disturbare la pace sociale, di aver incitato proteste contro l'autorità pubblica, di aver sostenuto il rovesciamento dello stato egiziano usando i *social network* e di aver istigato alla violenza e al terrorismo; Per quei messaggi Patrick rischia fino a venticinque anni di carcere. Si susseguono inoltre continui rinvii delle udienze preliminari per mezzo di provvedimenti pronunciati da una magistratura priva delle più elementari garanzie di indipendenza dal potere esecutivo. Proprio qualche giorno fa la corte d'assise del Cairo ha rinnovato di altri quarantacinque giorni la detenzione del ricercatore egiziano ed è stata inoltre respinta la richiesta presentata dalla difesa di un cambio dei giudici che seguono il caso. Secondo le stime di Amnesty International il tempo medio di detenzione in un penitenziario egiziano è di trecentoquarantacinque giorni, ma esistono casi che superano i mille giorni. Nel rapporto «Stato d'eccezione permanente» si evidenzia il disinvolto uso da parte della procura di forme di tortura quale mezzo per estorcere confessioni, nonché la complicità nelle sparizioni forzate operate dall'agenzia di sicurezza nazionale. Sempre nel documento, infine, si rileva che la procura omette sistematicamente di informare i detenuti dei loro diritti, nega loro l'accesso agli avvocati e li sottopone a interrogatori coercitivi in cui sono bendati, trattenuti in condizioni inumane e minacciati di ulteriori interrogatori e torture da parte dell'agenzia di sicurezza nazionale. Insomma, il ruolo della cosiddetta procura suprema per la sicurezza dello Stato, che è un ramo speciale del pubblico ministero responsabile di perseguire i crimini che riguardano la sicurezza dello Stato, ha poi subito una significativa espansione nel sistema giudiziario egiziano. egiziano. Queste violazioni hanno un impatto più ampio su altri diritti, tra cui quelli alla libertà di espressione, associazione, assemblea e partecipazione politica, creando un senso pervasivo di paura. È passato più di un anno da quel tragico arresto, ma nessuna petizione e protesta è purtroppo riuscita a esercitare una pressione tale da portare a una sua scarcerazione da parte del Governo egiziano.

rapporto del 2016 appare evidente un progressivo aumento di rapimenti di studenti, attivisti e manifestanti, anche minorenni, spariti per opera del sistema di repressione dello Stato. Quindi, come Patrick Zaki ce ne sono altri. sono altri. Occorre oggi fare una scelta. Dobbiamo prendere una netta posizione sulla questione dei diritti umani, in nome di una chiara adesione ai valori di libertà e giustizia che fondano la nostra Costituzione. Dobbiamo farci portavoce di questa battaglia di civiltà, schierandoci dalla parte di Patrick e di tutti gli altri che, come lui, sono ingiustamente detenuti in Egitto. La storia di Zaki non è una faccenda egiziana di cui l'Italia può disinteressarsi, come sostenuto anche dal Ministero dell'interno e dalla stampa egiziani. Sono state raccolte circa 200.000 firme e più di 1.000 Comuni italiani hanno votato per la cittadinanza onoraria di Zaki.

Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la dizione della mozione e poi dell'ordine del giorno in esame è che ricorre un eccezionale interesse dello Stato italiano a concedere la cittadinanza italiana allo studente Zaki. allo studente Zaki. La cittadinanza è l'appartenenza a un insieme di valori e di principi, in virtù dei quali si è titolari di diritti e di doveri in un sistema democratico e liberale questi diritti umani sono esigibili. Pertanto, la questione della cittadinanza è collegata collegata a un sistema compiuto di garanzie: l'effettività dei diritti umani è collegata a un sistema di garanzie ancorate alla Costituzione, che hanno hanno il baricentro in un diritto di libertà, in un diritto di opinione, come è stato ricordato, ma soprattutto anche in un diritto all'inviolabilità della persona, che può essere limitata soltanto in virtù di provvedimenti giudiziari in un sistema di garanzie motivate, trasparenti, impugnabili. Il *vulnus* della vicenda dello studente Zaki La cittadinanza prevede che non si possa essere privati della libertà senza un processo giusto, o in alternativa anche prima di un processo, se non con motivate esigenze

La libertà e la cittadinanza implicano l'inviolabilità della dignità della persona e, soprattutto, non può mai essere un arbitrio del potere politico, anche se legittimato dal voto, privare o limitare la libertà delle persone. La cittadinanza e questi diritti implicano anche un diritto alla verità, che appartiene ai cittadini, al popolo, nell'universalità dei diritti umani. Per questo ci richiamiamo alla Dichiarazione universale dei diritti umani diritti umani e questa idea di cittadinanza, questa idea di Europa, che però vogliamo sia universale, ci richiama a un diritto mite, a uno Stato che è per un diritto mite. Tuttavia, a questo diritto mite corrisponde la prepotenza del nostro grido, che si leva alto e chiaro, per la libertà delle persone, per la tutela dei loro diritti, per l'inviolabilità della dignità della persona. Con la mozione in discussione vogliamo anche affermare l'obiettivo che questa universalità dei diritti umani, che ha radici nella dichiarazione del 1948 (non a caso a Parigi), non potrà mai muoversi secondo una convergenza parallela, una linea parallela alle politiche degli Stati e ai rapporti tra di loro.

accusato di diffondere notizie false, di attentare alla sicurezza nazionale dell'Egitto, accusato cioè di battersi per i diritti civili nel tuo Paese dove è al potere il regime di al-Sisi. Amnesty international considera Patrick Zaki un prigioniero di coscienza, detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui *social media.*

a Patrick Zaki, ricercatore egiziano, studente dell'Università di Bologna, detenuto in una prigione egiziana dal 7 febbraio dell'anno scorso. La battaglia per la libertà di Zaki è una battaglia di tutti perché i diritti di Patrick Zaki sono i diritti di tutti. Questo è un caso di detenzione arbitraria che ha colpito l'opinione pubblica del nostro Paese. Non siamo i soli a essere preoccupati per le violazioni dei diritti umani in Egitto; 31 Stati hanno sottoscritto di recente una dichiarazione al Consiglio ONU dei diritti umani Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle violazioni dei diritti umani in Egitto, citando come esempi i casi di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016, e Patrick Zaki. Le autorità egiziane si rifiutano di rivelare il numero dei detenuti presenti nelle carceri. Organizzazioni non governative impegnate per i diritti umani stimano che il numero sia di 114.000, oltre il doppio della capienza massima indicata dal presidente al-Sisi. Dal 2014 in Egitto sarebbero state eseguite almeno 165 condanne a morte. poi l'omicidio di Giulio Regeni; sì, l'orrendo omicidio del ricercatore italiano rapito il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo,

Come possiamo coniugare i nostri interessi strategici, i rapporti diplomatici e di cooperazione con l'Egitto di al-Sisi, responsabile dell'omicidio di Giulio Regeni e della detenzione illegale di Patrick Zaki. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ci dà una risposta quando definisce il presidente turco Erdoğan un dittatore. Si deve essere franchi - ha detto il presidente Draghi - nell'esprimere le proprie diversità di vedute, di opinioni e di visioni della società si deve essere anche pronti a cooperare per assicurare gli interessi del proprio Paese. Bisogna trovare l'equilibrio giusto. Vi chiedo e mi chiedo quale sia l'equilibrio giusto con l'Egitto che tiene in carcere illegalmente Patrick Zaki e che è responsabile dell'omicidio di Giulio Regeni. Sappiamo che sta facendo rotta verso l'Egitto la seconda fregata Fremm, destinata alla Marina egiziana e stiamo sostenendo nei fatti il regime egiziano con forniture militari. Non si possono vendere armi a un Paese in cui si violano i diritti umani e civili. Colleghe e colleghi, abbiamo il dovere di chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni e approvando oggi la mozione per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki impegniamo il Governo ad intraprendere ogni ulteriore iniziativa presso le autorità egiziane per sollecitarne l'immediata liberazione. L'impegno che prendiamo oggi è quello di batterci perché Patrick Zaki possa riabbracciare al più presto, da uomo libero, la sua famiglia, i suoi amici e i suoi compagni dell'Università di Bologna. Caro Zaki, non ti lasceremo solo.

umani. La repressione del pensiero critico e la compressione dei diritti umani sono ancora troppo diffuse; penso non solo all'Egitto di al-Sisi, ma anche alla Turchia di Erdoğan, all'Arabia Saudita del principe bin Salmān. Si pensi al brutale assassinio di Jamal Khashoggi, ai territori occupati da Israele in Palestina, al Myanmar della giunta militare golpista. Quando si sente parlare di diritti umani, oggi si si fa sempre più riferimento a qualcosa di astratto e lontano, un ideale da perseguire solo perché è giusto portarlo avanti, perché certe convenzioni sociali ci dicono che è opportuno farlo. Presidente, colleghi, i diritti umani non sono negoziabili e il Parlamento oggi vuole dare un chiaro e forte segnale in tal senso. Siamo privilegiati, abbiamo la fortuna di vivere in una parte del mondo in cui non dobbiamo preoccuparci di cosa diciamo e di cosa pensiamo, siamo liberi di scrivere un *post* su un *social* o di manifestare in piazza contro quelle che per noi sono ingiustizie. I nostri studenti possono svolgere ricerche su ogni tematica, possiamo professare liberamente la nostra fede, senza temere ripercussioni da parte dello Stato. Colleghe e colleghi, prendiamoci un attimo per riflettere veramente su cosa ciò significhi e, ancor di più, su cosa significherebbe non avere queste possibilità. I diritti umani sono un elemento costitutivo della pace, che non è solo assenza di conflitto, ma significa creazione di sistemi giusti, che garantiscano la pace sociale, lo Stato di diritto e le libertà fondamentali di tutti gli individui. Esistono però, purtroppo, molti casi in cui le basilari fondamenta di uno Stato libero e moderno non riescono a tutelare i cittadini. Voglio ricordare con dolore i Paesi in cui le donne vengono sottoposte a orribili mutilazioni genitali quelli che puniscono gli individui per il loro orientamento sessuale. Signor Presidente, colleghe e colleghi, non dimenticheremo mai la barbarica uccisione del nostro Giulio Regeni, sulla quale non smetteremo mai di chiedere verità e giustizia. Rischiamo infatti di compiere un errore imperdonabile, di dare per scontate le libertà fondamentali e di diventare sempre più anestetizzati di fronte alle ingiustizie. Il moltiplicarsi dei casi di tortura fisica e psicologica nel mondo non deve lasciare indifferenti, solo perché sono lontani da noi. Oggi, come è stato detto, affrontiamo la dolorosissima vicenda del sequestro - perché di questo si tratta - di Patrick Zaki, cittadino egiziano, detenuto dal febbraio 2020 in carcere in Egitto, senza un giusto processo. motivo della detenzione sarebbero alcuni *post* sui *social*, che per il Cairo sono stati sufficienti a mettere Patrick in stato di fermo. Con una serie di udienze farsa, che rappresentano chiaramente un accanimento giudiziario, sono ormai quindici mesi che Zaki è privato della libertà, in un modo che viola ogni basilare principio dello Stato di diritto. I suoi avvocati hanno riportato che è stato bendato e ammanettato per ore, mentre veniva interrogato da professionisti della tortura. Come accaduto per Regeni, Zaki è stato sottoposto a scosse elettriche e percosse, in maniera da non lasciare tracce sul corpo. L'Egitto, come diceva anche il senatore Casini, ha un ruolo geopolitico di fondamentale importanza sul piano internazionale e ancor di più locale, ma nessun ruolo politico ed economico potrà mai giustificare certi metodi medioevali. La storia ci ha donato strumenti internazionali per assicurare che alcune linee non venissero mai superate e per assicurare che ogni essere umano potesse vivere una vita degna di essere chiamata tale. È il caso della Convenzione contro la tortura adottata dalle Nazioni Unite nel 1984. L'Egitto è parte della Convenzione dal 1986, tuttavia sembrerebbe non osservarne i principi fondanti. Concludo dicendo che quanto accaduto a Zaki, come a tanti altri attivisti, giornalisti e studenti, ci deve sconvolgere e far paura. È proprio questa paura, quella stessa paura che Zaki vive ogni giorno, ogni giorno, che deve spingerci non solo a condannare tali pratiche disumane, ma anche e soprattutto a chiedere con forza una soluzione, affinché nessun individuo debba mai più scontare il peso della negata libertà.

Signor Presidente, senatori e senatrici, il Governo segue con la massima attenzione il caso di Patrick George Zaki sin dalle prime ore successive all'arresto del giovane e condivide pienamente la preoccupazione espressa con l'atto parlamentare in oggetto, anche alla luce dell'ulteriore proroga della sua custodia cautelare in esito all'udienza dello scorso 5 aprile. L'azione di sensibilizzazione sulle autorità egiziane, che abbiamo svolto e continuiamo a svolgere sia a livello bilaterale - in particolare, tramite la nostra ambasciata al Cairo - sia nei *fora* multilaterali, è continua: sollecitiamo le controparti egiziane in ogni occasione di confronto a rilasciare lo studente. Seguiamo direttamente anche l'evoluzione del processo. Su nostra richiesta, infatti, il procedimento giudiziario nei confronti dello studente è stato inserito nel programma di monitoraggio processuale dell'Unione europea, pochissimi giorni dopo il suo arresto. Abbiamo insistito a tutti i livelli affinché il meccanismo europeo sopra descritto e coordinato dall'Unione europea, che era stato sospeso prima dell'estate per i rischi legati al Covid, venisse al più presto riattivato, non solo per Zaki, ma per tutti i casi qualificati come sensibili. Si tratta, infatti, a nostro avviso, di uno strumento fondamentale per la promozione dei diritti umani. Questa nostra posizione è stata condivisa dalla delegazione dell'Unione europea al Cairo e il meccanismo è stato immediatamente applicato al caso dello studente egiziano e ad altri. Anche nei mesi in cui il meccanismo era quasi del tutto inattivo per via della situazione epidemiologica, un gruppo di Paesi europei ed extraeuropei ha mantenuto un costante monitoraggio sulla vicenda di Patrick. Ciò è avvenuto grazie alla tenace opera di sensibilizzazione condotta dalla nostra ambasciata al Cairo, che ha continuato a inviare un proprio funzionario alle udienze, coinvolgendo di volta in volta altri *partner* europei e internazionali. Grazie a questa azione incessante, alle ultime udienze hanno partecipato, in varie forme, oltre ai diplomatici italiani, funzionari di Francia, Germania, Spagna, Belgio, Olanda, Danimarca, Stati Uniti e Canada. Anche in occasione della più recente udienza del 5 aprile, pur nelle circostanze collegate alla scelta della difesa del giovane di non partecipare all'udienza per sostenere la richiesta di una sostituzione del collegio giudicante, un funzionario della nostra ambasciata al Cairo si è recato presso il tribunale assieme ai colleghi di Francia e Canada, mentre gli Stati Uniti hanno depositato una lettera per rimarcare la loro attenzione verso il caso. L'Italia ha portato la questione del rispetto dei diritti umani nel Paese all'attenzione dell'Unione europea e del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Lo scorso 18 dicembre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui, citando esplicitamente Regeni e Zaki, si chiede un'indagine indipendente sui diritti umani in Egitto. Il 25 gennaio, quinto anniversario del sequestro di Giulio Regeni, il ministro Di Maio è intervenuto in occasione del Consiglio affari esteri dell'Unione europea per chiedere all'Unione di fare uso degli strumenti a sua disposizione affinché il Cairo compia progressi concreti in tema di diritti fondamentali. In occasione del segmento di alto livello della 46a sessione del Consiglio per i diritti umani dell'ONU, lo scorso 24 febbraio, il ministro Di Maio ha sollevato nuovamente il caso del giovane richiedendone il rilascio. Abbiamo inoltre sottoscritto la dichiarazione congiunta sull'Egitto e la situazione dei diritti umani nel Paese, pronunciata in Consiglio per i diritti umani l'11 marzo dalla Finlandia, a nome di 31 Paesi tra cui gli Stati Uniti, mentre il 12 marzo, su nostra iniziativa, è stato inserito un riferimento specifico alla vicenda dello studente nel discorso pronunciato dall'Unione europea al Consiglio. È importante sottolineare che l'impegno del Governo non riguarda soltanto il caso di Patrick Zaki, ma il complesso delle questioni relative ai diritti umani nel Paese e non solo. Conduciamo da anni un lavoro coerente e costante a difesa della centralità della persona e della sua tutela, in Egitto così come nel mondo, in linea con le nostre consolidate priorità di politica estera e con i valori su cui esse si fondano: il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e della tutela dei diritti umani. Sono valori su cui non arretriamo, avendo ben chiaro il quadro complessivo dei rapporti bilaterali. Sebbene le relazioni con Il Cairo restino fortemente compromesse dalla drammatica vicenda del nostro connazionale Regeni e perciò depotenziate fintanto che non sarà fatta piena verità su questo caso, l'Egitto rimane un Paese cruciale su *dossier* come la stabilizzazione della Libia, il Mediterraneo Orientale, la collaborazione nella lotta al terrorismo e ai traffici illeciti, la gestione dei flussi migratori, come è stato qui ricordato sia dal senatore Casini che dal senatore Ferrara. Ma sui valori non si arretra. Con riferimento all'eventuale attribuzione della cittadinanza italiana a Zaki, si riconosce la portata ideale, simbolica e umanitaria del possibile gesto, al pari delle altre numerose iniziative susseguitesi in questi mesi da parte di enti locali, ONG e associazioni, a testimonianza della sensibilità della società civile italiana su questi temi; una sensibilità in cui l'azione del Governo si rispecchia e di cui si avvale al fine di ribadire la propria fermezza in materia di diritti umani in ogni foro bilaterale e multilaterale. Sottolineo, tuttavia, l'importanza che la mozione oggi in discussione, nel testo da ultimo presentato - testo sul quale approfitto per esprimere fin da ora il parere favorevole del Governo faccia riferimento anche alla necessità di verifica di tutte le condizioni in vista della possibile concessione della cittadinanza. Vorrei attirare in questa sede l'attenzione sull'esigenza di una valutazione approfondita delle circostanze di contesto in cui tale eventuale riconoscimento andrebbe ad inserirsi. Invito me stessa e tutti noi a riflettere, in particolare, su due punti. In premessa, va considerata la circostanza per cui l'attribuzione della cittadinanza italiana a Zaki si configurerebbe, in definitiva, quale misura simbolica, priva di effetti pratici a tutela dell'interessato. Anche alla luce del diritto e dei principi internazionali, l'Italia incontrerebbe, infatti, notevoli difficoltà a fornire protezione consolare al giovane, essendo egli anche cittadino egiziano, poiché prevarrebbe la cittadinanza originaria, principio applicato peraltro dall'Egitto in maniera particolarmente stringente. Ancor più importante è addirittura il rischio, da valutare, di effetti negativi sull'obiettivo che più ci sta a cuore: ottenere il rilascio di Patrick. In questo senso, la concessione della cittadinanza potrebbe - dico "potrebbe", per questo chiediamo e accettiamo l'idea di una verifica - addirittura rivelarsi controproducente ed è responsabilità di tutti noi fare una riflessione su questo. Il Governo continuerà a seguire il caso Zaki con la massima attenzione, in raccordo con i *partner* che sostengono numerosi l'azione dell'Italia in questo campo. Porteremo avanti ogni possibile iniziativa di sensibilizzazione sul piano bilaterale nell'ambito del coordinamento europeo e a livello multilaterale, per raggiungere l'obiettivo cui tutti lavoriamo: la liberazione di Patrick.

ma tra queste non c'è Patrik, nonostante i problemi di salute. Quale sarebbe, allora, l'immane delitto compiuto da questo ragazzo, tanto da essere attenzionato dai Servizi egiziani mentre studiava a Bologna, arrestato non appena atterrato in Egitto, sottoposto ad atroci torture e, infine, trasferito in un carcere di massima sicurezza? Cosa c'è di così grave da rendere le autorità egiziane completamente sorde alle richieste dell'Italia e dell'Europa, alle manifestazioni di protesta, agli appelli delle organizzazioni umanitarie? Niente, se non un regime che già una volta è stato capace - come disse la mamma di Giulio Regeni - di tutto il male del mondo; un regime paranoico che vive come un'intollerabile minaccia ai giovani colti allergici ai pregiudizi e alle ingiustizie. È per questo che, pensando a Patrick, non solo viene in mente Regeni, ma tornano alla memoria anche Antonio Megalizzi, Fabrizia Di Lorenzo e Valeria Solesin. È proprio pensando a loro che Patrick è a tutti gli effetti un cittadino italiano ed europeo. Lo è perché con il suo giovane, ma intenso percorso di vita ha coltivato gli stessi valori fondativi delle nostre società. Abbiamo, quindi, un vincolo morale, come abbiamo un debito molto grande verso Giulio Regeni e la sua famiglia. Come ha scritto Luigi Manconi, qui non è in ballo un utopico idealismo contrapposto al realismo della ragion di Stato. Uno Stato esprime la propria legittimità attraverso pochi, ma chiari elementi e, tra questi, c'è la difesa dell'incolumità dei suoi cittadini e, quindi, nessuna sudditanza psicologica nei confronti di un regime dove i dissidenti vengono torturati e dove gli appelli alla ricerca della verità vengono sistematicamente disattesi. Negli ultimi tempi emergono frammenti di un'aggressività di regimi illiberali verso l'Italia e l'Europa. Penso non solo all'Egitto, ma anche alla vicenda dello spionaggio russo e allo sgarbo di Erdogan. La sensazione è che, al di là delle parole, poco o nulla si faccia per ripristinare la dovuta correttezza nei rapporti con quei Paesi. Presidente, credo allora che il lavoro del Senato non debba concludersi con l'approvazione di questa mozione. Mesi fa alcuni colleghi le hanno scritto per chiedere una missione del Senato nel carcere dove Zaki è detenuto. Credo che questa richiesta sia più che mai opportuna. Basta con i balletti di parole! L'Europa, l'Italia e anche il Senato si facciano carico di un'iniziativa per la liberazione di Zaki. Il riconoscimento della cittadinanza italiana sia solo il primo passo.

Bologna, Firenze, Bari, Milano, Procida, Bisceglie, Udine, Lauria, Pisa sono tra le sono tra le oltre 200 città italiane, da Nord a Sud, da Est a Ovest, che hanno accolto l'appello della società civile e si sono dette pronte a conferire la cittadinanza onoraria al giovane studente Patrick Zaki. Molte di queste città hanno anche già deliberato. A loro si aggiungono centinaia di migliaia di firme raccolte dagli attivisti di diverse realtà associative per trasmettere insieme un segnale di vicinanza al ragazzo e ai suoi familiari e per chiedere con forza al Governo di conferire, a sua volta, la cittadinanza onoraria italiana a Patrick Zaki, così da avere ancora più legittimità nel pretendere dall'Egitto la sua liberazione. Noi oggi facciamo nostra con convinzione la richiesta delle tante amministrazioni italiane e dei tanti cittadini che già si sono mobilitati per chiedere che il giovane ricercatore venga rimesso in libertà e possa tornare ai suoi studi. L'hanno già detto bene alcuni colleghi: Patrick è uno di noi; Patrick è un nostro studente, iscritto all'Ateneo di Bologna, l'università più antica del mondo, eppure così moderna nell'insegnarci ancora oggi il valore universale della difesa dei diritti, la tutela della libertà, ma anche il diritto allo studio; quel diritto che Patrick stava esercitando da ricercatore e che gli è stato negato la notte tra il 6 e il 7 febbraio dell'anno scorso, quando è stato arrestato all'aeroporto del Cairo, accusato dal Governo egiziano di diffondere notizie false attraverso i suoi canali *social* e di attentare alla sicurezza nazionale. Fino a quel momento Patrick era un giovane senza confini, un figlio del mondo, esattamente come i tanti nostri ragazzi e ragazze che ogni anno partono per ampliare il proprio sapere e la propria conoscenza. Noi oggi qui chiediamo che Patrick possa tornare ad esserlo. Chiediamo che il Governo italiano si prodighi nei confronti dell'Egitto per lasciarlo studiare in Italia, libero di imparare e libero di scegliere come vivere la sua vita. Al tempo stesso, chiediamo che l'Egitto fornisca finalmente chiarimenti sulla vicenda dell'altro nostro giovane ricercatore italiano, a sua volta arrestato dalla polizia egiziana in modo del tutto immotivato e poi purtroppo brutalmente ucciso: Giulio Regeni per il quale non si conosce ancora la verità sull'ignobile fine che gli è stata riservata. Il destino dei ragazzi è per forza di cose intrecciato ed entrambi ci stanno profondamente a cuore. Consapevoli delle riflessioni che adesso ci ha appena riferito la vice ministra Sereni, crediamo però che conferire la cittadinanza italiana onoraria a Patrick Zaki sarebbe un chiaro segnale alle autorità egiziane, un modo per attribuire più forza alle nostre istituzioni nella pretesa di rilascio di Zaki e nella richiesta di verità sul caso Regeni. Riteniamo che sarebbe non soltanto un fatto simbolico, ma anche uno strumento oggettivo attraverso il quale rendere più facile l'assistenza legale al ragazzo. Patrick è in stato di detenzione preventiva dal giorno del suo arresto, oltre un anno fa, senza che ci siano motivi fondati; i reati imputati a Zaki si riferiscono in realtà a legittime attività di denuncia o di normale commento critico. Fino a oggi non è mai stato avviato un processo a suo carico, anzi gli si rinnovano i giorni di carcerazione, quarantacinque giorni di carcerazione di volta in volta; e purtroppo la custodia cautelare - come avvenuto per molti altri attivisti prima di lui - può essere rinviata in modo indefinito, al punto che il rischio è che Patrick rimanga in carcere ancora a lungo, fino addirittura all'ergastolo. Ecco perché questa mobilitazione corale a favore del conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, e dunque a favore della sua liberazione, è così importante. Le accuse che gli vengono rivolte sono le stesse per le quali sono state incarcerate persone che svolgevano attività del tutto legittime secondo il diritto internazionale; accuse usate ad arte in Egitto in questi anni per arrestare centinaia di attivisti, ricercatori, avvocati, esponenti di organizzazioni per la tutela dei diritti umani. Ecco che con questa mozione indirettamente chiediamo all'Egitto anche il rispetto dei diritti umani per i tanti prigionieri detenuti ingiustamente nelle loro carceri, attraverso la loro liberazione, perché sappiamo che purtroppo sono in tanti in Egitto a essere nelle stesse condizioni. Lì la libertà di pensiero viene repressa e troppo spesso si calpestano i diritti di chi osa esprimere il proprio dissenso, attraverso l'arresto. Questa mozione vuole dunque essere anche un segnale di solidarietà nei confronti di coloro che vengono trattenuti in carcere senza motivo, magari solo perché sospettati di fare parte di movimenti che si battono a difesa dei diritti umani.

proprio per favorire il rilascio di Patrick Zaki. Un ringraziamento speciale va ai funzionari della Farnesina, sia a Roma che a Il Cairo, che si stanno prodigando per essere vicini e di aiuto già oggi, in questa fase di arresto, al giovane Patrick Zaki. Nell'esprimere questi ringraziamenti, a nome del mio Gruppo annuncio il nostro voto favorevole alla mozione che ci apprestiamo a votare. Chiediamo al Governo italiano di spendersi per il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Chiediamo il massimo impegno nel continuare a chiedere, in tutte le sedi istituzionali, a partire da quelle europee, il suo rilascio. E contemporaneamente chiediamo anche il massimo impegno dell'Italia nell'ottenere finalmente la verità sulla morte di Giulio Regeni. *(Applausi)*. Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, la vicenda di Patrick Zaki

quattrocentotrentadue giorni per reati presunti e comunque di opinione; un attivista per i diritti umani e per i diritti civili in carcere illegalmente, senza prove, con accuse gravissime, soltanto per avere espresso le proprie idee e per avere difeso i diritti delle minoranze, i diritti civili e i diritti politici dei suoi concittadini. È un fatto gravissimo per il quale oggi, giustamente, il Senato si impegna a fare tutto ciò che è possibile al fine di ottenere la liberazione di questo giovane, come quella di tanti altri perseguitati, in Egitto e nel mondo. Parlando di Patrick Zaki, si riapre - come altri colleghi hanno ricordato - una ferita mai rimarginata, che è quella di Giulio Regeni, torturato e assassinato cinque anni fa, per il quale ancora l'Italia e il mondo libero intero attendono giustizia e giustamente condannano i depistaggi, l'ostruzionismo, l'omertà delle autorità egiziane. Tuttavia, colleghi, credo che una riflessione in più la dobbiamo fare e ringrazio il Governo per averlo sottolineato. Ci dobbiamo cioè chiedere se davvero il modo migliore per aiutare Patrick e ottenere l'obiettivo principale, prioritario e assoluto che tutti ci dobbiamo proporre, e cioè la sua liberazione

dice che l'Italia può concedere la cittadinanza italiana a uno straniero in due soli precisi casi: qualora lo straniero abbia abbia svolto eminenti servizi a favore dell'Italia, oppure quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato. L'esempio che mi viene in mente è quello dei due ragazzi, Adam e Ramy, che nel 2019 riuscirono a sventare con grande coraggio il dirottamento di un bus, salvando la vita probabilmente a decine e decine di loro coetanei. In quel caso, certamente c'erano i presupposti per conferire la cittadinanza a quei due giovani, e noi,

sia utile conferirgli la cittadinanza italiana e se non sia un atto di provocazione nei confronti dell'Egitto che potrebbe avere l'effetto di irrigidire le autorità egiziane anziché di favorirne la liberazione. Lo

il paradossale risultato di confermare l'Egitto e l'autorità giudiziaria egiziana nei loro sospetti. Questo è il rischio che corriamo. La strada giusta - a nostro parere - era un'altra e lo voglio dire chiaramente:

La via giusta è stata, come è stata, quella di mobilitare il Parlamento europeo, di chiedere ed ottenere l'intervento delle Nazioni Unite, Unite, di appellarsi - come si dice nella mozione purtroppo ritirata - alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984. È un lavoro certamente più difficile, che dà meno spazio sui *media*, sui *media*, forse meno adatto a procurare consenso facile, ma certamente - a nostro avviso - molto più utile all'obiettivo di liberare questo ragazzo. Desidero qui ringraziare sinceramente il Governo per la comunicazione che oggi ci ha fatto, perché è precisa, puntuale e responsabile, che tiene davvero conto del contesto, non propagandistica, ma volta all'unico obiettivo utile che vogliamo realizzare. Ringrazio il Governo per l'impegno che ha sempre profuso a difesa di Patrick Zaki; per l'impegno che ha sempre profuso per ottenere la verità e la giustizia per gli assassini di Giulio Regeni. Ringrazio, a nome di Fratelli d'Italia, le nostre rappresentanze diplomatiche a Il Cairo, che hanno tenuto sempre alta l'attenzione sulle fasi processuali che hanno riguardato i continui rinvii della liberazione di Patrick e le continue conferme della detenzione preventiva, che in realtà è una vera e propria pena, molto grave, e non c'è nulla di preventivo in questo. Voglio anche

È giusto battersi per Patrick, ma è giusto battersi anche per tutti gli altri milioni di casi nel mondo di persone nelle stesse condizioni di Patrick.

Pensiamo, cari colleghi, a quello che succede a Cuba, perché fra poco voteremo una mozione encomiastica su Cuba, nella quale non c'è una sola riga dove si condanna la violazione dei diritti umani, civili e politici in quel Paese, Vergogna! Cari colleghi, queste sono le ragioni per cui noi, a malincuore, ci vediamo purtroppo costretti ad astenerci sull'ordine del giorno presentato unitariamente dalle forze politiche di maggioranza.

penso che si debba partire con un giusto ringraziamento a chi ha voluto promuovere l'ordine del giorno in esame, con un lavoro di confronto all'interno delle forze di maggioranza, a dimostrazione

Quando parli di Zaki parli delle centinaia di migliaia di persone i cui diritti umani, non solo in Egitto, ma in molti Paesi, non vengono rispettati. Parli dei casi di violazione, di uso della forza esagerato, di vera e propria tortura e di maltrattamenti. Ed è chiaro che,

Ma il contraltare è che il caso diventa simbolico anche per quei Paesi che invece non rispettano i diritti umani e tendono a irrigidirsi, evidentemente, davanti a casi di questo genere. Quindi, per la diplomazia e per i Governi è davvero complicato conciliare quei due principi che si scontrano spesso nella politica internazionale: la battaglia per i diritti civili e i diritti umani - una battaglia universale - e, dall'altra parte, il principio di sovranità che tende a chiudere i confini e a non rispettare quei diritti umani. Ci troviamo in una situazione davvero complicata e difficile come Governo che crede in quei diritti, crede nella tutela dei diritti umani, si batte e fa un lavoro straordinario. Noi l'abbiamo fatto a tutti i livelli, perché lo abbiamo fatto come società civile italiana, a partire dal Comune di Bologna, che ha abbinato - questo è il messaggio importante - il caso di Patrick Zaki a quello di Regeni, a dimostrazione che non facciamo distinzione fra cittadini italiani e cittadini che vengono da storie diverse. Per noi la battaglia dei diritti umani si fa a tutte le latitudini e la facciamo anche nei confronti dei Paesi amici, con cui c'è un lungo e consolidato rapporto. Quando c'è stato il caso di George Floyd, ucciso da un poliziotto americano, noi siamo intervenuti e l'abbiamo detto chiaramente: siamo un Paese amico degli Stati Uniti, ma allo stesso tempo - perché siamo amici e c'è un rapporto consolidato - ci sentiamo in dovere di denunciare quando alcuni dei diritti più elementari non vengono rispettati.

nelle sedi europee. Ricordo il passaggio in Parlamento europeo quando abbiamo richiamato l'esigenza della liberazione di tutti gli attivisti che in Egitto manifestano per la libertà di espressione, per la libertà di stampa e di orientamento sessuale; tutte quelle libertà che sono scolpite nella nostra Costituzione e nella Carta europea Lo abbiamo fatto alle Nazioni Unite il 12 marzo del 2021, quando insieme ad altri Paesi, Stati Uniti compresi, abbiamo richiamato la necessità di rilasciare tutti i prigionieri politici, tutti gli attivisti, coloro che si battono per i diritti umani in Egitto.

tutti i passaggi. Siamo mobilitati al massimo grado e a tutti i livelli. Perché anche la richiesta di cittadinanza? Come dicevo prima, ha assunto un valore simbolico la vicenda di Patrick Zaki e noi abbiamo voluto dire in maniera molto chiara che non facciamo distinzioni, a prescindere dalla cittadinanza. Allora, preannunciando la mia dichiarazione di voto, in cui esprimerò il voto favorevole delle donne e degli uomini del Partito Democratico, voglio fare due considerazioni: la prima è che questa deve essere una battaglia culturale, prima ancora che politica. Noi ci muoviamo in un quadrante complicato e difficile come quello del Mediterraneo orientale, dove è inevitabile mantenere canali di cooperazione con la Turchia e l'Egitto; un territorio fondamentale per la stabilità e la sicurezza dell'Europa e del nostro Paese, dove Turchia ed Egitto sono *partner* fondamentali nel lottare contro il terrorismo di matrice islamica e nel colpire il traffico di esseri umani e armi. Da e armi. Da questo punto di vista un canale di dialogo va tenuto aperto dal Governo. Allo stesso tempo questo non ci può e non ci deve impedire, soprattutto a livello parlamentare, di mettere in campo un'iniziativa molto forte a tutela dei diritti umani. È evidente che si scontra - come dicevo prima - quella dialettica complicata e difficile che noi viviamo giorno per giorno tra il rispetto della sovranità e delle scelte dei singoli Paesi e una battaglia universale come quella sui sui diritti umani, ma questo non ci deve far retrocedere. Abbiamo il dovere di andare avanti e fare questa battaglia soprattutto all'interno delle Aule parlamentari. C'è un cambiamento notevole rispetto al passato, in quanto la vittoria di Biden negli Stati Uniti apre una nuova fase nel Lo dico perché il rischio che alcune declamazioni sul rispetto dei diritti umani da parte dei Paesi europei finiscano per essere velleitarie è concreto e diciamocelo chiaramente senza ipocrisie. Avere gli Stati Uniti accanto è fondamentale e abbiamo visto il cambio di passo tra l'Amministrazione americana a guida Trump e quella a guida Biden: Trump impostava i rapporti, soprattutto a livello bilaterale, su logiche di forza, mentre con Biden si torna al metodo multilaterale e ciò è sicuramente un passo in avanti notevole. Il richiamo che il Presidente americano ha fatto alla comunità delle democrazie liberali aiuta a perimetrare il campo e avere alle spalle dell'Europa gli Stati Uniti che tornano così a garantire non solo la a garantire non solo la sicurezza internazionale, ma anche il rispetto di alcuni valori fondamentali delle democrazie liberali, come le libertà di espressione, di stampa e di orientamento sessuale, che sono scolpite

del Golfo, con lo stop e la sospensione di alcune forniture di armi perché impegnati a bombardare delle comunità dello Yemen senza *standard* minimi di rispetto dei diritti umani, la dicono lunga sul segnale

quando tre attivisti dell'organizzazione non governativa a cui aderisce Patrick Zaki avevano avuto l'ardire di incontrare 13 diplomatici europei (alla fine sono stati rilasciati). Blinken ha preso una posizione molto forte, dicendo che non è un crimine incontrare dei diplomatici europei. Si apre quindi una nuova fase, favorita anche dall'ascesa della nuova *leadership* americana,

il Patto atlantico è nato non solo con l'esigenza di garantire la stabilità e la sicurezza del nostro Continente, ma anche per mettere insieme una comunità che condivideva valori e principi comuni. Ci dobbiamo muovere dentro questo sentiero stretto. Condividiamo la mozione proposta dal collega Verducci, con la consapevolezza, attingendo alla tradizione, alla storia e alle nostre origini, che, come scritto nel Talmud, «Chi salva una vita salva il mondo intero». Penso che a questo dobbiamo fare sempre riferimento quando ci battiamo per i diritti umani. Grazie i colleghi Verducci e Montevecchi e tutti coloro che hanno contribuito in modo sostanziale a promuovere una discussione su una questione che ci sta a cuore e che - come dimostra anche il dibattito di oggi - è trasversale alle forze politiche. Il tema ci sta cuore perché parliamo della storia di Patrick

del filo che unisce noi a lui e che lui stesso sente sul piano della sua appartenenza, che vorrei dire doppia in quanto non solo al suo Paese d'origine, ma anche al nostro.

così come la storia di Giulio Regeni non era e non è quella di un ragazzo ammazzato ingiustamente. Se la derubricassimo a una vicenda di singoli, non ne capiremmo la natura e non riusciremmo ad affrontare nel migliore dei modi una discussione delicata che investe più piani. È la storia di un Paese, il nostro, che, come dicevo, ha accolto lo studente Zaki e sente Patrick come suo figlio, addirittura da chiederne, come stiamo facendo oggi, la cittadinanza italiana. Tuttavia è una storia di relazioni tra Paesi e di relazioni diplomatiche in difesa dei diritti umani.

ma dobbiamo essere consapevoli del ruolo e della funzione di un Paese come il nostro nel mondo, a tal punto da pretendere la difesa e il rispetto di diritti civili e dei diritti umani, quando questi non dovessero essere rispettati da altri Paesi, anche da quelli con cui intratteniamo

un passaggio come quello odierno, che deve far sentire tutta la solennità di questo strumento, non è semplicemente un atto di indirizzo, l'espressione del Parlamento italiano che chiede la cittadinanza italiana per un ragazzo che è stato imprigionato, torturato e ingiustamente detenuto, che non può avere diritto a un processo e che non ha contatti con il resto del mondo. Se non lo prendiamo da questo punto di vista, il passaggio odierno non è la votazione su una mozione o su un atto di indirizzo, ma diventa una mozione degli affetti una mozione degli affetti di cui possiamo farci ben poco sul piano della risoluzione dei problemi, ma soprattutto della possibilità di mettere al centro le grandi questioni di cui stiamo discutendo. Questa non è semplicemente la storia di un ragazzo,

richiedere misure restrittive per i funzionari egiziani responsabili di violazioni più gravi, perché l'impunità non può essere un elemento sostenibile sul piano democratico; non possiamo considerare democrazia un Paese che mette al riparo i suoi aguzzini, che si macchiano di reati gravi come quelli di cui stiamo discutendo. In secondo luogo, la risoluzione denuncia il tentativo da parte dell'Egitto di ostacolare le indagini su Giulio Regeni. È stato ricordato anche questo aspetto: la vicenda di Patrick Zaki è legata a doppio filo con quella di Giulio Regeni,

dei diritti umani. In questo senso, il nostro lavoro non è una mozione degli affetti, ma un lavoro tutto politico, che vuol dire diplomatico, perché investe la sfera dei rapporti tra i Paesi,

subordinando quindi la cooperazione al suo rientro nella Convenzione di Istanbul. Ne abbiamo discusso poco tempo fa. È un rapporto che dobbiamo stabilire con i Paesi verso i quali non abbiamo e non dobbiamo avere la pretesa di insegnare la democrazia, ma rispetto ai quali dobbiamo puntare i piedi e usare tutte le armi a disposizione per richiedere il rispetto dei diritti. In questo senso, signor Presidente, la domanda,

dove finisce la legittima volontà del nostro Paese di considerarsi amico dell'Egitto e di continuare a intrattenere relazioni commerciali e dove inizia,

arma piuttosto estrema, ma efficace, quella di immaginare persino il ritiro della missione diplomatica italiana in Egitto,

e non fornire - come non dovremmo fare, se vogliamo essere coerenti - commesse militari all'Egitto? Ci sono contraddizioni che ci riguardano, che investono il Governo e il nostro Parlamento e di cui dobbiamo sentire la responsabilità,

la questione che oggi ci troviamo a discutere in quest'Aula rappresenta l'essenza del nostro vivere le istituzioni democratiche e plasma il modo stesso di concepire le relazioni internazionali e la nostra presenza sullo scenario internazionale. Libertà e diritti umani non conoscono frontiere o colore politico, né sono orpelli da utilizzare alla bisogna, nelle varie contingenze, nella polemica politica o nel conflitto tra Nazioni, sono un patrimonio dell'umanità che, dichiarazioni e convenzioni a parte, riteniamo eticamente vincolante e su cui non ci possono essere distrazioni o compromessi. La vicenda di Patrick Zaki, che si protrae da oltre un anno, ha scosso le coscienze in tutto il mondo, o meglio in quella parte del mondo libero, l'Occidente, di cui siamo parte integrante, non solo per ragioni geografiche, quanto per appartenenza culturale e valoriale. Ha scosso ancor più il nostro Paese, l'Italia, in cui il giovane Zaki studiava e aveva trovato i suoi affetti. Nell'affrontare questa discussione e il voto che esprimerà il Parlamento sul testo al nostro esame, è necessario precisare che non si tratta di aprire l'ennesimo fronte di conflitto con le autorità egiziane, dopo la tragica vicenda di Giulio Regeni, che - lo dirò anch'io - ancora reclama verità. Si tratta di ribadire l'inviolabilità, ad ogni latitudine del globo, dei diritti umani riconosciuti a ogni singolo uomo. Personalmente - spero non si scandalizzino le anime belle - non contesto il diritto di un Paese sovrano, al di là della sua forma di Governo, di giudicare un suo cittadino. Contesto, come sancito dalla Carta dei diritti dell'uomo, che a un individuo possano essere sospesi i propri diritti inalienabili, specie in virtù delle sue opinioni politiche; pertanto, il procedimento giudiziario dev'essere giusto - è tale, se lo è anche nei tempi - e privo di discriminazioni. Constatiamo che Zaki si trova a vivere una vicenda giudiziaria non limpida, non trasparente e non giusta. Privato dei suoi legittimi diritti di difesa - di un giusto processo, diremmo noi - subisce una detenzione a tratti umiliante per la sua persona. Ricordo che Marco Pannella non perdeva occasione per ricordare e ricordarci che «dove vi è strage di diritto, vi è strage di popoli». È questo e non altro, onorevoli colleghi, il tema su cui soffermarci e su cui siamo chiamati a fare una battaglia politica. Non pensate, pur nella bontà delle vostre idee, che possiamo entrare nel merito della natura dei tanti Paesi che, dal Mediterraneo al Medio Oriente, passando per l'Estremo Oriente, presentano caratteri e forme di Governo a-democratiche. Siamo chiamati a difendere i valori sanciti nelle Convenzioni internazionali, base riconosciuta della nostra civiltà, che rappresentano la base naturale del nostro ordinamento costituzionale e della Repubblica. Possiamo e dobbiamo farlo, agganciando le nostre relazioni e lo sviluppo dei nostri rapporti economici e diplomatici al rispetto dei diritti umani e alla liberazione dei prigionieri politici. Dobbiamo farlo tanto con i Paesi che consideriamo deboli, come con quelli forti, ivi compresa la Cina, su cui molti degli stessi urlatori della difesa dei diritti umani nel Mediterraneo perdono poi la voce, pronti ad applaudire le nuove vie della seta, dimenticando la persecuzione religiosa di musulmani, buddisti, Falun gong e cristiani, perpetuata in questi anni da Pechino. Non dimentichiamo la nostra storia e le conquiste di civiltà di cui il nostro Paese è stato interprete. Infatti, nel passato l'Italia ha avuto la forza politica e istituzionale di difendere i diritti dei popoli oppressi in ogni dove, anche di fronte all'alleato americano. Forse qualcuno di voi, credo pochi, ricorderà le parole dell'allora presidente del Consiglio, Bettino Craxi, al Congresso americano, sulla repressione cilena. Dobbiamo poi difendere e subordinare al rispetto dei diritti umani non solo nel caso Zaki, ma anche quando siamo chiamati a determinarle e svilupparle, le politiche comunitarie. ho provato forte imbarazzo, lo scorso dicembre, quando è stato siglato l'accordo commerciale tra l'Unione europea e la Cina. Dovevamo pretendere che il rispetto dei diritti umani basilari fosse una parte importante di quell'accordo, approvato al *fotofinish* dalla presidenza tedesca, anche non tenendo in considerazione i dettami del Parlamento europeo. I risultati li abbiamo visti la scorsa settimana, con un gruppo di rappresentanti e parlamentari europei sanzionati da Pechino. È quindi questa l'occasione, onorevoli colleghi, di affrontare i nodi e i capisaldi intorno a cui ricostruire la nostra politica estera. Personalmente ho accolto con piacere le parole da *realpolitik* del presidente Draghi sui nostri rapporti internazionali necessari e la franchezza con cui, però, ha chiamato le cose con il loro nome. Credo e spero che questa formula istituzionale di emergenza nazionale possa servire per resettare alcuni sbandamenti del recente passato, riannodare il nostro legame atlantico, rilanciare una nostra presenza indispensabile nell'area del Mediterraneo allargato, dove ancora si giocano gli equilibri mondiali. L'Egitto, verso il cui popolo nutriamo sentimenti di grande amicizia, al pari di tante altre realtà della sponda Sud, è stato e può ritornare a essere - nella chiarezza dei rapporti e nel rispetto di quei diritti fondamentali che ho richiamato - un *partner* affidabile dell'Italia per la stabilizzazione dell'area e per lo sviluppo di feconde relazioni. Credo che l'ordine del giorno in discussione, per avviare tempestivamente, mediante le competenti istituzioni, le necessarie verifiche al fine di conferire a Patrick Zaki la cittadinanza italiana, possa essere un modo per porre l'attenzione sulla questione (che, mi permetto di dirlo, è una delle tante che si consumano in silenzio e tra l'indifferenza dei più in molte parti del mondo). e consentitici, pur tuttavia, di essere fortemente scettici che questa possa essere la strada che porti alla liberazione di Zaki e alla soluzione della sua vicenda; anzi, il nostro timore è che possa innescare un nuovo e più alto contenzioso giuridico sulla vicenda, esasperare i toni e gli animi e prolungare l'ingiusta detenzione di Zaki, alla cui condizione vogliamo dare una risposta e non già fare crociate sulla sua pelle. È una perplessità che condividiamo con la vice ministra Sereni e con il collega senatore Balboni, che però vogliamo mettere agli atti, non solo a futura memoria, ma perché abbiamo il dovere di abbandonare la retorica imperante, che, specie sui temi di politica estera, ha già fatto tanti danni all'Italia. Do atto al Governo, in questa particolare occasione, di averlo fatto. Non si possono infatti sostituire una buona e autorevole politica estera e l'azione politica e diplomatica di un grande Paese, come l'Italia dev'essere, con *escamotage* giuridici. Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, ritengo altresì che quella indicata nel testo, ossia sollecitare il Ministero degli affari esteri e le sue articolazioni a sviluppare ogni ulteriore iniziativa diplomatica che porti al più presto alla risoluzione della vicenda, sia la strada migliore e quella suscettibile di portare maggiori risultati. Sottosegretario, abbiamo particolarmente apprezzato il pragmatismo e anche la sua descrizione molto corretta dei fatti e dei rischi che si possono prefigurare, anche all'esito di questo nostro dibattito, rispetto alla alla persona stessa di Patrick Zaki, ma anche a chi come lui, in Egitto o in altri Paesi, vive in situazioni di costrizione e di mancato rispetto della libertà.

E lei, signor Sottosegretario, a nome del Governo ha molto correttamente precisato che lo stesso esito auspicato dall'ordine del giorno, che tutti ci accingiamo a votare, può produrre un effetto distorsivo rispetto ai presupposti di soccorso per i quali esso è stato presentato. Mi riferisco al fatto che il Governo egiziano potrebbe leggere come provocazione la concessione della cittadinanza italiana per le motivazioni - che ben conosciamo - inserite nella legge. Dobbiamo essere molto determinati nel fare rispettare i diritti umani e nel pretendere che le istituzioni internazionali, che dovrebbero essere preposte a farli rispettare, facciano la loro parte fino in fondo, evitando in ogni caso l'errore di considerare questa come un'azione bilaterale tra l'Italia e un altro Paese:

Penso innanzitutto alle istituzioni europee, all'Alto commissariato per la politica estera europea, ma certamente anche all'Organizzazione delle Nazioni Unite, che purtroppo - e dico tre volte purtroppo - appare totalmente evaporata.

si intravede, in maniera netta e stagliata, la figura di Regeni e quanto ancora oggi quella ferita sia aperta. È altrettanto indubbio, però, che il tutto non può essere ricondotto - lo ribadisco - a un rapporto tra l'Italia e l'Egitto.

la Farnesina e come ben devono fare i nostri rappresentanti all'estero, affinché l'esito di tutto ciò sia la liberazione di Patrick Zaki. Mi permetterei di correggere quanto inserito nell'ordine del giorno, non prevedendo semplicemente (come si legge al punto 4)

Certo che sì, ma - bontà di Dio - di tutto abbiamo bisogno, fuorché che la spinta dell'opinione pubblica deformi l'obiettivo finale, facendo sì che dall'altra parte ci sia un irrigidimento di posizioni tale per cui, al contrario, quello che andrebbe definito in maniera molto chiara tutt'altro che una democrazia, ossia un regime, voglia invece dare una dimostrazione muscolare alle spalle proprio di Patrick Zaki e delle organizzazioni che si battono in Egitto per garantire i diritti e la libertà delle persone. Abbiamo bisogno che tutto questo sia fatto in maniera intelligente dalla Farnesina. Abbiamo bisogno di sapere - cosa di cui siamo certi - che già ci stiamo muovendo in maniera intelligente, affinché non ci si trovi di fronte a un ulteriore caso Regeni, sapendo bene che ad ogni azione corrisponde una reazione proporzionale e inversa e che, se ci avventuriamo in dichiarazioni di un certo tipo, o facciamo seguire prese di posizione conseguenti oppure andremo incontro a una nuova frustrazione, per cui la politica estera italiana e il nostro Paese ne risulteranno ulteriormente indeboliti, alle spalle, per di più,

non di un nome e di un cognome. Tanti Patrick Zaki, infatti, in tanti altri Paesi, nel mondo e in Egitto, subiscono le stesse condizioni senza avere avuto

livello di privazione di libertà. Dobbiamo pertanto, tenerci sempre su valori importanti. Occorrono prese di posizione e credo lo stiamo facendo nella maniera più corretta, come il Governo prima ha delineato. Occorre anche avere consapevolezza che in questi dibattiti non ci si può limitare a un semplice ordine del giorno o a una risoluzione approvata in Senato, ma - ripeto - le istituzioni internazionali preposte

che ciò che abbiamo come obiettivo è la liberazione della persona e che siano rispettati i diritti umani in Egitto e negli altri Paesi nei quali non lo sono, con o senza cittadinanza. Non vogliamo infatti che quella cittadinanza italiana che non fu in grado di proteggere Regeni sia oggi un ulteriore fardello sulle spalle di Patrick Zaki.

Sono trascorsi quasi quindici lunghissimi mesi dal giorno in cui fui raggiunta dal messaggio di una docente dell'Università di Bologna che mi segnalava l'arresto di Patrick e mi chiedeva di attivarmi. In quel momento, ho sentito subito il dovere e la responsabilità di attivarmi e l'ho fatto - come dicevo - insieme ai miei colleghi della Commissione diritti umani per iniziare a seguire questo caso, quando ancora non era noto al mondo. vero che tutti i casi vanno seguiti, anche se non noti al mondo, perché ogni singola libertà va difesa, al di là del clamore mediatico che la circonda.

tendono inevitabilmente a rendere sfumata la nostra percezione dell'importanza di diritti astratti come quelli umani e civili. Essi, invece, insieme alla protezione dei loro difensori sono fondamentali, perché ci parlano della nostra libertà di esprimere le nostre idee,

infatti, non ha un figlio, un fratello, un fidanzato o un marito studente, ricercatore o difensore di questi diritti?

come lo era Giulio Regeni. Si tratta di un caso paradigmatico del pericolo e della deriva che stiamo vivendo a livello internazionale sulla libertà di essere studenti e ricercatori, di perseguire liberamente i propri filoni di ricerca e le proprie idee e di fare liberamente le proprie battaglie.

noi potremmo ritrovarci nelle condizioni dei genitori di Giulio Regeni. È perciò importante portare in Aula questi temi fondamentali e queste questioni, che siamo chiamati non solo ad affrontare, ma a risolvere.

sono incubatori di idee e di cambiamento come solo i giovani studenti e i giovani ricercatori sanno essere. E quegli incubatori di cambiamento e di idee non possono che portare beneficio anche a tutti noi e alla nostra società, perché di quei cambiamenti positivi beneficeremo tutti noi, non solo chi li avrà prodotti. Perciò è importante essere qui oggi a difendere un cittadino egiziano studente di un'istituzione prestigiosa come l'Università di Bologna. Grazie all'università per tutta la mobilitazione e a tutti i Comuni d'Italia che hanno voluto riconoscere

è da quasi quindici mesi in detenzione cautelare, in attesa di avere un processo per i capi di accusa che gli sono contestati; è in attesa di avere un processo. In una lettera dicembre 2020, Patrick già lamentava condizioni psicofisiche molto deteriorate e anche recentemente abbiamo notizia sua vita faticosa all'interno di un carcere di massima sicurezza, dove sono incarcerate altre persone come lui, con gli stessi capi d'accusa, anch'esse in attesa di un processo.

di alto valore simbolico nei confronti di questo ragazzo e di tutte le persone che si trovano nella sua condizione. La situazione di Patrick va inquadrata in un contesto internazionale e globale di deriva nei confronti dei diritti umani e delle libertà civili, ma noi ci siamo voluti spingere un po' oltre: un po' oltre: innanzitutto, dobbiamo batterci e chiedere, come sta facendo la nostra diplomazia, che sia ripristinato il monitoraggio processuale internazionale, al quale l'Egitto non può sottrarsi. Poi dobbiamo spingerci oltre e chiedere che sia valutata la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti messi in campo dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984. Questa è la via procedurale e giuridica per intraprendere un percorso pacifico e arrivare a una soluzione del problema attraverso una negoziazione. È inoltre molto importante un altro impegno che abbiamo chiesto di inserire e che è confluito in quest'ordine del giorno (e ringrazio il senatore Verducci, la senatrice a vita Liliana Segre e tutte le forze politiche che lo hanno voluto sottoscrivere):

seguente motto: persone, pianeta e prosperità. I diritti umani e le libertà individuali, in questa prospettiva, non sono dunque negoziabili e l'Italia dev'essere promotrice di una riflessione sul rispetto dei diritti umani in questo consesso, che nasce nel segno di tali principi e obiettivi. Ricordiamolo di nuovo: persone,

ancora si dovesse chiedere, dopo questo mio intervento, perché siamo qui oggi, ricordo una frase estratta dal film «Milk»: «Se non ti mobiliti per difendere i diritti di qualcuno che in quel momento ne è privato, quando poi intaccheranno i tuoi, nessuno si muoverà per te. E ti ritroverai solo». Oggi perciò votiamo a favore di quest'ordine del giorno, che - lo ricordo al senatore Balboni

in questi giorni ha consegnato all'interno di un romanzo, che è un monumento della letteratura mondiale, «Cent'anni di solitudine» di Márquez, un messaggio scritto in un italiano un po' zoppicante: «Anchora resetendo.

e non ci sposteremo di un millimetro fino alla tua liberazione.

Si è così conclusa la discussione sulle mozioni sulla concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki e sulle iniziative per la sua liberazione. I lavori dell'Assemblea riprenderanno alle ore 15,30. La seduta è sospesa.

di reclusione per corruzione. Questo è un fatto gravissimo che cancella un percorso per il quale la mia forza politica si è battuta per anni e che va contro la delibera

quest'argomento è molto all'ordine del giorno

spiego anche il motivo. È evidente che ieri, come abbiamo tutti appreso dalle agenzie di stampa, c'è stata una decisione della giurisdizione interna del Senato della Repubblica

il Consiglio di garanzia, per l'aspetto giurisdizionale, e il Consiglio di Presidenza per gli aspetti deliberativi, tanto è vero che si discute di delibere prese dal Consiglio di Presidenza. Pertanto, il merito di questi argomenti, per la loro rilevanza, va discusso in queste sedi. Naturalmente la Presidenza non può che prenderne atto

la questione dei vitalizi restituiti a due persone condannate, come dice lei, ha avuto la sua genesi in organismi giurisdizionali, tuttavia mi permetto di dissentire circa il fatto che la questione sia meramente giuridica. In un momento come quello attuale, in cui una pandemia ha messo in ginocchio l'intero Paese, in un popolo che sta manifestando e la rabbia comincia a crescere perché c'è una crisi economica che morde fortissimo, un segnale come quello verificatosi in questi giorni, cioè la restituzione con gli arretrati e anche con gli interessi, dei vitalizi a persone condannate, che quindi hanno rubato alla collettività (uno è condannato per corruzione e l'altro anche per fatti gravissimi che hanno danneggiato la collettività) è qualcosa che può far esplodere la rabbia sociale, ancora di più rispetto a quello che abbiamo visto nei giorni scorsi. Pertanto, la questione non è meramente giuridica, ma è politica e se ne deve discutere in questa sede. Chiedo quindi che si trovi il modo di parlarne e di superare questo *vulnus* evidentissimo all'eguaglianza e all'equità sociale *(Applausi)*.

di cui non a caso fanno parte gli esponenti di ciascun Gruppo. In ogni caso l'argomento ha una sua rilevanza, e ora possiamo procedere oltre con la trattazione del punto all'ordine del giorno.

di Roma Capitale, e quindi con la presa di Porta Pia il 20 settembre 1870. Le celebrazioni ovviamente riguarderanno il biennio 2020-2021. Rispetto alle ragioni di una mozione come questa,

di molti parlamentari, alcuni dei quali eletti a Roma ma non solo, che da due anni cercano in tutti i modi, con convegni, riflessioni e iniziative, di porre al centro dell'attenzione del Parlamento e delle istituzioni la questione che riguarda il ruolo, di Roma Capitale. Alla Camera - lo dico, ma molti colleghi lo sanno perfettamente - sono stati incardinati

pandemia; il Comune ha organizzato una serie di iniziative; vi è stata soltanto l'iniziativa di un concorso

di prestare una particolare attenzione, rilevando che anche le celebrazioni sono un modo per significare che il Governo e il Paese hanno a cuore la propria capitale.

purtroppo è una situazione assai imbarazzante. Sono ormai vent'anni che parliamo di forme di adeguamento della capitale d'Italia alle altre capitali europee e non si è fatto nulla. Grazie a Dio c'è questo osservatorio trasversale, che sta discutendo in modo concreto non di dare più poteri alla capitale d'Italia, ma di renderla adeguata alle sfide, non solo dell'oggi, ma anche del domani. Gli inglesi lo hanno fatto con The Greater London Authority, con cui hanno reso autonoma la città di Londra. È stato fatto per Berlino, capitale da poco più di venti anni, che stata elevata al rango di *Land*, quindi con pieni poteri legislativi, tutti finalizzato allo sviluppo della città capitale

una fase di profonda metamorfosi, perché si rendono conto di quanto sia difficile governare una comunità, ma abbiamo visto fotografie della sindaca della capitale d'Italia, con degli alberi potati o con un manto stradale rifatto: non la critico, ma ciò dà la dimensione della coscienza e della consapevolezza del ruolo che si occupa. Non è stata tradita la fiducia dei cittadini, ma si è semplicemente inadeguati.

di chi fa il sindaco della capitale d'Italia ed è ridicola. Non è colpa della sindaca Raggi: sono tante altre le sue responsabilità. Ho letto stamattina che ieri è stata salvata, perché non ha la maggioranza in consiglio comunale: neanche il presidente Conte ce l'aveva e si è dimesso. Sarebbe utile, come ha chiesto l'UDC a Roma, che la sindaca Raggi ne prendesse atto e che almeno il 20 Giugno si dimettesse, dando finalmente luogo a un commissariamento della capitale d'Italia.

a Roma non si è mai fatto nulla. Lo dico come esponente politico che è stato anche avversario di chi ha governato per tanti anni la capitale d'Italia: le ultime opere pubbliche o le ultime opere che hanno dato una prospettiva alla città, le abbiamo inaugurate venti anni fa. all'auditorium o al sottopasso di Castel Sant'Angelo: non le ho certamente inaugurate come amministratore di maggioranza, ma ne rendo atto. Qual è l'ultima opera pubblica inaugurata in questa città? Non c'è niente! Sono vent'anni che non si costruisce il futuro di Roma. Sono vent'anni che non si va a costruire un'opera pubblica, che dia una maggiore fruizione e una maggiore prospettiva. Per concludere, mi auguro che questa non sia l'ennesima occasione in cui si contempla e si esalta il ruolo di Roma, lasciando poi a Roma il destino di un qualunque Comune d'Italia.

culla del diritto, centro della cristianità, con 6.000 chilometri di strade, dove si stratificano tremila anni di storia, e sede di tre tipi di ambasciate (presso la Capitale, le organizzazioni internazionali e la Santa sede). Roma, che all'interno dei suoi confini vanta un museo a cielo aperto. Roma, che si estende su un territorio che potrebbe contenere otto delle principali città italiane e ben nove capitali europee: Amsterdam, Atene, Berna, Copenaghen, Dublino, Lisbona, Parigi, Vienna Bruxelles. Il centocinquantesimo anniversario della sua proclamazione come capitale d'Italia deve essere l'occasione per impegnarci tutti insieme, senza steccati ideologici e logiche di appartenenza partitica, affinché Roma torni ad occupare uno spazio importante nel contesto sia nazionale che internazionale. Roma deve riappropriarsi del suo fondamentale ruolo di traino economico e soprattutto culturale, che la storia le riconosce da sempre. Roma capitale da sempre. Roma capitale della cultura europea: non deve soltanto essere uno *slogan*, ma un impegno che oggi tutti noi dobbiamo prendere in quest'Aula votando la mozione. Roma, orma: restituire la giusta dignità che merita alla capitale d'Italia significa seguire - da orma - quella traccia che segna il giusto cammino, per far sì che questa città torni a essere grande nel mondo, ma allo stesso tempo capace di farsi piccola e prendersi cura di tutti i suoi cittadini, nessuno escluso. Una città che deve ambire a una maggiore autonomia di funzioni sia per governare il suo enorme patrimonio storico sia per la gestione efficiente di una macchina amministrativa così complessa. Roma, infatti, è una delle poche capitali che a livello mondiale non gode di una particolare autonomia.

stante il suo particolare *status*, non può essere governata in modo esclusivamente verticistico e centralizzato. L'esperienza amministrativa dimostra che, soprattutto in enti territoriali molto estesi, il decentramento puntuale e non generalizzato può essere la chiave per migliorare la qualità dei servizi al cittadino in termini di maggiore efficienza. E noi a questo teniamo, al bene dei cittadini. Ecco perché sarà necessario procedere a conferire ai municipi specifiche funzioni amministrative il cui esercizio risulti più efficiente la devoluzione a un ente di prossimità e riconoscere una maggiore autonomia finanziaria di spesa finalizzata all'erogazione dei servizi ai cittadini residenti. L'obiettivo in questo caso è incentivare l'azione amministrativa decentrata nei municipi (che in altri enti sarebbero città) attraverso il conferimento di nuove funzioni e il riconoscimento di maggiore autonomia finanziaria, quest'ultima anche quale meccanismo premiale della gestione virtuosa ed efficiente. Roma, amor, orma: la strada che ci porterà a una rinascita di questa città, la Città eterna, non può che essere incarnata nell'amore proprio per la città: Roma, amor, orma. Viva Roma!

ringrazio i colleghi senatori per aver posto la questione in oggetto con la mozione. Ricordo brevemente, *in primis* a me stessa, che sono state effettuate alcune celebrazioni centocinquant'anni di Roma capitale d'Italia: ricordo che nella legge di bilancio 2019 sono stati stanziati 500.000 euro, cui ha fatto seguito un bando del Mibact proprio per selezionare progetti da finanziare sulle associazioni territoriali. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport che mi ha preceduto ha costituito un tavolo tecnico di coordinamento al quale sono stati invitati i rappresentanti del Mibact, del Ministero dell'istruzione e di Roma Capitale. Il tavolo era coordinato dalla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e si è riunito tre volte. Il Ministero dell'istruzione ha promosso un concorso per gli studenti di ogni ordine e grado, «Tutte le strade portano a Roma», anche questo nell'ottica di ricordare ma altresì di includere i giovani, e Roma Capitale ha avviato le celebrazioni lo scorso 3 febbraio 2020 con un evento di apertura al Teatro dell'opera: c'è stata, in sede di Musei Capitolini, una *lectio magistralis* tenuta dal saggista e storico Paolo Mieli, alla quale ha partecipato una delegazione di giovani studenti. Da quando ho assunto le deleghe, ho avviato la ricostituzione della struttura di missione, alla quale, però, ho voluto anche dare una nuova forma. Quindi, accanto alle celebrazioni nazionali, vi è anche il coinvolgimento dei giovani, proprio in un'ottica partecipativa: ricordo e coinvolgimento dei ragazzi. È mia intenzione anche confermare il comitato che è stato nominato lo scorso dicembre, valutando la possibilità di allargarne la composizione. Ciò detto, per quanto riguarda la mozione in esame esprimo parere favorevole sulle premesse e sugli impegni, con una proposta di riformulazione degli impegni 4) e 5).

il punto 5) con il seguente: «a valutare, nel caso di insufficienti disponibilità del bilancio dello Stato, la possibilità, sulla base delle necessarie verifiche tecniche, di destinare in via del tutto eccezionale una quota parte degli incassi delle biglietterie dei principali siti archeologici e monumentali e dei musei della capitale alla celebrazione del 150° anniversario e alla realizzazione dei progetti individuati».

già nel marzo 1861 Cavour, in un discorso alla Camera del Regno d'Italia, affermava: «Tutta la storia di Roma, dal tempo dei Cesari al giorno d'oggi, è la storia di una città la cui importanza

Partendo da questa frase pensiamo al danno culturale per l'umanità che questa pandemia sta creando da un anno alla nostra capitale, privando anche i turisti di tutto il mondo della possibilità di godere della bellezza e della storia di Roma. Una volta mi colpì la frase di un ragazzo - e ringrazio la ministra Dadone per aver citato la partecipazione dei giovani e per aver proposto la riformulazione di quel punto della mozione

Ebbene questa mozione, a prima firma della collega De Petris, chiede di celebrare in maniera forte i centocinquant'anni della proclamazione di Roma Capitale. Certo, in questo anno non abbiamo potuto farlo come Roma e l'Italia avrebbero meritato e come è stato fatto per altri eventi, tra i ricordato nella mozione, del 2018, in occasione dell'anniversario della vittoria nella Prima guerra mondiale, con un evento finale al quale ha partecipato il Presidente della Repubblica. A questo proposito, ancora una volta mi piace ricordare l'impegno nel comitato per gli anniversari di interesse nazionale del senatore Marini, che purtroppo abbiamo perso da poco a causa del Covid-19 e che è stato autorevole presidente di questo Senato.

compiere una grande operazione culturale ed educativa, come la mozione chiede, con il coinvolgimento di centri studi, università pubbliche e private, associazioni culturali, terzo settore, sindacato, mezzi di comunicazione, aggiungendo adesso, su impulso della ministra Dadone, come ricordavo prima, come ricordavo prima, giovani e associazioni giovanili. Ma richiede anche un impegno straordinario per la riduzione dell'inquinamento e la realizzazione di un programma di opere pubbliche e di riqualificazione del tessuto urbano. Abbiamo le risorse del *recovery* e anche su questo dobbiamo impegnarci

All'altro ramo del Parlamento sono in corso le audizioni per l'*iter* di proposte di legge di intervento nella nostra Costituzione per ampliare il ruolo di Roma Capitale. Riteniamo che questo sia il momento. C'è un osservatorio - anche questo lo si ricordava - in cui sono presenti tutte le forze politiche per rilanciare il ruolo e le funzioni di Roma Capitale. È, dunque, questo il momento.

oggi discutiamo la mozione su Roma Capitale, che risale ad agosto 2020 e che è gemella di un'omologa mozione presentata alla Camera. Entrambe sono uno dei frutti e degli intenti trasversali, come è stato ricordato, del lavoro dell'Osservatorio parlamentare per Roma. L'oggetto è la ricorrenza dei centocinquant'anni dalla proclamazione di Roma a capitale. La data di riferimento è quella del 3 febbraio 1871, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia della legge n. 33, appunto del 3 febbraio 1871, che trasferiva la capitale da Firenze a Roma. Il 3 febbraio scorso, complice la pandemia e le note ristrettezze, le celebrazioni sono state ridotte e la ricorrenza è passata quasi inosservata,

una questione di celebrazioni, peraltro dovute, ma anche di sostanza e cercherò di spiegarlo. Potrei impiegare interamente i dieci minuti a mia disposizione

Come non ricordare alle origini la legge per Roma Capitale n. 396 del 1990 di Craxi e Andreotti, con relativi stanziamenti, definanziati purtroppo nel 2012. Mi piace Mi piace sottolineare che Roma Capitale entra nella Costituzione con la legge costituzionale n. 3 del 2001, che modifica il comma 3 dell'articolo 114 della nostra Costituzione con la definizione: «Roma è la capitale della Repubblica». altri interventi legislativi nel 2009 e nel 2010 in attuazione del federalismo fiscale, il decreto legislativo del 2011 per funzioni e valorizzazioni e il già citato ridimensionamento del decreto legislativo

Questo è il senso propositivo e l'intento della mozione che Fratelli d'Italia ha sottoscritto alla Camera e al Senato e che quindi - anticipo - convintamente voterà. però, sottolineare talune cose. Non è stata solo la pandemia a contribuire a questa distrazione istituzionale verso Roma e la ricorrenza in oggetto. Infatti, non si era predisposto il calendario degli eventi a partire dalla data del 20 Settembre 2020, cioè l'anniversario della Breccia di Porta Pia, fino al citato 3 febbraio, mentre il 50° anniversario dell'unione di Roma all'Italia nel secolo scorso fu ampiamente celebrato con iniziative istituzionali. Lo stesso dicasi per la ricorrenza dei cento anni dalla proclamazione di Roma Capitale, celebrata come completamento dell'unità d'Italia e come chiusura dell'epopea risorgimentale. centocinquant'anni sono stati trascurati. Mi piace ricordare un bel francobollo celebrativo di Poste italiane e qualche iniziativa quel giorno; però poca roba. Ma qual è il *vulnus*, al di là di là del 3 febbraio scorso? Il *vulnus* è più profondo, cari colleghi, ed è l'attribuzione a Roma Capitale di poteri speciali, cui devono o dovrebbero corrispondere fondi speciali. Questa è peraltro la storica posizione di Fratelli d'Italia, che siamo contenti abbia visto anche la convergenza di altre forze politiche, come dimostra l'approvazione dell'ordine del giorno alla Camera a firma Meloni e Rampelli nel febbraio scorso, ma anche l'assemblea capitolina del 24 febbraio scorso dedicata a maggiori fondi e poteri per Roma Capitale, con un consenso trasversale. Mi riferisco alla richiesta di poteri speciali per la città di Roma, per le altre capitali europee: Parigi, Berlino, ma anche Londra pre e post Brexit. Qual è il punto, cari colleghi? La piena attuazione della riforma in materia di poteri, risorse e funzioni di Roma Capitale. È evidente a tutti che non sono bastati gli importanti dispositivi introdotti nella Costituzione, né la legge ordinaria sui poteri e le competenze speciali, perché sono rimasti senza conseguenze concrete e perché la legge ordinaria è rimasta senza i decreti attuativi. C'è un passaggio interessante di previsione nella legge di bilancio 2021, che ci auguriamo venga attuato, mentre - e questo non lo notiamo solo noi, ma direi che è stato notato in termini *multipartisan* - c'è un insufficiente stanziamento nel *recovery plan*. Spiace dover ricordare - lo dico in questo caso senza polemica - che il 31 marzo scorso è stata bocciata la proposta di Fratelli d'Italia di destinare alla capitale nel PNRR un miliardo all'anno

è anche la sede di organismi internazionali che rafforzano la vocazione internazionale di Roma. A Roma si concentra un immenso patrimonio artistico e monumentale; il centro storico di Roma è è un sito dell'UNESCO. Rilanciare Roma Capitale, colleghi, significa rilanciare l'Italia intera, significa investire sul futuro della Nazione, perché il futuro della Nazione passa per le strade di Roma. Senza Roma non ci sarebbe stata l'Italia unita e libera che noi abbiamo conosciuto e che ci piace ricordare. È per questo che che dobbiamo recuperare tutti (non è una questione di parte) l'orgoglio della romanità e anche della capitale di una Nazione. Per Fratelli d'Italia i poteri speciali di Roma Capitale non sono un problema della città di Roma, ma una questione di rango e di livello nazionale. Rilanciare Roma significa appunto puntare sul futuro dell'Italia, perché, cari colleghi, Roma è storia, è civiltà, deve essere orgoglio. Roma Capitale, però, non deve soltanto essere evocata, deve ricevere strumenti e risorse che la mettano in condizione di affrontare le sfide che ci attendono e anche di primeggiare, come può o come potrebbe, tra le capitali europee. Voglio anche aggiungere che Roma nell'immaginario collettivo mondiale è il centro della storia. Goethe ha scritto: «Roma è la capitale del mondo» e di Roma capitale del mondo, di Roma capitale d'Italia, di Roma centro della storia non dobbiamo dimenticarcene noi

consentitemi, un finanziamento particolare, per il finanziamento con il quale viene oggi trattata, la capitale d'Italia sostanzialmente

dei ruoli, delle rappresentanze, un peso non solo perché è capitale del Paese, ma perché è un *unicum* in quanto capitale mondiale della cristianità. La sua funzione capoluogo del Lazio, capitale d'Italia, capitale mondiale della cristianità.

tutte le cose che si dicono e si fanno in un periodo elettorale, come è quello a pochi mesi dal rinnovo del Consiglio comunale del Campidoglio, forse può essere strumentalizzato,

da tanti anni del suo *status* istituzionale, alla Camera sono in discussione in Commissione affari istituzionali alcuni provvedimenti. La discussione è delicata,

dalle risorse normali legate alle funzioni straordinarie che per sua natura la capitale d'Italia, capoluogo della Regione e capitale mondiale del cattolicesimo e della cristianità deve affrontare. Dichiaro quindi, anche a nome Dichiaro quindi, anche a nome del Partito Democratico, il voto favorevole a questa mozione, perché è giusto porre in quest'Aula, al centro della nostra discussione, un tema così importante e vitale per il nostro Paese. *(Applausi)*. Grazie,

è diventata capitale del nostro Paese e certamente questo è stato un fatto straordinariamente importante, che ha segnato davvero la nascita dello Stato italiano.

torno a ripetere - riguarda soltanto i cittadini romani, i cittadini dell'area metropolitana, del Lazio o i parlamentari di Roma, ma è una questione nazionale. Così com'è stata una questione nazionale Berlino, capitale Grazie,

come per tutte le altre capitali. Poi sceglieremo le forme; il dibattito è aperto da molti anni, ma credo sia necessario assumere, tutti insieme, una decisione su questo. Contemporaneamente vi è un disegno di legge ordinario, perché

di un governo vero del territorio. Questo non riguarda chi in quel momento governa la città, perché in quest'Aula praticamente abbiamo governato un po' tutti Roma e in un modo o nell'altro vi sono state alternanze, ma le questioni davanti a noi sono rimaste praticamente le stesse. le stesse. Credo sia arrivato il momento di fare questo salto di qualità e finalmente spero che alla Camera

Siamo, alla vigilia del rinnovo del consiglio comunale e delle elezioni, ma, torno a ripetere, non si tratta di una questione di parte. È una questione che riguarda

istituzionale e poteri speciali che permettano di governare al meglio, è importante per tutto il nostro Paese. Quindi, con l'auspicio che questa mozione possa portarci rapidamente a definire sia il ruolo che i finanziamenti

fa, a Roma, è nato un coordinamento, un osservatorio dei parlamentari eletti a Roma e, quindi, insieme abbiamo redatto una mozione per richiamare, per la verità già da mesi, le istituzioni, i Governi, il Governo dell'epoca, a celebrazioni adeguate per i centocinquant'anni di Roma Capitale. Non è solo per retorica. Potrei fare una citazione: «L'Italia è restituita a se stessa e a Roma. Qui, dove noi riconosciamo la patria dei nostri pensieri, ogni cosa ci parla di grandezza». È scritto dietro la presidente Rossomando. Nessuno di noi le guarda, ma ci sono queste lapidi.

Non voglio fare qui una lezione di storia: non sarei all'altezza né i colleghi ne hanno bisogno. Tuttavia, credo che avere consapevolezza del ruolo della nazione e del ruolo della capitale un fatto importante. Roma, poi, è stato un luogo controverso, di polemiche, addirittura definita mafiosa. Poi, però, non lo era: c'era la corruzione, come c'è stata in tante parti d'Italia e del mondo. La Corte di cassazione ha però tolto quel marchio, che era stato con superficialità appioppato alla Capitale, con un danno di immagine gigantesco al Paese di cui qualcuno poi dovrebbe essere chiamato a rispondere. Per questo, però, basta leggere i libri di Sallusti e Palamara, non c'è bisogno che io ne parli qui.

Credo, pertanto, che si debba riflettere sul ruolo della nazione, sul ruolo della capitale e, certo, anche sui poteri. Nel dibattito è emerso qualcosa. Dico alla collega Rauti, che conosco e stimo da tempo e che è alla sua prima legislatura, che, che, negli anni Ottanta, il Governo Craxi fece una legge speciale per Roma; nel 2008 e nel 2009 il Governo Berlusconi ha fatto norme e leggi per Roma. È stata cambiata la Costituzione, introducendo la dicitura Roma Capitale. Non basta, però, cambiare il nome.

che vuole introdurre in Costituzione dei poteri maggiori per Roma, affinché venga equiparata ad una Regione. Come in altri Stati del mondo, dell'Occidente, la città capitale ha dei poteri che non sono quelli degli altri Comuni: per gli oneri,

le lapidi e la storia ce lo ricordano. Poi, noi ce ne dimentichiamo nel percorso che ha portato a questo traguardo. Io credo, quindi, che questa mozione impegni il Governo a fare qualcosa in più, da qui alla fine dell'anno, per celebrare i

su temi di varia natura. Credo si possa tranquillamente, a costo zero, avere un momento più solenne di celebrazione con il Presidente della Repubblica e le massime istituzioni. Si promuovono

non dico l'anzianità, ma l'esperienza politica maturata sia sul territorio che in queste Aule. Noi avvertiamo il dovere di porre una questione storica, culturale, identitaria, costituzionale e normativa. Roma può stare anche antipatica perché è sempre al centro delle polemiche. Peraltro, Roma ospita i difetti suoi e dell'Italia, perché a Roma tante vicende negative

un servizio e un'esigenza della comunità nazionale intera e non una rivendicazione di natura campanilistica. Mi auguro che la mozione in esame venga approvata - il nostro Gruppo la sostiene

la spinta per leggi utili alla capitale e quindi alla Nazione.

con l'intento di voler diffondere e valorizzare il suo ruolo di capitale, promuovendo lo sviluppo futuro della città, tramite una serie di iniziative celebrative e commemorative, in occasione della ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione a capitale d'Italia. Riteniamo che il ricorrere il ricorrere del 150° anniversario dalla proclamazione di Roma Capitale debba però rappresentare l'occasione per affrontare più compiutamente un tema di importanza strategica, non solo per la città di Roma, ma per l'intero Paese, con l'auspicio che questa discussione possa rappresentare un primo ma importante tassello nel percorso che veda il Parlamento riconoscere a Roma una maggiore autonomia nell'esercizio di poteri e di funzioni, dotando la capitale d'Italia delle necessarie risorse, utili a una migliore gestione del suo patrimonio archeologico, storico e architettonico. Proprio oggi che Roma si appresta ad affrontare il 150° anniversario dalla sua proclamazione a capitale del Paese, ritengo che non sia più rinviabile il riconoscimento di uno *status* che in termini di autonomia possa realmente garantire l'obiettivo di poter preservare il valore di città eterna, di città aperta, simbolo di vittoria e liberazione, che le è riconosciuto a livello internazionale. Se guardiamo Roma con uno sguardo alle altre capitali europee, come correttamente sottolineato dalla mozione che stiamo discutendo, non si può non constatare come le maggiori capitali europee e occidentali godano di finanziamenti specifici per l'espletamento delle funzioni connesse al loro ruolo in seno all'ordinamento statale, indispensabile anche per contribuire alla conservazione e alla valorizzazione di un patrimonio storico e culturale di enorme valore che raramente appartiene alle sole amministrazioni locali, che necessita dunque di interventi dei rispettivi Stati nazionali. Non possiamo parlare di Roma senza considerare che il suo suo territorio da solo risulta più grande di quello delle altre otto più grandi città italiane messe insieme ed è equivalente alla somma di nove tra le maggiori capitali europee: parliamo di Amsterdam, Berna, Atene, Bruxelles, Copenaghen, Dublino, Lisbona, Parigi e Vienna. Nonostante questi dati pongano in evidenza la grandezza di Roma, non si può fare a meno di evidenziare come a ciò non corrisponda un adeguato riconoscimento normativo in termini di autonomia che spetta invece alle principali capitali europee che, sia pure con specifiche diverse, godono di forme di autonomia riconosciute dai rispettivi ordinamenti. A titolo esemplificativo, in Germania e Austria, Berlino e Vienna sono *Länder;* in Spagna, Madrid rappresenta una comunità autonoma; in Belgio, Bruxelles è divenuta la terza regione. Guardando oltreoceano, Washington non è solo la capitale degli USA, ma è anche uno Stato. è l'unica città al mondo che ospita tre circuiti di ambasciate: come capitale della Repubblica, come sede dello Stato della Città di Vaticano e come sede Al contempo, però, Roma è una delle poche capitali mondiali che ancora oggi non gode di una particolare autonomia. Condividiamo la preoccupazione espressa nella mozione in esame per la drammatica emergenza economica causata per la città di Roma dall'epidemia da Covid-19, in particolare con la paralisi del settore del turismo, da sempre asse portante dell'economia cittadina, per cui si rende necessario un sostegno straordinario da parte dello Stato nei confronti della città. Riteniamo che oltre a questo sostegno straordinario, in occasione della ricorrenza dei centocinquant'anni dalla sua proclamazione a capitale, Roma meriti anche una nuova considerazione all'interno dell'ordinamento italiano. Ricordo infatti che oltre ad essere la nostra capitale, come riconosciuto dall'articolo 114 della Costituzione, Roma è stata definita dalla legge n. 42 del 2009 come ente territoriale Roma Capitale. In virtù di ciò, le sono state riconosciute specifiche funzioni amministrative sul tema dell'edilizia pubblica e privata, dello sviluppo economico, dei beni culturali e della protezione civile. Il primo *vulnus* normativo che riteniamo debba essere quanto prima superato sta nel fatto che le prerogative riconosciute a Roma Capitale insistono solo sul territorio comunale e non sull'area della Città metropolitana, così come istituita nella legge n. 56 del 2014. Una soluzione a questa incongruenza consisterebbe nel voler costringere l'area metropolitana con quella comunale, costituendo una Roma centrale cui la Regione Lazio dovrebbe inevitabilmente cedere alcune competenze. Attraverso un decentramento municipale, si tratterebbe di riconoscere anche ai singoli municipi, oggi nell'area metropolitana, maggiori poteri e maggiore autonomia, anche finanziaria, sui propri territori nell'interesse dei cittadini e dei servizi che ad essi vanno erogati. Solo così potremo veramente riconoscere a Roma il ruolo di capitale del Paese, valorizzando al contempo i singoli municipi che ad oggi ricadono nell'area metropolitana e che spesso faticano a godere delle risorse di cui necessiterebbero perché il più delle volte trattenuti a livello centrale. Sono questi gli obiettivi che si prefigge di poter raggiungere la nostra proposta di legge disposizioni sull'ordinamento della Città metropolitana di Roma Capitale che, riconoscendo ad essa una propria autonomia, creerebbe indubbi benefici anche agli altri capoluoghi della provincia del Lazio. Parliamo di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina che il più delle volte vedono sottratte dai propri territori risorse regionali che con l'ordinamento attuale vengono perlopiù fagocitate da Roma, alla quale dovrebbero invece essere destinate risorse specifiche dello Stato. Per tale ragioni un voto favorevole alla mozione in esame con l'auspicio che essa possa rappresentare il primo tassello di un percorso legislativo che veda finalmente il Parlamento discutere di Roma e di quanto necessario affinché quella che da centocinquanta anni è la capitale del nostro Paese, sede delle principali accademie di arte e cultura, centro della cristianità del mondo e culla culla del diritto, possa vedere pienamente riconosciuto il suo *status* di capitale italiana.

per aver presentato la mozione sulla celebrazione del 150° anniversario dell'unione di Roma allo Stato italiano e quindi della sua proclamazione a capitale d'Italia.

come spesso accade c'è una parte dell'emiciclo che è molto rumorosa e non consente di ascoltare l'intervento della collega.

abbastanza scontato. Roma è già una celebrazione vivente. Bisogna ricordare Roma non solo per il Giubileo o per le polemiche sterili, che si sentono spesso. Bisogna lavorare insieme, concretamente. *(Commenti).*

Desidero ricordare le parole del presidente Mattarella, che è stato presente, insieme a tutte le istituzioni e anche al vicario di Roma, il portavoce del Papa, alla prima celebrazione che ci fu nel febbraio 2020. Egli disse proprio che «Roma può dare tanto allo sviluppo del Paese» e che «la comunità nazionale deve assicurare il sostegno necessario, affinché le funzioni della capitale siano svolte al meglio

quindi mi auguro che, dopo le parole, seguano i fatti. Ovviamente Roma ha bisogno di risorse *ad hoc* e sono indispensabili anche per contribuire alla conservazione e alla valorizzazione di un patrimonio storico e culturale di enorme valore. patrimonio nazionale, prima ancora che della singola amministrazione comunale. Vengo al punto:

Fermi restando gli argomenti già previsti dal calendario corrente, la prossima settimana l'Assemblea si riunirà a partire da martedì 20 aprile, dalle ore 16,30 alle 20, per la terza lettura del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, ove concluso della Commissione, nonché per le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri. Nella giornata di mercoledì 21 si procederà alla discussione del decreto-legge sul riordino dei Ministeri, ove concluso della Commissione; diversamente si proseguirà con la discussione delle ratifiche di accordi internazionali. Giovedì 22 aprile avrà luogo la discussione congiunta del Documento di economia e finanza 2021 e della Relazione sullo scostamento dall'obiettivo programmatico di bilancio. Per quest'ultima è previsto il voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. La replica del Governo e le dichiarazioni di voto finale avranno luogo con trasmissione diretta televisiva. Martedì 27 aprile, alle ore 15, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per la discussione sono state ripartite tre ore e trenta minuti, escluse le dichiarazioni di voto. Per la replica del Presidente del Consiglio dei ministri e le dichiarazione di voto è prevista la trasmissione diretta televisiva. Il calendario della settimana dal 27 al 29 aprile prevede inoltre, oltre all'eventuale seguito del decreto-legge sul riordino dei Ministeri, la discussione del decreto-legge in materia di trasporti e traffico crocieristico nella laguna di Venezia. Giovedì 29, alle ore 15, avrà luogo il *question time.*

e che lo faccia con sempre maggiore attenzione e incisività: in sede ONU, nelle sedi dell'Unione europea e in tutte le sedi internazionali opportune, fino a che non sarà raggiunto l'obiettivo della rimozione definitiva dell'embargo contro la Repubblica di Cuba che dura da quasi sessant'anni. Coerentemente, questo, con tutti gli appelli umanitari che si sono sollevati in questi ultimi tempi di atroce pandemia globale, che sono partiti dal Pontefice, dal Segretario generale delle Nazioni Unite a marzo 2020, dal *leader* dei Paesi del G20, affinché ci sia un allentamento delle sanzioni economiche, esortando a sospendere le sanzioni che minano la capacità dei Paesi di rispondere alla pandemia e a continuare ad adoperarsi, soprattutto in coordinamento con i Paesi dell'Unione europea e nei fori multilaterali, affinché il meccanismo sanzionatorio, tutt'ora applicato nei confronti di Cuba, non contempli ostacoli alla fornitura di generi di prima necessità, inclusi medicinali e strumentazioni mediche. Ciò coerentemente, inoltre, con il voto, quasi unanime, di condanna del blocco, che per 28 volte consecutive ha visto l'Assemblea generale dell'ONU esprimersi in tal senso. Il drammatico periodo causato dalla rapida diffusione del Covid-19 e la conseguente situazione di emergenza in cui è precipitato il mondo hanno messo in difficoltà tutti; ma, più di tutti, quei Paesi che subiscono embarghi, come Cuba, che lo subisce, appunto, da sessant'anni, ma non solo Cuba. I blocchi economici, commerciali e finanziari, mossi da interessi economici, commerciali e finanziari, ma soprattutto politici (diciamocelo), ricadono inevitabilmente sempre sui più deboli, sulle popolazioni. La pandemia è stata una lente di ingrandimento su una situazione, quella di Cuba, oramai insostenibile, mettendo in evidenza i danni socio-economici del blocco, aggravati dagli inasprimenti messi in atto dall'Amministrazione Trump proprio nel periodo peggiore, proprio nel periodo di maggior bisogno sanitario e sociale, bloccando anche l'approvvigionamento di medicinali e del materiale sanitario. Non dovrebbe essere necessario ricordare all'Italia che, mentre questo accadeva nell'indifferenza di tanti, Cuba era tra i Paesi che hanno prestato soccorso al nostro Paese nel marzo 2020, inviando, su richiesta delle Regioni Lombardia e Piemonte, che in quel periodo erano davvero sotto una pressione indicibile, due brigate mediche composte da immunologi e infermieri specializzati in interventi di contrasto alle pandemie; medici e logisti che hanno operato a Crema e Torino, due dei focolai più rilevanti del Nord Italia. La nostra valutazione, infatti, deve prescindere da questo, anche se non lo si può ignorare. Quindi il nostro impegno su questo deve essere inteso solo a vantaggio della popolazione, qualunque sia la nostra valutazione di tipo politico.

il nostro Gruppo ha voluto dare un contributo, spero fattivo, non ideologico e molto più pratico, alla discussione

può dimenticare che Cuba è stata protagonista per molti decenni di gravi e prolungate limitazioni dei diritti delle persone, delle libertà economiche e anche di diritti fondamentali e che questo purtroppo prosegue anche dopo la riforma costituzionale del 2019. A Cuba infatti vige un regime fondato su un partito unico. Deve però essere ricordato, per fare chiarezza, un aspetto che forse pochi conoscono, ossia che né l'Italia, né l'Unione europea in questo momento hanno in vigore sanzioni contro Cuba. Le sanzioni contro Cuba sono degli Stati Uniti. È chiaro che gli Stati Uniti applicano sanzioni unilaterali con portata extraterritoriale e che questo ha un riflesso anche sulle attività economiche degli imprenditori italiani. Quindi, è giusto ricordare che l'Italia e l'Unione europea in questo momento non hanno in vigore sanzioni e provvedimenti restrittivi del commercio nei confronti dell'isola di Cuba. L'ordine giorno ricorda anche che il 23 marzo il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato con il voto contrario dell'Italia un provvedimento che andava a criticare l'impatto negativo di alcune misure coercitive. Più in generale, noi vogliamo sottolineare la necessità di passare da sanzioni indiscriminate che rischiano di avere scarsa efficacia e che vanno a colpire la vita delle persone normali a sanzione più mirate. Da questo punto di vista, ricordiamo la risoluzione approvata dalle Nazioni Unite con il voto contrario dell'Italia, che ha suscitato parecchie polemiche. Brevemente in questa risoluzione dell'ONU si faceva riferimento alla condanna dello strumento delle sanzioni unilaterali. Il documento, infatti, «esorta vivamente tutti gli Stati ad astenersi dall'imporre misure coercitive unilaterali»

Andando al dispositivo, ricordiamo sicuramente che l'Italia è uno dei principali *partner* commerciali dell'isola di Cuba e non si può neanche dimenticare - è un nostro dovere di riconoscenza - la presenza di molti medici cubani che l'anno scorso in soccorso dell'Italia durante i tristissimi e drammatici mesi dell'inizio della pandemia. Spero che la nostra proposta possa ottenere ascolto, considerazione e attenzione da parte del Governo, che mi pare impegnato a fare altro in questo momento.

l'attenzione del Governo rispetto alla parte dispositiva del nostro ordine del giorno che impegna l'Italia a cambiare il registro delle sanzioni, passando da sanzioni unilaterali generalizzate a sanzioni più oculate

dei Governi e non la generalità della popolazione. Su questo argomento, che ho dovuto sintetizzare per necessità di tempo, il Gruppo Fratelli d'Italia - lo dirà più tardi il collega Urso - sollecita un confronto vero con il Governo affinché l'Italia possa adoperarsi per tutelare gli interessi nazionali ed economici delle nostre imprese rispetto alle sanzioni unilaterali extraterritoriali degli Stati Uniti. Speriamo che il Governo voglia accogliere il nostro ordine del giorno che - ripeto - non è ideologico, ma pratico e concreto. È rivolto alla tutela degli interessi nazionali, senza colpire la popolazione, ma i responsabili politici delle restrizioni della libertà nei Paesi come Cuba.

che il testo è stato presentato il 26 maggio del 2020, in una fase di estrema emergenza e in risposta a un segnale arrivato dal popolo cubano. Detto questo, a fronte della votazione

Vorrei entrare un po' nel merito di queste sanzioni. Di cosa stiamo parlando? Se facciamo un passo indietro nel secolo scorso, tutto avvenne intorno ai primi giorni di gennaio del 1959, quando i cosiddetti *barbudos* entrarono finalmente all'Avana (8 gennaio 1959). Un anno e mezzo dopo avvenne la nazionalizzazione di tutte le industrie che risiedevano che risiedevano sul suolo cubano; a seguito di quella nazionalizzazione partì l'embargo da parte degli Stati Uniti. Quindi stiamo parlando sostanzialmente di un rapporto tra gli Stati Uniti e l'isola di Cuba, che non ci riguarda. Perché dico che non ci riguarda? Non ci riguarda perché, se andiamo sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, notiamo che alla voce sugli embarghi finanziari da parte dell'Italia l'isola di Cuba non c'è. Quindi l'Italia non deve vergognarsi, come ha detto qualcuno, ma deve essere fiera del fatto che, in risposta a quell'atto fatto dai dai medici cubani, noi non abbiamo applicato delle sanzioni dirette. Ma c'è di più: se andiamo sul sito della Commissione europea a vedere quali sono le restrizioni finanziarie che l'Unione europea ha applicato ai vari popoli del mondo che sono in una *black list*,

Facciamo il punto sulle sanzioni. Queste ultime sono uno strumento di politica estera, sono un atto diplomatico sancito dal diritto internazionale; non stiamo parlando di atti criminali o di cose di questo tipo. Se volessimo seguire il solco tracciato da questa mozione,

L'embargo non ha intaccato minimamente questo aspetto, tant'è che addirittura solo nel 2016 nell'isola di Cuba è stato permesso l'uso dei telefoni cellulari. Non è che sono arrivati i cellulari: era proprio vietato usarli. Quindi l'embargo ha effetti paradossali su questi aspetti, che molto spesso dipendono dalle scelte proprie dell'isola. Ma veniamo ancora al punto. Come possiamo aiutarli? Ad esempio chiedendo che aderiscano al *Cuban democracy act*, nel quale si chiedono elezioni libere. Giusto per lasciarla agli atti, ho stampato la scheda elettorale delle scorse elezioni, che sono avvenute proprio in concomitanza con le nostre: una scheda elettorale del 2018, in cui c'è un solo partito (ancora nel 2018). Questo forse dovremmo fare: aiutarli a

sono fermi addirittura al 1903; mi riferisco ai rapporti bilaterali di amicizia, di scambio economico, di crescita economica, culturale e democratica. Questo possiamo fare; per il resto, credo si tratti di rapporti che non riguardano

di un Paese, ma il fatto che medicinali e generi di prima necessità non arrivino alle popolazioni, perché c'è un embargo politico. Il 29 marzo centinaia di cubani hanno manifestato a L'Avana con una sfilza di auto e moto d'epoca per chiedere agli Stati Uniti, certo, e non all'Italia, che non ha niente di cui vergognarsi perché si è sempre prodigata in questo verso, di revocare l'embargo contro l'isola in vigore da oltre sessant'anni. La protesta ha avuto luogo anche in altre 50 città in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti. Le manifestazioni erano per chiedere all'Amministrazione Biden di eliminare l'embargo. «Chiediamo la fine del blocco», ha dichiarato il ministro Rodriguez. «L'inasprimento opportunistico del blocco durante il governo Trump, nel bel mezzo della pandemia Covid-19, lo rende ancora più genocida», ha aggiunto. Il 23 marzo il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione sull'impatto negativo delle misure coercitive unilaterali e sul godimento dei diritti umani e ha sottolineato che tali misure impediscono la piena realizzazione dello sviluppo economico e sociale delle Nazioni, influendo anche sulla piena realizzazione dei diritti umani. La risoluzione approfondisce le conseguenze drammatiche che misure come l'embargo creano sulla popolazione e sottolinea, inoltre, che queste colpiscono sempre le frange più deboli della società. Ci sembra importante anche ricordare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e Cuba, firmato nel dicembre 2016, che ha inteso imprimere un nuovo corso alle relazioni euro-cubane, per una migliore cooperazione bilaterale, in controtendenza all'extraterritorialità del blocco, che colpisce, tra l'altro, la possibilità di rapporti economici tra Cuba e l'Europa. L'Accordo riapre il rapporto di *partnership* tra l'Europa e Cuba e deroga alla posizione comune del 1996,

Non si può dimenticare, però, che l'Amministrazione Trump ha inasprito l'embargo contro Cuba e ha portato indietro l'orologio del tempo, oltre ad aver abrogato una serie di norme che consentivano agli statunitensi di viaggiare a Cuba per turismo e aver limitato le rimesse degli emigranti, colpendo così le due principali fonti di reddito dell'isola. Le mosse di Trump hanno segnato il totale capovolgimento degli sforzi dell'Amministrazione Obama per ricostruire i legami con l'isola. L'attuale presidente degli USA Biden ha promesso in campagna elettorale che avrebbe cambiato la politica verso l'isola, affermando che le politiche di Trump avevano inflitto danni al popolo cubano e non avevano fatto nulla per promuovere la democrazia e i diritti umani. Al momento afferma che la revisione dell'approccio verso L'Avana è in corso, ma la Casa Bianca non ha indicato ancora quando agirà e cosa farà e se intende davvero proseguire con la storica distensione tra Cuba e gli Stati Uniti che era stata avviata da Obama. quindi che il Governo accetti questo nostro invito in linea con gli appelli che sono venuti, soprattutto in quest'anno, anche dal Pontefice.

la proposta del Governo è di modificare nel seguente modo: «*premesso che*: a Cuba persistono gravi limitazioni dei diritti civili e politici e diffuse violazioni delle libertà fondamentali confermate dall'esistenza tuttora

anche dando applicazione alle Convenzioni internazionali dell'ONU sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1996, firmate da L'Avana nel 2008 ma finora non ratificate dal Parlamento cubano

questione interessante ed importante, ma perché nell'economia di una riflessione che parte da un Paese singolo forse meriterebbe un altro tipo di discussione in un'altra sede.

Signor Presidente, la discussione di oggi mi offre l'opportunità di evidenziare brevemente le linee di fondo della politica italiana ed europea verso Cuba, nonché la posizione tradizionalmente espressa dall'Italia in ambito ONU nei confronti dell'embargo che gli Stati Uniti hanno imposto all'isola all'inizio degli anni Sessanta. I rapporti italo-cubani, pur nel contesto di una concezione della democrazia e dei diritti umani evidentemente non coincidenti, sono improntati dei diritti umani evidentemente non coincidenti, sono improntati a una tradizionale amicizia e vengono periodicamente passati in rassegna nel quadro di un meccanismo di dialogo politico che si riunisce a cadenza regolare alternativamente a Roma e L'Avana, nel corso del quale non manchiamo di rappresentare alla controparte le nostre aspettative in termini di aperture sul versante delle libertà fondamentali. Cuba è anche un Paese prioritario della nostra cooperazione allo sviluppo, uno *status* che consente la programmazione e l'attuazione di importanti progetti che interessano settori cruciali della società cubana e la rilevanza dei quali oggi è ulteriormente accresciuta visto il duro impatto che la pandemia da Covid-19 ha prodotto sull'isola. Nel dicembre 2016, l'Unione europea ha firmato con L'Avana un accordo di dialogo politico e di cooperazione che ha ridefinito il quadro complessivo delle relazioni euro-cubane. In linea con questo rinnovato slancio l'Italia sta contribuendo ad accompagnare il complesso percorso di attualizzazione del sistema economico dell'isola, una sfida che il Governo cubano ha intrapreso da alcuni anni e che ha quindi trovato un inquadramento istituzionale all'interno della Costituzione del 2019. Uno dei dialoghi settoriali che discendono dal citato Accordo di dialogo politico e di cooperazione è interamente dedicato alle tematiche relative alle misure coercitive unilaterali. L'ultima sessione, tenutasi lo scorso 25 marzo, ha permesso pertanto di discutere in dettaglio le conseguenze dell'embargo statunitense e della recente applicazione dei titoli III e IV della legge Helms-Burton, i cui effetti extraterritoriali pongono una seria minaccia agli interessi di operatori economici europei e sulla quale l'attenzione di Bruxelles rimane particolarmente elevata. Un altro dialogo settoriale che nel contesto dell'Unione europea conduciamo con Cuba su base regolare, certamente non meno importante, è invece quello sui diritti umani, la cui ultima sessione si è tenuta lo scorso 26 febbraio, nella quale sono state affrontate anche le note e perduranti criticità dell'isola in questo settore. Il solido ma anche franco rapporto con Cuba fa sì che l'Italia sia bene a conoscenza delle complesse relazioni che intercorrono tra L'Avana e Washington, sulle quali grava in maniera preponderante l'embargo che gli Stati Uniti mantengono nei confronti dell'isola. Durante il mandato dell'Amministrazione Trump, l'embargo ha subito un progressivo inasprimento del meccanismo sanzionatorio ed è stato applicato senza più alcuna eccezione, com'è dimostrato dall'inserimento di Cuba lo scorso gennaio tra i Paesi *sponsor* del terrorismo, provocando tra l'altro una sensibile contrazione dei partenariati economico-commerciali di Cuba su scala internazionale. La nuova Amministrazione statunitense ha adottato un atteggiamento di cautela verso l'isola e ha mostrato sinora scarsa propensione ad intraprendere azioni in discontinuità con il passato. Nello scorso mese di febbraio è stata decisa la proroga di un anno del provvedimento di *national emergency* funzionale all'attuazione dell'embargo, in attesa di completare l'esame della fitta rete di restrizioni vigenti. Qualsiasi eventuale cambio di rotta, inclusa l'ipotesi della ripresa del dialogo con L'Avana, che comunque non sembra rientrare tra le priorità della nuova amministrazione, sarà fondato sul pilastro dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L'Italia si è sempre espressa, di concerto con gli altri Stati membri dell'Unione europea, promuovendo con essi una linea contraria al blocco economico e ai suoi effetti extraterritoriali verso Paesi terzi ritenuti contrari al diritto internazionale e votando tradizionalmente a favore della risoluzione che il Governo cubano presenta annualmente all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Si tratta di una linea coerente e consolidata, come confermato dall'ultimo voto del novembre 2019, di cui il Governo cubano ci è grato e che confidiamo possa contribuire a migliorare il clima complessivo dei rapporti tra L'Avana e Washington, con positive ricadute per entrambi. La nostra contrarietà all'embargo, peraltro, è dovuta non solo alle ripercussioni sulla popolazione o alla già citata portata verso altri Paesi, ma anche dalla constatazione del fatto che esso non abbia in effetti contribuito a promuovere processi di apertura e di dialogo sui diritti e le libertà fondamentali. Vorrei pertanto cogliere l'occasione per ribadire che l'Italia non ha mai votato a favore delle sanzioni contro Cuba, come già chiarito dal ministro Di Maio durante l'audizione tenutasi lo scorso 31 marzo sulle linee programmatiche del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'annuale progetto di risoluzione per richiedere la fine dell'embargo statunitense verrà presentato da Cuba in Assemblea generale delle Nazioni Unite per la ventinovesima occasione consecutiva il prossimo 23 giugno. In quella sede l'Italia, in stretto coordinamento con i *partner* europei, si impegnerà a considerare favorevolmente il progetto di risoluzione per confermare il tradizionale appoggio accordato all'istanza cubana.

migliorano la comprensione del nostro testo. Sono elementi aggiuntivi e anche significativi, che vanno nella stessa direzione. Per questo motivo, le accogliamo in pieno.

intervengo molto brevemente. L'illustrazione del vice ministro Sereni è stata estremamente chiara ed esaustiva, per cui c'è poco da aggiungere. C'è da sottolineare una cosa in particolare: il il testo, che ha raggiunto una larghissima convergenza parlamentare, sottolinea in modo particolare un aspetto, riprendendo quelle che sono state le dichiarazioni del Pontefice e del segretario generale delle Nazioni Unite rimarcando una questione fondamentale. Anche in presenza di sanzioni, mai e poi mai queste possono in qualche modo riguardare la fornitura di generi di prima necessità e di strumentazioni mediche. È chiaro che la posizione del Governo italiano è quella appena illustrata. Speriamo che nella ventinovesima occasione che Cuba presenta alla prossima Assemblea delle Nazioni Unite ci sia, questa volta, la volontà e la capacità di approvarla. Così come è importante continuare nell'opera, da sempre sostenuta dal Governo italiano, di superare definitivamente l'embargo. Per questo, il nostro sarà un voto convintamente favorevole.

Impegnata da sempre nel sociale, Cuba è un Paese in cui si hanno ancora tanti problemi. Continua ad essere una realtà controversa, oggetto di molte critiche, cui bisogna guardare, però, in modo differenziato, riconoscendo lo sviluppo in atto. Anche Papa Francesco vi si è recato alcuni anni fa. La sua stretta di mano a Fidel Castro interpreta bene l'immagine del cambiamento in corso. Nonostante i tanti limiti, si iniziano a vedere i primi segnali di apertura. Il Paese - ad esempio - ha fatto passi avanti importanti in campo sanitario, nel campo della ricerca, della scuola, dell'emancipazione femminile. Ecco perché crediamo che sia il caso di dare un'opportunità a questo Paese. In piena pandemia, nei mesi scorsi Cuba si è distinta attraverso un bel gesto umanitario nei nostri confronti. Sulla bacheca dell'ospedale *covid hospital* di Torino ci sono ancora tanti messaggi lasciati da *ex* pazienti: «Mi avete donato una seconda vita»; «Avete lasciato le vostre famiglie e siete venuti qui per mesi in mezzo all'inferno della pandemia»; «Siete stati i miei angeli custodi»; messaggi che riportano, in modo semplice ma diretto, i tanti *gracias* di chi è guarito dal Covid-19 dopo settimane di sofferenza; messaggi che trasmettono la profonda gratitudine verso quei medici cubani che hanno supportato le nostre strutture ospedaliere. Non era scontato decidere di aiutarci. Cuba viveva, a sua volta, una situazione molto seria, perché i problemi strutturali, già causati dall'embargo sotto cui Cuba vive da anni, erano ulteriormente aggravati dal Covid-19. Negli stessi giorni in cui si apprestava ad aiutarci, Cuba era costretta, a sua volta, a chiudere le frontiere per settimane nel tentativo di arginare i contagi. Questo voleva dire, in pratica, mandare a rotoli la principale fonte di reddito: il turismo; turismo; un duro colpo all'economia locale, dunque, in un periodo già fortemente provato dalle politiche messe in atto dall'allora Presidenza Trump che, con il divieto imposto alle navi da crociera, aveva già provocato un calo del 15 per cento delle delle entrate del settore turistico, poi ulteriormente calato in modo drastico. In questo quadro generale di certo non facile, Cuba, sin dall'inizio della pandemia, ha scelto lo stesso di mobilitare un esercito di camici bianchi o medici, non bombe, a sostegno di diversi Paesi amici, tra cui anche l'Italia, messi in ginocchio dal coronavirus. Attraverso l'invio di personale sanitario, Cuba ha dimostrato la sua grande generosità. Nell'isola da decenni scarseggiano generi di prima necessità, medicinali compresi (nelle farmacie de L'Avana, per esempio, non ci sono antibiotici) e ciò è il frutto dell'embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti a Cuba da oltre quando si trattava di contrastare i conflitti scaturiti dalla rivoluzione castrista. Ciò vuol dire che, ancora oggi, Cuba sta subendo le conseguenze di un embargo determinato da condizioni storiche, politiche e sociali totalmente diverse da quelle odierne, tant'è che il presidente Obama, nel corso del suo mandato, aveva provato a rimuovere l'embargo senza però riuscirvi, a causa dell'opposizione messa in atto dai repubblicani che detenevano la maggioranza al Senato. al Senato. Il presidente Trump, invece, ha ulteriormente inasprito il blocco con l'aggiunta di nuove sanzioni e ha stoppato di fatto l'arrivo di una serie di prodotti, tra cui petrolio, generi di prima necessità e materiali sanitari. L'attuale presidente Biden, invece, durante la campagna elettorale ha annunciato la sua intenzione di modificare le politiche degli Stati Uniti nei confronti di Cuba, lasciando intravedere un possibile allentamento delle sanzioni. Ci auguriamo che questi intenti espressi durante la campagna elettorale possano trovare realizzazione. Anche noi di Italia Viva siamo convinti che i tempi siano maturi affinché si arrivi a un superamento di questo embargo che

di Cuba. Gli appelli per la sospensione delle sanzioni all'isola sono ormai molteplici e arrivano da voci autorevoli, a partire dal segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, che ha esortato i *leader* del G20 a rivedere la loro posizione sull'embargo a Cuba. Un appello analogo è arrivato anche dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che per ben 28 volte consecutive ha espresso a larga maggioranza un voto di condanna dell'embargo. C'è poi anche un collega democratico, il senatore Ron Wyden, Presidente della Commissione finanze del Senato degli Stati Uniti, che ha depositato un disegno di legge sulla questione e si è espresso a favore del ripristino di normali relazioni commerciali tra Cuba e gli Stati Uniti. Con il nostro voto possiamo dare forza al suo progetto e - ci auguriamo - anche agli intenti del presidente Biden, rimarcando l'importanza della ripresa dei rapporti anche al fine di alleviare le difficili condizioni di vita della popolazione cubana. Le sanzioni continuano infatti a provocare gravi disagi al popolo dell'isola. Dal punto di vista economico, gli effetti dell'embargo si sentono ancora più forti di prima. Cuba sta attraversando un periodo molto nero a causa dell'assenza di turisti impossibilitati a raggiungere l'isola anche a seguito delle restrizioni anti-Covid e ciò sta mettendo ulteriormente in crisi la già fragile economia. economia. Il superamento dell'embargo è reso ancora più urgente dalla pandemia in corso e le logiche geopolitiche che hanno determinato l'applicazione delle sanzioni tanti anni fa sono oggi superate degli eventi, a maggior ragione a seguito della situazione problematica nella quale versa l'isola. Voler continuare a mantenerle è antistorico e rischia di essere controproducente. Nei mesi scorsi Cuba si è distinta per un'operazione di grande solidarietà nei nostri confronti. Oggi abbiamo modo di esprimere, a nostra volta, gratitudine attraverso un voto che può aiutare Cuba a uscire da una paralisi che è già durata sin troppo. «Gracias Cuba» hanno scritto i pazienti di Torino. Oggi lo diciamo anche noi in quest'Aula. Così come quest'isola con i suoi medici ha contribuito a preservare un pezzo del nostro futuro, allo stesso modo con il nostro voto possiamo contribuire a nostra volta a preservare un po' del futuro dell'isola. È per questo che salutiamo con favore

di diversa cultura politica, a prima firma della senatrice Nugnes, per presentare il nostro ordine del giorno che affronta la questione di Cuba, ma che va oltre per cercare di delineare quale possa essere oggi l'uso sapiente delle sanzioni per colpire regimi o anche sistemi autoritari senza arrecare danno diretto e continuativo alle popolazioni. Una cosa sono i regimi e un'altra sono le popolazioni di quei Paesi, anche perché molto spesso le popolazioni già subiscono quei regimi. Ringraziamo il Governo di averci proposto delle modifiche integrative che sono

Credo che ciò sia importante in questo momento. Stamattina un collega di Liberi e Uguali notava come fosse importante approvare un documento unitario sulla politica industriale del Paese; in quel caso eravamo noi i proponenti della mozione e siamo stati noi anche a realizzare, con le altre forze di maggioranza, l'ordine giorno finale che reca comunque la nostra prima firma. Abbiamo dato un indirizzo e siamo felici che in quell'indirizzo di politica industriale che riguarda il settore strategico della siderurgia il Parlamento per la prima volta si sia trovato insieme a indicare al Governo, e quindi al Paese, alle forze sociali, sindacali e produttive, la strada che insieme vogliamo percorrere per riaffermare il valore della siderurgia e rassicurare non solo le imprese della filiera, ma soprattutto le imprese che utilizzano l'acciaio in Italia, che sono centinaia di migliaia. Dopo la politica industriale - lo diceva proprio il collega stamattina - c'è la politica estera; sono due *asset* in cui, per il loro valore strategico, un Paese deve delineare, possibilmente maggioranza e opposizione insieme, la sua postura.

Ancora oggi la Costituzione, ratificata non quarant'anni fa ma nel 2019, prevede che Cuba

quando era delegato al commercio estero del nostro Paese durante il Governo Berlusconi, promossi una delegazione politica e imprenditoriale a Cuba, all'Avana; pur essendo in un Governo di destra, sapevo bene qual era l'interesse del mio Paese e come era opportuno rapportarsi con un regime comunista, ovviamente nell'ambito delle regole internazionali. Quella missione la ricordano bene i cubani, perché fu anche l'occasione per siglare un accordo

conoscere prima di giudicare. Pertanto Cuba è un regime in cui i dissidenti vengono ancora oggi puniti e in cui nella Costituzione vi è soltanto il Partito comunista. Cuba è però anche un popolo generoso, uno straordinario patrimonio culturale e che si riconosce nella comune religione cattolica. Il ruolo della Chiesa a Cuba è fondamentale ancora oggi perché quel regime, a differenza di altri regimi comunisti, non ha conculcato la Chiesa. È una differenza sostanziale che bisogna percepire, pur contrapponendosi. Cuba ha uno spirito generoso al punto tale che ha inviato - e noi lo riconosciamo una sua delegazione nel momento più acuto della pandemia. A Cuba il sistema comunista ha investito soltanto nella scolarizzazione e nel sistema sanitario, come sapete meglio di me voi che l'avete frequentata anche per motivi ideologici. Tralasciando tutto il resto, dobbiamo riconoscere questo aspetto. Si parla di vaccini cubani che arriveranno tra breve. Riconosciamo che l'atto di generosità, ovviamente avallato dal regime, ha colpito anche noi italiani,

e lo sa il nostro Paese. Per tale ragione abbiamo colto l'occasione per ribadire la politica italiana ed europea nei confronti di Cuba, senza intrometterci nella politica americana perché è diversa la sensibilità. Noi non diciamo cosa deve fare l'America,

Detto questo, noi abbiamo tanto rispetto verso quel popolo che nella mozione che abbiamo presentato affermiamo che comunque la politica delle sanzioni non può essere la politica dell'embargo. Chiediamo - e il Governo ha fatto bene a precisarlo sanzioni mirate, e non solo in quel caso, ma possibilmente in ogni caso; sanzioni mirate alle quali ormai anche nella legislazione internazionale ci si sta orientando sapientemente che colpiscano personalmente gli autori dei crimini

Se colpiamo le vittime degli autori dei crimini, se colpiamo le vittime dei regimi, li rafforziamo e, quando le sanzioni durano troppo a lungo, vuol dire che sono inefficaci. vera politica di sanzioni è quella che colpisce in maniera selettiva e mirata gli autori dei crimini e gli autori o le cricche di regime.

È efficace in quanto colpisce, potete dire rieduca o comunque ottiene effetti, altrimenti le sue conseguenze sulla popolazione sono controproducenti e rafforzano il regime. Vi è tale consapevolezza nella destra italiana

il Movimento dei Paesi non allineati, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, a Ginevra, ha sollevato la questione delle sanzioni come strumento generale, applicato in maniera non proporzionale rispetto

e individuali hanno un effetto deterrente, vanno a colpire gli autori dei reati o dei comportamenti contrari al diritto internazionale, mentre le sanzioni più generali rischiano a volte di colpire la popolazione, avendo un impatto sul versante del rispetto dei più elementari diritti umani. Penso sia utile che una riflessione generale sull'utilità delle sanzioni, ma soprattutto sull'efficacia di alcuni tipi di esse, venga svolta anche dal Parlamento italiano, nelle modalità più opportune e coinvolgendo gli organismi competenti. Quindi, questa può essere l'occasione per riflettere insieme sulle modalità con cui farlo. Per arrivare a Cuba, è evidente che, che, da anni, a livello europeo e italiano abbiamo relazioni bilaterali molto forti, con accordi di collaborazione in campo economico, sociale, culturale, politico e diplomatico. Da questo punto di vista, all'interno di questo quadro di collaborazione, nel

della Regione Lombardia. Eravamo in un momento di grandi difficoltà, tanto che un contingente di medici e operatori sanitari cubani arrivò nella città di Crema fu di grande aiuto, proprio in una delle aree più colpite della Lombardia, in quel momento, svolgendo un servizio

da ultimo nel novembre 2019, così come annunciato da Marina Sereni in qualità di Vice Ministro degli affari esteri. E mi sembra di capire che lo saremo anche il 23 giugno dando mandato

bilaterale, scaricano con effetti extraterritoriali su altri Paesi. Questo in riferimento al dibattito su come le sanzioni rischiano a volte non solo di colpire la popolazione a cui si rivolgono - quindi, persone che non sono responsabili per gli atti del proprio Governo - ma anche di penalizzare i legittimi interessi di aziende e imprese di altri Paesi. saluto in maniera positiva il contributo che è stato dato oggi dai colleghi perché ci permette di parlare di Cuba, del contributo importante che hanno dato al Paese in un momento di difficoltà, delle esigenze di superare l'embargo e anche di una riflessione più generale da fare in prospettiva con strumenti diversi e coinvolgendo gli organismi competenti sul sistema delle sanzioni.

più difficile per noi, quello del primo impatto. Ricordo a tutti che noi siamo stati il Paese su cui il virus ha impattato per primo, con tutte le situazioni drammatiche che ricordiamo nel Nord Italia. sono arrivati e hanno operato bene nella città di Crema e a Torino. Tra l'altro, non soltanto la sindaca di Crema ma anche oggi le istituzioni

del processo di riforme, sia economiche sia politiche, all'interno di Cuba. della Presidenza Trump ha riportato indietro quel processo che pure era stato avviato, così come accaduto per altre questioni (penso all'accordo di Parigi).

percorso verso un rapporto diverso e di collaborazione, soprattutto per arrivare alla sospensione - e io dico alla rimozione - dell'embargo. In questo momento è particolarmente urgente operare in tal senso,

ho sentito in quest'Aula riecheggiare più volte un riferimento alla nuova Amministrazione Biden. Mi permetto di inviare immediatamente un telegramma a chi lo ha fatto, non per congelare il pensiero e un sentimento - che immagino alberghi nel cuore di ciascuno di noi - finalizzato a cercare di guardare al meglio del popolo cubano. Voglio però ricordare che lo stesso Biden pochi giorni fa ha dichiarato che il problema delle sanzioni a Cuba non è una priorità del Governo americano. È fin troppo ovvio che Forza Italia considera ogni gesto di solidarietà, come quello che si è verificato nell'ultimo anno a Crema e a Torino, da parte dei medici e degli infermieri che provengono da Cuba, come un atto di amicizia e sicuramente di benevolenza nei confronti del popolo italiano. Non possiamo però sottacere, visto che abbiamo l'occasione di parlarne, la situazione drammatica che vive in questo momento Cuba. Evidenziamo immediatamente che Forza Italia è vicina al popolo cubano. Sono stato a Cuba qualche tempo fa; è un Paese del quale mi sono innamorato. Dico subito

per correttezza. È una realtà meravigliosa, con gente molto mite e incredibilmente buona, ma c'è un Governo comunista e militare ormai da sessantadue anni che ha oppresso quel popolo e dobbiamo prendere in considerazione anche questi aspetti.

nei gulag del regime castrista. È stato torturato; ha cercato più volte la fuga. È una sorta di «Papillon», ma nessuno ne ha mai parlato e sarebbe un libro consigliabile a tanti che oggi ascoltano e sanno perfettamente che quel regime ha commesso nefandezze inenarrabili. Vogliamo ricordare - dobbiamo farlo per correttezza - gli 8.000 esecutati da quando nel gennaio del 1959 Fidel Castro raggiunse il potere. Non possiamo nemmeno dimenticare

Costituzione, le libertà di parola e di stampa sono garantite conformemente ai fini della società socialista. Ciò significa che personaggi e poeti come Armando Valladares potevano e possono ancora oggi - a Cuba ci sono ancora detenuti politici - essere incarcerati per queste cose. Nelle ultime pagine di quel libro c'era l'indicazione di tutti i *gulag*, di tutti i campi di concentramento presenti a Cuba.

14 istituti penitenziari. Oggi gli istituti penitenziari a Cuba sono più di 200. Vorrà dire qualcosa? Oggi abbiamo una percentuale di incarcerati per ogni 100.000 persone superiore a 500. È il *record* dell'America Latina.

degradante efficacia, che può portare anche a reazioni. Queste sono le ragioni per le quali credo che dobbiamo fare un'attenta riflessione su ciò che sta avvenendo. Anche questi medici che sono venuti sono una cosa un po' strana, perché non abbiamo mai saputo, pur essendo state presentate alcune interrogazioni, quale sia stato il emolumento o il loro salario; pare che fosse dai 4.000 ai 6.000 euro, quindi non è che stiamo parlando, in questa situazione, di un'attività filantropica o solidaristica. Il Governo italiano ha pagato e pare addirittura che ai medici cubani, oltre naturalmente ad essere stato sequestrato il passaporto all'arrivo, perché in molti casi sono anche scappati via (non in Italia, ma in altre parti del mondo),

per un pacco di detersivo ci vuole il 20 per cento dello stipendio. Si era promesso il benessere e ci siamo ritrovati in una situazione di crisi, anche alimentare, di quel popolo. Allora giustamente diciamo che non lo possono pagare i bambini e i deboli. Quali strumenti abbiamo per farlo pagare a questo regime sanguinario, che ha dimostrato nella storia di essere tale, nonostante la cecità di tanti? Voglio ricordare il carcere di La Cabaña, che era gestito da Che Guevara, e le torture che avvenivano lì. Le vogliamo dimenticare? Oppure i campi di lavoro nei quali ancora oggi si lavora per dodici ore, incessantemente. Come ha detto con molta eleganza il Governo, diritti umani tra noi e loro non sono coincidenti; certo, non sono coincidenti, siamo su strade diametralmente opposte. opposte. C'è la necessità, in questa situazione, di guardare in faccia alla realtà, come ho detto tante volte intervenendo in Aula. Cosa possiamo fare? Vi anticipo che il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'ordine del

la speranza che si possa davvero trovare una soluzione positiva al dramma che sta vivendo Cuba in questo momento. È una situazione davvero disastrosa

il presidente dell'ordine dei medici venezuelani ci ha indicato che in Venezuela circa il 70 per cento non erano nemmeno medici.

e, di fronte a questa situazione, non possiamo dimenticare tutto ciò che è avvenuto in quella realtà, che è drammatica. E non capisco perché, nonostante ci fosse la possibilità di avere oltre 200 medici venezuelani specializzati a disposizione, questi non siano stati presi in considerazione, ma siamo andati a guardare altrove. Se togliamo le sanzioni a Cuba con questo sistema,

e soprattutto il Brasile una Nazione da non fustigare, come stiamo facendo raccontando il numero dei morti. Se ci guardiamo in casa, forse avremmo anche noi qualche cosa di cui vergognarci per ciò che è avvenuto prima dell'arrivo di questo Governo. mi permetto di ricordarle - non è una correzione, ma un'informazione - che comunque un gruppo di medici venezuelani

e per questo, di cui è stato dato atto sia dalla Regione sia dalle amministrazioni locali, sicuramente dobbiamo dire grazie a coloro che ci hanno dato una mano in un momento in cui è scoppiata una tempesta, una tragedia devastante che nessuno si poteva aspettare. Io stesso - posso citare questo episodio - nel settembre 2019, quando ho fatto parte della Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ho avuto modo di confrontarmi con il rappresentante del Governo cubano, che ha portato avanti proprio l'eccellenza medica che poi abbiamo sperimentato sulla nostra pelle.

che nella propria Costituzione richiama comunque ancora l'elemento socialista come fondamentale. Dobbiamo riportare al centro il vero oggetto della discussione, cioè il rispetto dei diritti umani,

Nel momento in cui le istituzioni internazionali e la diplomazia vanno ad affrontare questo discorso, allora sì, siamo assolutamente d'accordo con l'intraprendere un percorso che possa arrivare anche ad allentare o a eliminare determinate sanzioni. Non possiamo peraltro dimenticare un'altra cosa. Dobbiamo ricordare che l'interlocutore principale - è stato citato tantissime volte che insiste sulla manovra dell'embargo sono gli Stati Uniti, con cui abbiamo una storica e fondata relazione di amicizia e di collaborazione, al netto delle Amministrazioni che si succedono. Se è vero, infatti, che nella mozione e anche negli altri atti che abbiamo esaminato si fa riferimento a una scelta dell'ex presidente Trump di inasprire comunque la posizione degli Stati Uniti nei confronti di Cuba, è pur vero che il nuovo presidente Biden ha chiarito immediatamente che l'intenzione degli Stati Uniti è di promuovere la democrazia e i diritti umani. Questo è il vero oggetto della discussione che ci deve riguardare. Quindi, se vogliamo intraprendere un percorso per far sì che le sanzioni siano mirate e oculate e che vadano a colpire, come ha riferito il senatore Urso poco fa, i veri responsabili di comportamenti che sono di fatto antigiuridici e contrari alla morale che ci deve tenere tutti uniti

D'altro canto, nella mozione - lo ricordo perché probabilmente a qualcuno sfugge - non si fa cenno, ad esempio, ai movimenti interni cubani, che non sono decisamente allineati e ovviamente poi devono subire determinate repressioni. Credo che dobbiamo veramente fare un lavoro di diplomazia e su questo dobbiamo interloquire ancora di più con gli Stati Uniti e con tutte le altre istituzioni tutte le altre istituzioni internazionali, a cominciare dall'Unione europea, che deve farsi interlocutore e da questo punto di vista sicuramente non possiamo che

attenti a portare avanti un cammino che però non deve rischiare di rompere determinati equilibri, anche perché - lo ricordo sempre a beneficio mio, ma anche di tutti gli altri

Ricordo anche alla senatrice Nugnes che il mio Gruppo parlamentare, il mio partito politico, è quello che ha fatto dell'autodeterminazione del popolo un elemento fondante e quindi su questo dobbiamo ritornare, ossia al fatto che il popolo dev'essere il nostro primo interlocutore e il nostro primo tesoro da custodire. da custodire. Nel ribadire quindi quanto già detto in merito alla dichiarazione di voto, auspico che davvero nel prosieguo della discussione si possa riuscire ad arrivare

prima di tutto lasciatemi esprimere ancora una volta la più profonda e sincera gratitudine nei confronti di Cuba per il sostegno che ci ha offerto durante le ore più buie dell'emergenza Covid, inviando medici e infermieri. Questo gesto di vicinanza e generosità non sarà mai dimenticato dal popolo italiano. *(Applausi)*. Quella cubana è una realtà complessa e tale complessità non deriva soltanto dalle numerose sfide interne che il Paese si trova ad affrontare, ma soprattutto dalle pressioni esterne, esterne, miranti a sanzionare la politica dell'Avana, ma che nei fatti hanno avuto pesantissime ripercussioni sulla popolazione civile, il cui sviluppo è fortemente ostacolato da più di sessant'anni. Eppure, nonostante il blocco economico, la Repubblica di Cuba è riuscita a ottenere sorprendenti risultati, ad esempio nell'ambito del diritto allo studio e del livello delle cure mediche che riesce a garantire. L'avanguardia dell'industria biofarmaceutica pubblica cubana ha permesso al Paese di produrre vaccini anti-Covid di altissima qualità e senza brevetto. Questi vaccini potranno essere venduti ai Paesi più sviluppati, ma verranno anche offerti agli Stati più svantaggiati, in uno spirito di protezione e assistenza da cui dovrebbero prendere spunto alcune multinazionali dell'industria farmaceutica. Pensiamo quindi al grande potenziale che un Paese del genere ha e potrebbe sprigionare, se liberato da costrizioni anacronistiche, ingiuste e sproporzionate. Il MoVimento 5 Stelle è fermamente convinto che, rispetto alla coercizione sanzionatoria, il dialogo e la cooperazione siano strumenti migliori in termini di risultato. La medesima posizione è stata espressa dall'Unione europea nell'ambito della decisione del Consiglio UE del 2016 sull'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Cuba. Quella del blocco contro Cuba è una strategia che si è rivelata inefficace e lo prova il fatto che non ha prodotto risultati sostanziali in più di mezzo secolo, o meglio ha prodotto un risultato di cui nessuno Stato moderno dovrebbe andare fiero: ha affamato un popolo. Cari colleghi, il popolo cubano sta soffrendo tanto. Ricordo ancora quando visitai l'isola, lo sguardo degli anziani e dei bambini, generazioni a confronto unite in una sofferenza di cui non sono colpevoli, puniti per crimini che non hanno commesso, privati della dignità, ma sempre disponibili a condividere quel poco che hanno, a regalare un sorriso. Il voto dello scorso 23 marzo del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha destato molto scalpore e diverse voci male informate hanno accusato il nostro Paese di essersi opposto alla rimozione delle sanzioni su Cuba. Tengo a precisare in questa sede, come ha già fatto il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio, che quel voto aveva natura e finalità differenti. Si votava, infatti, sulla richiesta di abolire in generale lo strumento delle sanzioni quindi, non si è trattato di un voto contro Cuba. In sede ONU l'Italia ha sempre votato a favore della rimozione delle sanzioni contro Cuba (l'ultima volta, il 7 novembre del 2019, quando votammo per la fine del blocco economico insieme ad altri 186 Paesi; ad opporsi furono solo Stati Uniti, Israele e Brasile). Presidente, colleghe e colleghi, vorrei che soffermaste la vostra attenzione su questo dato: da aprile 2019 a marzo 2020 si stima che il blocco abbia causato a Cuba perdite di circa 5,5 miliardi di dollari. Complessivamente, negli ultimi sessant'anni le perdite dovute alle sanzioni supererebbero i 1.000 miliardi di dollari, una cifra astronomica per un piccolo Paese. Ancora oggi il popolo cubano non ha accesso ad alcuni generi di prima necessità. È stato riportato che le richieste a compagnie americane di medicine necessarie per i bambini e i malati oncologici rimangono inevase. I prodotti cubani non possono essere esportati negli Stati Uniti e L'Avana non può importare beni che contengano almeno una certa porzione di componenti statunitensi, anche se prodotti da aziende europee. Pensate quanto più grave sia la situazione oggi, con le difficoltà imposte dall'emergenza sanitaria connessa al Covid. è sostanzialmente impossibilitato a perseguire qualsiasi forma di sviluppo economico e la drammatica situazione è stata ulteriormente inasprita, tra l'altro in piena pandemia, dalle politiche dell'Amministrazione di Donald Trump. Auspichiamo pertanto che gli Stati Uniti del neopresidente Biden accolgano finalmente l'appello che Papa Francesco lanciò nel 2015, in occasione della sua visita a Cuba, quando chiese ai responsabili politici di proseguire sulla strada della normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi come servizio a favore della pace e del benessere dei loro popoli e di tutta l'America e come esempio di riconciliazione per il mondo intero. Concludo dicendo che siamo fiduciosi che la nuova guida statunitense potrà portare al superamento delle posizioni estremiste dei suoi predecessori, aprendo finalmente la strada a un ormai necessario e non più differibile cambio di atteggiamento nei confronti di Cuba e del suo splendido popolo. Per questi motivi, annuncio convintamente il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sui due ordini del giorno.

intervengo brevemente per parlare di dotazione organica e produzione in rapporto al Teatro dell'Opera di Roma, dal 1996 fondazione di diritto privato come gli altri enti lirici italiani, ai quali è comunque riconosciuto senso pubblicistico, nonostante la privatizzazione. Come per le altre fondazioni lirico-sinfoniche, anche nel caso dell'Opera di Roma il piano di risanamento previsto dalla legge Bray del 2013 non è stato attuato nei tempi previsti; da qui lo spostamento dei termini in avanti, che però non ha risolto il problema.

imponendo alle fondazioni lirico-sinfoniche di inviare ai Ministeri competenti la loro proposta di dotazione organica formulata secondo uno schema tipo predisposto *ad hoc.* Orbene, nel triennio 2017-2019 l'Opera di Roma ha avuto bilanci in attivo con l'organico che ora viene messo in forse. Dal 2020, poi, data la chiusura

Com'è possibile allora che la proposta di dotazione organica di Fuortes, stando a quanto reso noto dalla direzione del teatro il 16 marzo, sottostimi di oltre 100 unità la dotazione finora ritenuta adeguata, soprattutto per il settore produttivo? Com'è possibile che il numero dei contratti a tempo determinato e indeterminato proposti contrasti con la disciplina transitoria della legge n. 81 del 2019? Eppure la norma afferma che la proposta dev'essere mirata a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento ai fini statutari comuni alle fondazioni lirico-sinfoniche, che sono la tutela e la diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano, lirico-sinfonico e del balletto. Occorre ricordare al sovrintendente Fuortes, emanazione del "Sinistro" della cultura, che non è possibile fare le nozze con i fichi secchi. Se si vuole tenere l'organico produttivo al minimo, bisogna per forza puntare al precariato e dunque verosimilmente su spettacoli *prêt-à-porter,* con tanti saluti per la produzione artistica di qualità e nessuna *chance* di competere con i grandi teatri stranieri. Né lo *streaming,* che pure rappresenta un'importante opportunità soprattutto in questo momento, può sostituire gli spettacoli di tipo tradizionale.

Signor Presidente, il mio intervento è teso a portare la vicinanza della Lega e dei piemontesi perbene alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che da due giorni cercano con estrema professionalità di mantenere l'ordine in Val Susa. Nella giornata di ieri 400 antagonisti, più della metà mascherati e pronti a dare battaglia, hanno invaso il Comune di San Didero (500 anime). Sono state ore di guerriglia terribile tra le forze dell'ordine e i per nulla pacifici manifestanti, che in più occasioni hanno tentato di assaltare l'area che sarà sede della nuova autostazione internazionale per impedire agli operai di Tunnel Pietre e oggetti contundenti sono stati lanciati contro le Forze dell'ordine e massi anche di cinque chili sono stati scagliati contro il parabrezza dei furgoni che portavano gli operai. Sono stati feriti un lavoratore e tre poliziotti, tra i quali un vicequestore ancora ricoverato all'ospedale di Rivoli per accertamenti. I delinquenti hanno anche occupato i binari, interrompendo i collegamenti Italia-Francia e bloccando un treno passeggeri diretto a Torino, con immensi disagi per i viaggiatori, in quanto l'unica via d'accesso al paese era bloccata dai manifestanti e gli autobus navetta non riuscivano a raggiungere i pendolari per portarli a destinazione. I sindaci no TAV si indignano perché non avvertiti in tempo della recinzione dell'area. I lavori dovevano partire a dicembre, oggi siamo ad aprile e mi indigno del fatto che un'amministrazione abbia concesso l'uso della sala polivalente per un'assemblea organizzata dai no TAV. perché è lì che i contestatori hanno pianificato le azioni da compiersi a danno dell'installazione e delle Forze dell'ordine. I dati aggiornati a luglio 2019 vedevano spesi 143 milioni di euro per i sette chilometri di gallerie scavate e 146 milioni di euro (stimati per difetto) per la sicurezza e il ripristino dei danni causati dalle contestazioni. Se non si cambia registro, gli effetti collaterali costeranno ben più dell'opera. Simili comportamenti e atti di violenza non sono più tollerabili, così com'è intollerabile l'atteggiamento di chi governa quei territori, che prende le distanze dagli scontri, si lamenta dell'eccessiva militarizzazione della valle, ma al tempo stesso autorizza e concede locali dove riunirsi a gruppi sfascisti con chiari e dichiarati intenti Voglio concludere questo mio intervento citando il segretario generale provinciale del Sindacato «una cosa è certa: altri dieci anni di queste condizioni dimostrerebbero la fine dello Stato di diritto, incapace di mettere in atto la volontà di ammodernamento delle opere pubbliche senza attivare un perenne massiccio impiego delle Forze dell'ordine». La TAV rischia dunque di diventare l'emblema della debolezza dello Stato, costretto a dispiegare tutte le sue forze per consentire la realizzazione di opere pubbliche moderne e innovative. Una risposta risolutiva sul piano politico e legislativo va data e in fretta, che vada ben oltre l'obsoleta indignazione a cui poi segue un insopportabile nulla di fatto. La ringrazio, Presidente, e dalla parte delle Forze dell'ordine sempre.

lo scorso 9 aprile, a Fabriano, il presidente del consiglio comunale Giuseppina

assurdo e di crisi socio economica globale e totale, che coinvolge il mondo, ha deciso di spostare la propria produzione in Polonia, mettendo sulla strada 410 persone,

Il piano di ristrutturazione annunciato dall'Elica, *leader* mondiale nella produzione di cappe aspiranti, «è inaccettabile. Le lavoratrici e i lavoratori hanno da subito iniziato la mobilitazione e hanno scelto di restare in presidio permanente per protestare contro la decisione del *management* che prevede 409 esuberi su 560 dipendenti, nel comprensorio di Ancona, la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi e l'organizzazione del 70 per cento della produzione in Polonia».

assolutamente la situazione del lavoro in Italia perché è troppo labile e troppe situazioni si creano a causa di aziende che delocalizzano il lavoro all'estero. Non abbiamo più tempo, dobbiamo agire.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento vuole richiamare ancora una volta l'attenzione sulla lotta al cancro, in particolare nell'età infantile e ancora di più dopo il provvedimento che il Senato ha adottato ieri sulla necessità di un nuovo Piano nazionale oncologico. La diagnosi dei tumori nei bambini al tempo del Covid è costellata purtroppo da ritardi e dalle conseguenze problematiche che ciò comporta. Diagnosi, interventi e cure si sono ritardati, in molti centri oncologici, durante la pandemia. Tutto ciò comporta gravi ripercussioni e negativi risvolti sul corretto approccio al bambino con sospetta diagnosi di tumore. Si è ridotto il numero delle diagnosi e degli interventi chirurgici e, d'altronde, molte sedute di chemio e radioterapia sono state rinviate. L'incidenza e il peso della grave situazione che stiamo vivendo, legata alla pandemia, ha stravolto l'organizzazione di molti ospedali e dei centri oncologici, soprattutto nei paesi e nelle Regioni economicamente più deboli, in cui la situazione sanitaria, organizzativa e strutturale pre-pandemia era già molto carente e nelle quali il SARS-CoV-2 ha letteralmente stravolto la debole rete oncologica, la cui sopravvivenza, indispensabile per seguire i tanti piccoli pazienti con patologie neoplastiche nei loro *follow-up*, si reggeva e si regge sui tanti sacrifici e sulla lodevole abnegazione di tanti operatori sanitari. Proprio questi ultimi sono stati spostati e trasferiti nei reparti Covid dedicati, distogliendo una risorsa umana importante nei difficili equilibri esistenti nei reparti di oncologia pediatrica. A tutto ciò si aggiunga che una parte importante delle risorse economiche è stata dirottata verso l'emergenza sanitaria pandemica, con tagli cospicui dei finanziamenti, riduzione dei posti letto e del personale, fino alla chiusura di interi reparti e la loro riconversione in reparti Covid. Come era logico supporre, i paesi e le Regioni a basso reddito pagano ancora una volta il prezzo più alto. La pandemia ha reso più difficile ottenere cure di qualità tutto questo, purtroppo, non sono nel campo della patologia oncologica. La lotta al tumore anche nell'età pediatrica, grazie alla ricerca, è via via costellata di sempre più numerosi successi. Occorrono solo un'attenta programmazione, opportuni investimenti e un'adeguata riorganizzazione della rete oncologica, che vada oltre le problematiche complesse della pandemia. Concludendo, signor Presidente, non dimentichiamo che il binomio tra diagnosi precoce e qualità della terapia è fondamentale per sconfiggere il cancro,

una strage autorizzata dalla ASL. Questo dimostra che la proroga della sospensione delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano, disposta 2021, non è purtroppo una misura sufficiente. Certo, in questo modo è stata risparmiata la vita ed enormi sofferenze a migliaia di cuccioli, circa 35.000, che sarebbero nati proprio ora, nel mese di aprile e in quello di maggio, i quali però, dopo otto o nove mesi di prigionia in anguste gabbie, sarebbero stati uccisi con il gas, il tutto per il solo e ignobile scopo di realizzare delle pellicce. La pelliccia di visone non è necessaria all'uomo, ma è necessaria agli animali. È sconcertante che oggi, in tempi di transizione ecologica, con un nuovo e apposito Ministero, il Governo non prenda in considerazione l'ipotesi di chiudere definitivamente questi allevamenti, come hanno fatto, del resto, in molti Paesi d'Europa. Ne cito alcuni: Regno Unito, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Serbia, Germania, Norvegia, Belgio, Olanda, Svezia e Danimarca hanno sospeso l'allevamento, l'Ungheria ha disposto il divieto di importazione di visoni al fine di evitare la delocalizzazione e, infine, la Francia ha disposto il divieto dal 2026. Occorre tutelare l'ambiente e gli ecosistemi, è necessario porre fine allo sfruttamento degli animali selvatici. L'industria delle pellicce deve definitivamente abbandonare la produzione di questi animali, in favore di materiali sostenibili e ciò non solo per tutelare l'ambiente, ma soprattutto per ragioni di salute pubblica. È probabile che gli allevamenti di visoni siano stati l'origine delle linee virali che hanno diffuso il coronavirus nelle prime ondate. Infatti, Infatti, non sempre negli allevamenti, come ha dimostrato l'associazione animalista LAV, le regole di sicurezza sono state rispettate. La stessa Organizzazione mondiale della sanità ha identificato gli allevamenti di visoni come possibili serbatoi del virus, anche le pericolosissime varianti. Basterebbe che il Ministero della salute obbligasse gli allevatori ai test sierologici. Ecco che allora occorre chiudere questi allevamenti subito, per importantissime ragioni etiche, attesa l'enorme sofferenza inferta ai bellissimi e poveri animali. Concludo, Presidente, con l'auspicio che il Governo intervenga immediatamente sia per la tutela degli animali, ma soprattutto per la tutela della salute pubblica.